nostro esame consente ora non soltanto di discutere sulle importanti misure in esso contenute, ma soprattutto di fare un bilancio complessivo sulle politiche economiche e di finanza pubblica degli ultimi cinque anni e sull'eredità - a nostro giudizio positiva - che lasciamo al prossimo Governo. Il nostro Paese si trova oggi in una situazione di conti pubblici in ordine, che continuerà anche nei prossimi anni, e con un'economia in decisa ripresa. In breve, siamo nelle condizioni di guardare finalmente al futuro con maggiore fiducia e con la consapevolezza di poter migliorare ulteriormente i nostri fondamentali. fondamentali. Il quadro è completamente diverso da quello da noi ereditato a inizio legislatura, che ci ha visto duramente impegnati nel corso di questi anni per capovolgere in positivo la situazione. Il quadro economico e di finanza pubblica di inizio legislatura

In tale contesto, pur impegnando 15 milioni solo per la manovra, non era pensabile permettere l'innalzamento dell'IVA, che avrebbe sicuramente ucciso i pochi elementi di ripresa e i chiari segnali presenti. Nella manovra si sta attenti alla crescita e allo sviluppo. Si danno incentivi affinché il mondo delle imprese si riprenda. Si danno incentivi per aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro. previste misure che partono dalla prima infanzia per arrivare fino all'ingresso nel mondo del lavoro. Il lavoro del Senato è stato importante e strategico. Abbiamo preso in mano una legge di bilancio già buona e utilizzato tutti gli spazi possibili per inserire

Ritorno ora a parlare degli elementi di politica e di economia e finanza. Negli ultimi quattro anni la politica economica e finanziaria messa in atto dal Governo ha dovuto procedere all'interno di un sentiero stretto - per usare un'espressione così soventemente ripresa dal ministro Padoan - spesso concordato con l'Unione europea, i cui confini risultano compressi - da un lato - dagli effetti di una crisi economica senza precedenti nella storia recente e - dall'altro - dall'esigenza di riduzione del disavanzo e del debito pubblico. Il provvedimento - come già accennato - focalizza gli interventi prioritari su alcune direttrici: in primo luogo, le misure volte a realizzare le clausole di salvaguardia su IVA e accise, che cubano per ben 15 miliardi; le riforme e le diverse *policy* approvate negli ultimi anni hanno ridotto ulteriormente il differenziale dell'Italia rispetto alla media dell'Unione europea hanno restituito credibilità al nostro Paese. E il disegno di legge di bilancio al nostro esame si inserisce in tale contesto con l'obiettivo di continuare a innalzare il potenziale di crescita dell'economia nazionale, l'occupazione e le capacità innovative e competitive delle imprese. Al prossimo Governo spetterà, pertanto, il compito di non disperdere i risultati raggiunti e di proseguire nel percorso delineato in questa legislatura.

Credo si possa tranquillamente pensare a una legge di bilancio rivolta allo sviluppo e alla crescita. Ora le misure ci sono tutte. I segnali di crescita sono presenti e spetta a noi fare in modo che si prosegua su questa strada.

ci hanno fatto ampiamente discutere in questi giorni e ci hanno fatto pensare a cosa è meglio per il nostro Paese, pur nelle diversità pur nelle diversità delle posizioni. Si è lavorato davvero tanto insieme, anche con le opposizioni, in un clima complessivamente costruttivo, tant'è vero che molti degli emendamenti di sintesi che, come relatori, abbiamo prodotto sono stati approvati all'unanimità. E questo perché molti temi erano sentiti da tutti i Gruppi e, quindi, la sintesi ha cercato di tener conto di tutte le esigenze e differenze.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, questa notte in 5a Commissione si è concluso l'esame del disegno di legge per il 2018. I lavori si sono svolti in un clima di buona collaborazione, consci tutti (maggioranza e minoranza al Senato, così come il Governo) delle ricadute delle nostre scelte e delle decisioni che stiamo prendendo. Dopo settimane di intenso lavoro giungiamo nell'Aula del Senato con l'ultima legge di bilancio di una legislatura estremamente delicata, per le particolari condizioni economiche e politiche del nostro Paese, in uno scenario nazionale e internazionale in costante e continua mutazione. La manovra di finanza pubblica per l'anno 2018 si sviluppa in un quadro di ripresa economica e occupazionale. Chiaramente, non tutti i dati macroeconomici e le stime numeriche sono positivi, ma la costante che ha caratterizzato l'azione governativa e della maggioranza in Parlamento è stata quella di mettere in campo azioni efficaci e volte al miglioramento della politica del nostro Paese. Pertanto, nel giorno in cui l'ISTAT certifica il crollo - ahimè - delle nascite nel nostro Paese, il *bonus* bebè diventa una misura strutturale. Mi piace sottolineare come la Commissione bilancio abbia votato all'unanimità l'emendamento in questione, a dimostrazione del fatto che la famiglia e il sostegno alla genitorialità Siamo tutti chiaramente consapevoli dell'esiguità delle risorse a disposizione per il prossimo triennio e in particolare per il prossimo anno. Questo, non farà sicuramente venir meno l'impegno ad ampliare le misure approvate in tema di famiglia. L'adeguamento delle soglie reddituali per le detrazioni per i figli a carico sembra essere una necessità rilevante e speriamo che questo innalzamento possa essere introdotto alla Camera. La mia collega poco fa è intervenuta su tantissimi temi. Io vorrei sottolineare che sono stati fatti grandi interventi, nei campi pensionistico, della famiglia,

grandi interventi e azioni mirate. Ringrazio fortemente anche gli Uffici, riscontrandone l'alto senso del dovere

il disegno di legge comprende di tutto, fuorché ciò che possa essere pertinente al significato della legge stessa, e racchiude al suo interno una serie di favori

quando a un certo punto, nell'interregionalità, non sono stati presi in considerazione la volontà e il parere degli enti locali, dei sindaci, degli amministratori, delle associazioni di categoria del mondo dell'agricoltura e della pesca e di quanti altri avrebbero avuto titolo - e in effetti hanno titolo - a esprimere un parere.

piaccia o no, dipende da ciò che mangiamo e da come mangiamo, ma soprattutto da ciò che mangiamo. Il mondo dell'agricoltura è un settore primario e va difeso. Non posso accettare che sia respinto un emendamento che chiede l'innalzamento dell'età per accedere a facilitazione e sgravi contributivi a favore

cercare di fare beceri risparmi a vantaggio di pochi e non di chi veramente ha bisogno di lavorare, creare impresa e credere in questo settore, checché se ne dica del *made in Italy* di cui molti si riempiono la bocca. Faccio parte della Commissione agricoltura e tante volte

nulla si è fatto per le gravi situazioni che investono ormai da troppi anni il mondo dell'agricoltura.

come l'agricoltura sia un settore che riguarda tutti. Dobbiamo essere competitivi per poter valorizzare quello che tanto viene decantato come *made in Italy*.

o dello stabilimento di produzione, così definito in un gergo un po' maldestro. Dobbiamo garantire chi produce

che c'è ripresa non più timida del PIL e, tutti sono soddisfatti; abbiamo gli 80 euro e tutta una serie di manovre che ci stanno accompagnando in maniera serena verso le prossime elezioni. Ovviamente non è così, perché sappiamo che questo è semplicemente un ciclo

del nostro anno politico, venga discussa in siffatto modo. Noi abbiamo avuto sessioni della Commissione bilancio che si sono protratte fino alla mattina, in condizioni di lavoro estreme, e ciò determina soltanto un fatto:

nella condizione di poter svolgere un dibattito politico all'interno dei palazzi, senza costringere e comprimere il dibattito in maniera repressiva.

nelle convenzioni tra Regioni, enti locali e protezione civile, ospitalità sociale. Cosa significa? Che molte attività ricettive hanno ospitato cittadini purtroppo sfollati a causa del terremoto

intervengo non tanto per criticare questa legge di bilancio, che è, né più, né meno, una serie di piccoli interventi dettati dall'imminenza del momento elettorale. Si tratta di piccole mance, ma anche di interventi che incidono sulla stessa funzionalità del sistema del nostro Paese.

responsabilità di garantire che il processo democratico di legislazione avvenga secondo determinate regole. Le confesso avevo molta fiducia nel fatto che fosse lei a seguire la legge di bilancio, insieme al presidente Tonini. L'articolo 80, che è stato approvato e che era inserito nella legge di bilancio,

a settant'anni l'età della pensione dei magistrati, ha pensato di dare un contentino, non preoccupandosi di risolvere il problema della sezione tributaria della Corte di cassazione. Avete sentito dire tutti in quest'Aula che la sezione tributaria della Corte di cassazione è gravata non solo da un enorme arretrato, ma anche da un afflusso di ricorsi ogni anno che sono pari a un terzo dell'intero ammontare dei ricorsi che arrivano presso la Corte di cassazione. Ebbene,

che voleva significare: istituiamo per legge la sezione tributaria presso la Corte di cassazione e consentiamole di operare con un numero di magistrati idoneo.

sono profili d'incostituzionalità? La nostra Costituzione prevede la possibilità di nominare magistrati onorari per la funzione di giudici singoli.

non può determinare quel numero di magistrati che soltanto quella modifica avrebbe potuto invece garantire nel numero di 45. Questo avrebbe significato la seria

e dunque viene meno la funzione di nomofilachia.

non si può toccare una cosa che è stata fatta, non si comprende perché. Vi rendete conto che per tre anni si utilizzano i magistrati che vanno in pensione e che dovrebbero risolvere i problemi? Come si utilizzano i magistrati che vanno in pensione? Nominandoli magistrati onorari. Vi rendete conto? Si forza una norma della Costituzione e si tenta di farsi perdonare

Signor Vice Ministro, io credo che il lavoro del Parlamento non possa essere ridotto ad un mercanteggiamento determinato da da chi ha più influenza per ottenere una determinata normetta o articolo. Il problema di fondo è che noi dobbiamo renderci conto che quando si chiede il parere ad una Commissione tecnica di questo Parlamento, occorre poi avere la forza, la possibilità, il dovere giuridico e politico di rispondere in Parlamento e di spiegare le ragioni che portano a discostarsi da un parere dato all'unanimità che solleva da un lato dubbi di costituzionalità e dall'altro di funzionalità del sistema, suggerendo di adottare un determinato emendamento. So che non

non posso che ripetere quanto scritto in quel rapporto. Si è in presenza di un tripudio di fondi rifinanziati, riprogrammati, definanziati o addirittura soppressi. Si disperdono le risorse in una miriade di piccoli interventi con effetti molto limitati, rispondenti a molteplici obiettivi, ignorando le vere priorità e utilizzando la flessibilità dell'Unione europea per sterilizzare il meccanismo delle clausole IVA e aumentare il *deficit* e la spesa corrente, senza riuscire a far ripartire gli investimenti pubblici, leva fondamentale per creare crescita, sviluppo e buona occupazione, scesi in valore del 4 Si sono votate norme "manifesto" perché le elezioni si avvicinano. E quindi sbandierare provvedimenti rende. Forse. Ma credo, sono convinto che questa volta avete fatto i conti sbagliati. Non voglio nemmeno rimarcare come, una parte politica ben nota in questa Aula, abbia condizionato diverse decisioni per affermare una propria primazia su una serie di stanziamenti, grazie anche ad un esplicito ricatto politico a cui la maggioranza non si è opposta, anzi! Mi preme però rimarcare che il Movimento 5 Stelle, come fa dall'inizio di questa avventura in Parlamento, ha proposto una serie di idee per risolvere problemi reali, ed anche in questa legge di bilancio è rimasto inascoltato. Ognuno di noi, nel proprio campo di azione, ha proposto soluzioni utili alla collettività e con lo scopo di mirare al bene comune. Ad esempio, per quel che mi riguarda ho tentato di esentare dalla restituzione di quanto percepito, a titolo di benefici pensionistici previsti per i lavoratori esposti all'amianto, i soggetti per i quali sia stata riconosciuta, seppure solo nei gradi di merito del processo, l'esposizione all'amianto. Costava un milione di euro ed avete detto no. Ma nel contempo avete trovato 10, 100 volte tanto per localistiche, mirate e redditizie (l'espressione è dovuta) "marchette". Così come, tramite il credito di imposta si è provato a facilitare la bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto nei locali pubblici e aperti al pubblico, puntavamo alla progressiva sostituzione dei materiali in amianto con altri prodotti di uso equivalente. Molto si è proposto sulla mobilità sostenibile a partire dal sostegno al ciclo turismo per proseguire la realizzazione del Corridoio verde adriatico nella regione Abruzzo per il recupero e la riqualificazione ad uso ciclo pedonale dei tracciati già esistenti e per la realizzazione degli interventi necessari nei Comuni interessati così come si è provato ad incentivare, tramite erogazione di contributi a fondo perduto, l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita. Tramite concessione di finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che operano nei settori della *green* *economy* e della ricerca nel campo delle *smart cities* credevamo di trovare il vostro sostegno ad una azione utile a dare forza alla occupazione, problema principale del nostro Paese. Anche qui: picche! Al fine di favorire gli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale e di promuovere il concorso dello Stato al raggiungimento degli *standard* europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale si è tentato di aumentare la dotazione del fondo per l'acquisto di veicoli adibiti al miglioramento dei servizi offerti offerti per il trasporto pubblico locale. Poi bonifica isochimica, Bussi sul Tirino, fondo per le ciclovie turistiche, aiuti ai piccoli Comuni tramite aliquote IVA agevolate, credito imposta per imprese e coltivatori, agevolazioni gasolio e gpl, incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tutto respinto! Nessuna soluzione alternativa, diversa proposta dalla maggioranza. Nulla. Per principio al Movimento 5 Stelle si deve dire no! E così anche questa volta, verrà vanificata l'azione che una vera legge di bilancio potrebbe avere se affrontata con criteri diversi e con una visione di Paese che non sia legata solo ed esclusivamente all'immediato ritorno elettorale. Tutto questo è stato reputato inutile. Viene rabbia! Non perché la non approvazione di alcune di queste proposte provenga da una scelta politica; in quel caso avrei accettato; non compreso ma accettato. Avete fatto scelte quanto meno discutibili. La *ratio* del piano Industria 4.0, voluto e rivendicato a più riprese dal Ministro dello sviluppo economico, era tanto chiara quanto semplice: costruire due pilastri, gli

poco o nulla si è mosso. La concentrazione pressoché totale del piano nazionale Industria 4.0 del Governo italiano sulla produzione manifatturiera e sulla fabbrica non è positiva in un momento storico nel quale, proprio grazie all'Internet delle cose, industria e servizi sono sempre più interconnessi tra loro dando origine a modelli di *business*, mercati, processi, prodotti e dinamiche del consumo, non solo nuovi ma anche integrati. La tecnologia ha inciso profondamente anche nelle modalità di guardare al mondo dei viaggi, ampliando a dismisura la possibilità di reperire informazioni, rivoluzionando il tradizionale concetto di intermediazione e riducendo di conseguenza l'asimmetria informativa tra produttore e consumatore. Occorreva indirizzare e qualificare maggiormente le risorse da impegnare nel settore del turismo per supportare la crescita della dimensione digitale, ormai inarrestabile. Se le opportunità di questa nuova sfida non dovessero essere colte, gli effetti negativi prodotti dalla diffusione dell'automazione e delle nuove tecnologie

di buon senso sono state affossate per accontentare interventi localistici. Ma tant'è e forse, anzi sicuramente, questo è il motivo per cui tanti cittadini come noi hanno deciso di venire con l'obiettivo di sostituirvi il più presto possibile.

alla discussione e al varo della legge di stabilità oggi al nostro esame. Non ragionando mai infatti all'insegna del tanto peggio, tanto meglio, abbiamo cercato con proposte puntuali, concrete, motivate e con tanto di coperture, di richiamare l'attenzione su una serie di temi.

dei giornali leggo oggi notizie riguardanti l'andamento della natalità in Italia. Ci sono dati allarmanti; diminuisce, come da tempo avviene, il numero delle nascite,

che incidono sul tasso di natalità. Ebbene, noi, a fronte di queste notizie, leggiamo sui giornali di queste ore, da un lato, i dati demografici ISTAT e, dall'altro, l'annuncio che il *bonus* bebè

altro che coperture! Ci sono le stracoperture per la famiglia, il *bonus* bebè e la natalità; è che non ve ne importa niente di queste cose e le avete tagliate.

lo dico anche a chi ci dovesse seguire fuori di qua - dimezza il *bonus* bebè dal 2019, mentre non si dimezzano ma si riducono considerevolmente le nascite. Non c'è un rapporto di causa ed effetto, ma un andamento del Paese che dovrebbe comportare politiche abitative, fiscali e sociali invece, non l'avete fatto. emendamento - voglio dare atto alla collega Bignami di aver avuto grande tenacia nel perseguire questa causa trovando ampio consenso - però non possiamo non dire che la cifra è esigua. Si apre un capitolo

Noi, come al solito (lo sa il vice ministro Morando con il quale su questo tema ci confrontiamo da tempo), avevamo sottolineato l'esigenza della sicurezza.

delle Forze di polizia, che forse potranno disporre - si spera se non verranno fatti trucchi contabili in qualche ufficio di Governo - di una cifra residua nel 2017 e 2018 per un parziale pagamento degli straordinari.

Fate in modo che da qui al 31 dicembre qualcosa ci rimanga. Vorrei che rimanesse al verbale. Non vorrei che da qui al 31 dicembre quel capitolo venga prosciugato così nel rinvio di quelle cifre al 2018 per gli straordinari non resti niente. In questa legge avevamo proposto uno stanziamento per il comparto sicurezza e difesa

perché anche adesso che si avvicina il Natale c'è il Piano sicurezza delle città e dei mercatini di Natale. Certo, sono belli, ma oggi girano in Europa persone che li considerano un bersaglio. Insomma, c'è una esigenza di sicurezza che cresce: esigenza militare e di forze di polizia. Noi abbiamo proposto di fare questo stanziamento. Come lo si copre? Noi lo abbiamo indicato in maniera dettagliata. Sono molti i tagli e quant'altro a spese produttive. Ricordo che noi spendiamo cinque miliardi per l'immigrazione quest'anno. Invece, per il contratto delle forze di polizia, niente. Il blocco contrattuale è antico; lo so che vari Governi di ogni orientamento ne sono colpevoli, ma c'è stata una sentenza della Corte Il comparto sicurezza e difesa, grazie a una legge voluta dal Governo Berlusconi, ha la sua specificità in quanto svolge un lavoro rischioso e pericoloso, che viene considerata una specificità all'interno del pubblico impiego. Ma dov'è il contratto?

1,2 miliardi sono troppi (5 miliardi agli immigrati sì, ma al comparto sicurezza e difesa no), bene, stanziamo 200 milioni. E la cifra non l'abbiamo inventata, ma l'abbiamo letta anche sui giornali. Il «Corriere della sera» giorni fa, raccogliendo il grido di allarme di alti esponenti di forze di polizia aveva quantificato questa lamentazione pubblica di alti esponenti, non della politica, ma delle forze di polizia, definendo in 200 milioni le esigenze minime:

dove si concede, tipo per l'assistenza familiare alle persone con disabilità, si parla di 7 euro per ogni caso. Sulla famiglia e sulla sicurezza questa legge di stabilità non solo delude ma non dà risposte.

la data, ma la legislatura comunque volge a termine. E voi sarete bocciati dal vostro fallimento, dalla vostra arroganza, dalla vostra incapacità e dalla vostra disattenzione a temi di prioritaria importanza. Su famiglia e sicurezza vi chiameremo a rispondere, non tanto in quest'Aula dove vi blinderete con l'ennesima fiducia, ma davanti al Paese che quella fiducia non ve la darà.

Li saluto a nome della Presidenza e di tutti i senatori e faccio loro i complimenti perché sono ragazzi che hanno raggiunto risultati di eccellenza nei loro studi e che sicuramente avranno un ruolo importante in futuro. Benvenuti in Senato e molti auguri a tutti voi.

rese evidenti durante i lavori di Commissione, e restituisce al Paese un quadro con molte ombre e poche luci, una istantanea di una legislatura caratterizzata troppo spesso da ostentati "vorrei ma non posso", da false promesse o da promesse mantenute che spesso sanno di *spot* elettorale. Il lavoro della Commissione bilancio ha certamente corretto il tiro di un provvedimento per molti versi deludente. Ci si aspettava qualcosa in più: il Paese attendeva misure più incisive, strutturali, concrete e definitive. Si è preferito invece, ancora una volta, intervenire per limitare i danni e non scontentare nessuno. Questa, almeno, è la sensazione che in tanti - in troppi - abbiamo avuto. È mancata quindi, anche in questo caso, una visione strategica e d'insieme, una visione capace cioè di fornire risposte adeguate alle istanze del Paese e dei ceti meno privilegiati. Anche questa volta ha pesato, e non poco, l'invito formulato dalla Commissione europea ad evitare passi indietro sul fronte delle riforme strutturali, in particolare su quella pensionistica. Passando alle misure che noi componenti del Gruppo Misto-Fare! abbiamo proposto, spiace dover segnalare, tra le altre cose, che non si sia voluta trovare una soluzione per la proroga del cosiddetto meccanismo "opzione donna". Come tutti noi ben sappiamo, si tratta di donne chiamate a confrontarsi con una quotidianità tutt'altro che agevole e che, con encomiabile abnegazione e determinazione, sopperiscono spesso - possiamo dire sempre - a carenze del nostro sistema socio-assistenziale. Invito pertanto il Governo, anche in questa sede, ad attivarsi per dare una risposta concreta su una tematica tanto delicata

è stata invece data ai risparmiatori, che si sono visti sottrarre i loro beni all'interno di un sistema che, alla luce anche del lavoro che la Commissione di inchiesta sul sistema bancario sta svolgendo, li ha resi vittime. Si è trattato di un atto dovuto, a parziale ristoro del trattamento riservato da quelle banche a correntisti e azionisti. Grazie alla collaborazione tra le diverse forze politiche - dobbiamo darne atto - e all'interazione sulla questione si è riusciti a dare una prima risposta.

L'istituzione di un fondo per i risparmiatori, a nostro avviso, è solo un timido primo passo, ma l'aspetto dinamico della norma ci porta nella giusta direzione e auspichiamo che questo sia davvero il punto di partenza, per dare di nuovo fiato ai risparmiatori, alle famiglie, ai pensionati e a tutti coloro che hanno creduto ad un sistema che, invece, li ha portati alla rovina e, a volte, purtroppo, anche alla scelta definitiva del suicidio. Quindi davvero ci sentiamo responsabili per un sistema fallimentare, che

Gli enti locali, molti in situazioni economiche problematiche, in questi anni hanno visto decrescere in modo allarmante le loro capacità programmatiche. Particolare attenzione - e su questo mi permetto di sollecitare un intervento del Governo nel passaggio del provvedimento alla Camera

Nella direzione auspicata va anche la modifica approvata, relativa all'ulteriore semplificazione del documento unico di programmazione per Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Noi alla Camera continueremo a sostenere le loro giuste istanze, al pari di quanto certamente faremo per tutti gli altri temi che purtroppo in Senato non hanno trovato risposta. Mi sia consentito, signora Presidente, esprimere la mia personale soddisfazione e quella del Gruppo Fare! per

La strage del Vajont non è solo una questione veneta o bellunese, ma riguarda l'Italia tutta intera. È giusto quindi che in questo disegno di legge di bilancio si siano finalmente trovate delle risorse da destinare a quello che, con decreto del Presidente della Repubblica del 2 ottobre 2003, è stato dichiarato monumento nazionale.

di un Esecutivo impegnati a dare risposte e trovare soluzioni, mettendo da parte inutili quanto stucchevoli personalismi e anteporre l'interesse del Paese ad ambizioni e ingiustificabili smanie di *leadership*.

che vi vorrei parlare, perché in questo momento c'è un duplicato: il segnale che arriva da quest'Aula viene infatti trasmesso simultaneamente sia su Radio Radicale che su Rai GrParlamento. Questo avviene - è giusto che tutti i cittadini lo sappiano - con soldi pubblici:

dal canone, non è in grado di assicurare una copertura totale. Noi allora facciamo un duplicato: diamo a una radio privata, che poi è una radio di partito - tra l'altro,

trasmettere sul digitale terrestre i due segnali di Camera e Senato, in modo che da casa qualsiasi persona di qualsiasi età che non avesse accesso o dimestichezza con Internet e con i canali satellitari

Cosa vuol dire? Oggi c'è la prima versione del digitale terrestre, ossia il DVB-T1. Accadrà che chi trasmette dovrà cambiare modulazione e trasmettere con il segnale DVB-T2. Ma a casa,

DVB-T2. Accade che questo Governo ha deciso di fare un doppio passaggio: per un anno o un anno e mezzo passeranno al sistema DVB-T2 prima le locali, e poi con calma seguiranno le nazionali. Ovviamente accadrà che chi non ha il ricevitore digitale terrestre DVB-T2 a casa, praticamente quasi tutti, di colpo non vedrà più le locali.

accorge che il mondo va in un'altra direzione: sarà tutto in digitale e tra un po' la televisione, così come la conosciamo, non ci sarà più. Lo stesso dicasi per il DAB. C'è quest'altro inganno sulla radio digitale, ne avrete sentito parlare: che bella la radio digitale, il futuro e il cosiddetto DAB+. Però sono

può tenersi le frequenze sperimentali; in quelle zone dove non è ancora stata assegnata la frequenza del digitale radiofonico, non può trasmettere nessun altro. Quindi, oggi la sperimentazione può essere fatta solo dai grandi *network* e in quelle zone (si tratta di tante Regioni, che coprono circa la metà dell'Italia) dove il Ministero non ha assegnato le frequenze non si possono

In ultimo, apprezziamo l'approvazione di un ordine del giorno che riguarda le persone affette da obesità.

Questo ordine del giorno, quindi, impegna il Governo a reperire le risorse necessarie per garantire la mobilità e l'accessibilità delle persone affette da questa problematica. Per questo ringrazio tutte le associazioni che ci hanno segnalato il problema e le persone che l'hanno raccontato, come Fabio De Nunzio e Vittorio Graziosi. Signora Presidente, ci troviamo ad affrontare l'ultima legge di bilancio di questa legislatura ma, in realtà, l'ultima legge di bilancio di un lungo periodo, caratterizzato dal Governo del Partito Democratico, iniziato alla fine del 2011, con l'arrivo, inaspettato e anche un po' discutibile, di un Governo pseudotecnico, quello di Monti, proseguito poi con i Governi PD Credo quindi sia il momento di fare dei bilanci sull'efficacia dell'azione di questi Governi e di questa forza politica, che - ormai è evidente - è in caduta libera agli occhi degli italiani, come dimostrano le recenti elezioni elezioni che si sono tenute in Sicilia. Credo sia evidente a tutti che la situazione che ci troviamo ad affrontare è ben più grave rispetto a quella che vivevamo sei anni fa. Ci troviamo in una situazione in cui molte imprese e molte attività economiche sono fallite, in cui vi è stato un aggravio della pressione fiscale (soprattutto sotto il Governo Monti), che ha messo in ginocchio il Paese invece di risollevarlo. È una situazione in cui ormai i cittadini non hanno più fiducia nelle istituzioni e hanno perso tutte le proprie certezze, in termini di sicurezza, ma soprattutto rispetto al futuro, al lavoro, alla possibilità di avere una speranza di migliorare le proprie condizioni di vita, e hanno perso perfino la certezza di poter considerare al sicuro i propri risparmi e di avere una pensione dignitosa una volta terminata la propria vita lavorativa.

una manovra snella; credo, invece, che ci troviamo ad affrontare una manovra assolutamente inconsistente, più che snella. Infatti, l'unica risposta reale che dà è quella di rinviare l'applicazione delle clausole di salvaguardia, cioè un aumento della pressione fiscale, soprattutto per quanto riguarda l'IVA;

È una continua rincorsa nel tentativo di non applicare queste scellerate tasse e questi scellerati aumenti sull'IVA e sulla benzina, che potrebbero deprimere ulteriormente la nostra economia, prima o poi, si troverà ad affrontare. Non vorremmo che questo rinvio fosse solo funzionale al fatto che, magari nella prossima legislatura, a causa di prese di posizione più severe da parte della Commissione europea, un Governo, magari di unità nazionale

da parte del Governo, l'azzeramento di queste sciagurate misure, non certamente un rinvio. Siete stati bocciati anche dalla Commissione europea, sempre, però, con un un rinvio di decisioni, che dovranno essere prese in primavera dal prossimo Governo, magari con richieste di nuove manovre, stimate nell'ordine di 5 miliardi di euro, quindi manovre serie. Avete poi imbastito, a parte questo rinvio di aumento di tasse, una legge di bilancio che cerca di affrontare, a *spot*, alcuni temi veri e reali,

non possiamo ridurci a ritenere che l'unica cifra rilevante per considerare il vostro successo sia l'aumento del prodotto interno lordo. Si tratta di un aumento irrisorio rispetto alla media europea, è quasi un effetto trascinamento: non siete stati voi a

Non è la politica dei *bonus*, quella tanto cara a Matteo Renzi, che può creare sviluppo. Queste sono politiche assolutamente fallimentari e ne è dimostrazione la sofferenza che c'è ancora nel nostro Paese. Si può cercare di tenerla nascosta in quest'Aula, ma è evidente per chi per chi frequenta le nostre città e le nostre comunità. Ci sono ancora un vastissimo malessere, rabbia e assenza di speranza nel futuro: questi sono i mali reali del Paese, che voi non avete aggredito. E non sarà certo il *bonus* bebè, con quegli 80 euro per un anno - che poi diventano 40 nei successivi - a creare prospettive di crescita dei nuclei familiari. C'è il tema degli asili che dev'essere affrontato: si pagano rette altissime, che devono essere azzerate. La frequentazione degli asili deve essere considerata un diritto dei cittadini, al pari della scuola dell'obbligo; questo sarebbe un salto di qualità nella cultura italiana. Certamente anche la riduzione dei *superticket* imposta dallo Stato e dai Governi negli anni passati è assolutamente irrisoria. È una cifra simbolica quella che viene stanziata, anche qui nel tentativo illusorio di dimostrare ai cittadini che si danno risposte.

sono poi temi anche di altro carattere, e mi riferisco al vostro approccio all'autonomia dei nostri territori. Dopo ripetute manovre, che hanno ridotto in termini insostenibili i trasferimenti agli enti locali, Comuni, Province e Regioni che sono quelli che erogano effettivamente i servizi quotidiani che stanno a cuore ai cittadini, perché non siete riusciti a tagliare la spesa pubblica statale; cosa che non avete mai voluto,

strade e i servizi sociali), dopo tutte queste manovre continuate dunque nella politica di riduzione degli spazi di autonomia. Non solo ci avete provato con il *referendum* dell'anno scorso, quello del 4 dicembre, che ha mandato a casa Matteo Renzi,

di un parco, quello del Delta del Po, interregionale e nazionale, ignorando totalmente le richieste, non solo della Regione, dei territori e delle Province, ma anche dei Comuni, delle associazioni dei cittadini e di chi lavora e ha bisogno di

che non si fidano più dei Governi centrali, che vogliono e pretendono di gestire competenze e risorse sui propri territori, e andate avanti per la vostra strada. Ma la strada per voi è chiusa, è finita, siete al capolinea,

C'è poi un'ultima norma che è un insulto, un'offesa a decine di migliaia di risparmiatori che sono stati truffati dalle banche, dal Governo, da questo Paese, che avevano fiducia in un futuro dignitoso, nel tentativo di mettere da parte il frutto del proprio lavoro in alcuni istituti bancari.

tra l'altro difficile da ottenere, perché ci vorrà un decreto del Governo per stabilire i criteri, i requisiti, le modalità e le condizioni per accedere a questo fondo,

che questi risarcimenti avverranno solo in seguito a sentenze passate in giudicato, sostanzialmente quindi con l'obbligo per questi risparmiatori truffati di fare causa alle banche, con un percorso difficile, complicato, impossibile. Questa è l'ultima - ennesima - vergogna di questo Governo, che invece di dare risposte al Paese ha vissuto di *bonus*, di promesse, di inganni, di comunicazioni che sono state assolutamente non veritiere. Ma, guardate i cittadini si ricorderanno di quest'esperienza, di questi sei anni di malgoverno, di bugie, di illusioni. Il tempo per voi è scaduto - o scadrà presto - e mi auguro che il prossimo Governo punti su uno sviluppo che dia certezze alle nostre famiglie, e certezza di un futuro migliore per quei giovani italiani che vogliono ancora costruirsi un futuro in Italia, nei nostri territori, e non essere costretti a emigrare, la più grande vergogna che abbiamo vissuto negli ultimi anni. signor rappresentante del Governo, colleghi, la legge di bilancio stabilisce le priorità di un Governo, di una maggioranza, di un soggetto politico rispetto alle spese del Paese.

ma la legge di bilancio stabilisce per l'appunto le priorità e le quantità. È una bella cosa che siano stati toccati questi due argomenti, ma quando si parla di soldi, c'è poco da fare, evidentemente il punto è la quantità.

l'accoglienza immediata degli immigrati. I 600.000 immigrati che con grande determinazione l'attuale Governo e quello precedente hanno voluto portare in Italia in ogni modo, fatto, come detto pochissimi giorni fa dal presidente del Consiglio Gentiloni Silveri, che l'Italia è l'unico Paese ad avere una politica decente sull'immigrazione. Ciò nel suo pensiero significa una politica di vasta accoglienza. Nessun altro Paese in Europa lo fa, noi lo facciamo.

Parlando del beneficio per la singola famiglia, sappiamo che al di sopra di un reddito non certo stellare, una famiglia italiana ha zero benefici per un figlio a carico, o meglio può avere una detrazione di circa 600 euro l'anno, pari a circa 50 euro al mese,

senza contare i circa 200 euro al mese che costa l'assistenza sanitaria per ogni residente in Italia, sia italiano che stranieri e gli stranieri si ammalano tanto quanto noi;

nostre scuole. Ogni bambino che va a scuola, italiano o straniero, costa allo Stato circa 700 euro al mese, ivi inclusi i mesi estivi. Quindi, senza contare questo, per ogni immigrato si trovano più di 1.000 euro al mese, per ogni famiglia con bambino, forse, quando va bene, 140 euro, nei casi medi intorno ai 50 euro, in molti casi zero assoluto. Questo ci dice che evidentemente le priorità che si danno sono diverse da quelle che credo la maggior parte degli italiani vorrebbe. Come già detto, proprio in questi giorni, perché è un tema di attualità (e teniamo presente che la legge di bilancio dura un anno), l'Istat ha

La questione dei *caregiver* è giustissima. Nel medio termine - e forse addirittura - nel breve può essere un risparmio per lo Stato, se è uno stimolo vero per le famiglie a

in tre anni: 20 milioni di euro all'anno. Qualcuno - spero - abbondando un po' nelle cifre ha detto che le persone che dovrebbero fruire di questa assistenza, ovvero le loro famiglie, sono 3 milioni; il che farebbe la bellezza di sette euro all'anno, che non credo cambi la situazione neanche nelle famiglie però già un segnale positivo, anche se rimane solo tale. Noi troviamo appena 20 milioni di euro per le famiglie che si prendono cura in casa delle persone non autosufficienti e che hanno bisogno di assistenza continua

che il gruppo internazionale specializzato in questo settore ritiene a grave rischio, perché sono Paesi inaffidabili o aggressivi verso i loro vicini. Ci sono Paesi minori, ma tutti sanno che il centro di questo provvedimento è l'Iran. Tre giorni fa il vice capo dei pasdaran, che sono il vero regime in Iran, ha dichiarato

Meno di 2.200 chilometri dall'Iran alla Puglia, meno di 2.600 dall'Iran a Roma, meno di

come centrodestra, dobbiamo prenderci l'impegno di cambiare radicalmente nella prossima legislatura dopo le elezioni.

(circa 14.600 persone e quindici categorie; si va dal lavoro siderurgico a quello edile, agli insegnanti della scuola d'infanzia, ad altre categorie) ad altre categorie) il principio che non tutti i lavori sono uguali di fronte alla pensione, come giustamente ha stabilito un accordo tra due organizzazioni sindacali e il Governo. L'*iter* parlamentare è stato molto rispettoso della dialettica tra Governo e parti sociali: si è stabilito davvero un circolo virtuoso tra Governo, Parlamento e parti sociali. Quindi, si sostengono

si decide anche un principio fondamentale: la portabilità dell'esonero contributivo, che apre la strada a un principio importante, come dicevo; nello stesso tempo, si aiutano le persone ad andare in pensione derogando all'automatismo dell'aspettativa di vita. Si tratta di una legge di bilancio in cui la maggior parte delle risorse, come anche miei colleghi esponenti dell'esposizione

giovani e persone accompagnate alla pensione sono sicuramente misure per la crescita, l'occupazione e lo sviluppo del nostro Paese. Sempre in tema lavoro, sono particolarmente contenta di un emendamento approvato in Commissione bilancio che riguarda risorse ad ANPAL Servizi SpA, strettamente collegate all'assegno di ricollocazione, altro diritto fondamentale, importante e nuovo nel panorama giuridico italiano: accompagnare e aiutare le persone a ritrovare il lavoro quando lo perdono. Altrettanto importanti sono le risorse destinate all'INAPP, l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche. Noi abbiamo tanto bisogno di monitorare e capire come impattano le leggi per costruire Sempre nella dinamica parlamentare si è dato spazio anche a risorse per il sistema duale e l'incontro tra scuola e lavoro, di cui abbiamo tanto bisogno, perché è la vera politica del lavoro: sostenere le competenze dei nostri giovani, soprattutto anche competenze digitali, come qualcuno ricordava. Inoltre, sulle politiche sociali è la prima volta che - dal 1° luglio di quest'anno - la legge di bilancio prevede un ulteriore rafforzamento del contrasto alla povertà:

Abbiamo rafforzato, anche nel corso dell'*iter* parlamentare, le risorse ai servizi territoriali per consentire di attuare e gestire questa riforma.

dopo che c'è stata, appunto, una dialettica positiva tra maggioranza e opposizione sul tema. Stabiliamo un fondo per dare sollievo a queste persone, a queste figure, che spesso non hanno neanche il tempo di fare una passeggiata, perché si dedicano

il sistema dei servizi socioassistenziali, capire i loro bisogni e consentire, ad esempio, l'aumento delle ore di assistenza domiciliare, perché le persone che si dedicano alla cura - soprattutto le madri di figli con disabilità

questa legge di bilancio possa essere ulteriormente rinforzata, soprattutto nel reddito di inclusione, perché abbiamo bisogno di rafforzare ancora di più l'infrastruttura sociale per accompagnare le persone fuori dalla povertà, sostenendo per questo il lavoro degli assistenti sociali, che si devono prendere cura delle persone persone che hanno bisogno. C'è una questione che mi sta particolarmente a cuore, che parla di un sostegno al tessuto economico e sociale delle piccole e medie imprese. Abbiamo avuto un grande risultato con i piani individuali di risparmio: auspico che ciò possa essere davvero

una legge di bilancio, che sarà più equa e più giusta, come ho detto, sia per i giovani, sia per le persone in età di pensione. Credo che si legga in questi interventi, trasversalmente, anche un abbraccio tra generazioni, oltre alle azioni che serviranno allo sviluppo e alla crescita, perché di questo abbiamo bisogno, anche per prenderci cura del tema della denatalità. La politica pubblica deve infatti sostenere trasversalmente, con il lavoro e anche con interventi che favoriscano l'accesso alla pensione, la scelta libera delle famiglie, delle persone e soprattutto delle donne, di mettere

signore e signori Vice Presidenti, Vice Ministri, Sottosegretari, membri di questa Assemblea, onorevoli senatori, ma preferisco chiamarvi, semplicemente, colleghi, voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno dato la piena fiducia e che mi - e ci - hanno riscaldato il cuore durante tutti questi anni di lavoro, silente e solitario, con le loro talvolta ferme, ma sempre sagge parole, anche se durissime, come nel caso della ministra Anna Voglio ringraziare coloro che mi hanno supportato e, certamente, spesso sopportato. Ringrazio coloro che erano amici e che si sono persi, ma grazie ai quali comunque sono qui. Ringrazio coloro che sono divenuti nuovi amici e anche coloro che ho ritrovato, grazie al comune sentire su temi comunemente condivisi e aggreganti. Grazie colleghi, a tutti voi veramente grazie, perché avete contribuito a rendermi forte nelle mie convinzioni, perché avete contribuito a spingermi oltre i miei limiti e oltre ogni ragionevole audacia, perché, in alcuni casi, insieme, abbiamo dimostrato che è vero che l'unione fa la forza. Io, noi e voi abbiamo spinto il cuore oltre l'ostacolo e abbiamo dimostrato al Paese, e a quanti erano diffidenti, che unirsi attorno a temi veri, di interesse comune, era ed è possibile, oltre ogni differenza di colore e credo politico. Tra tutti voi, ma senza con questo voler escludere nessuno, il mio grazie (in tal senso credo di interpretare un comune sentire di affetto di quest'Assemblea) va al presidente Zavoli, che mi ha sempre sostenuta. Non posso che ringraziare Aldo Bonfrisco e Anna Cinzia che, dal primo ordine del giorno, hanno abbracciato questa causa mettendomi a disposizione anche le loro risorse. Noi abbiamo dimostrato che fare del bene al Paese oggi è ancora possibile e non è una *fake news*. Voglio ringraziare infine tutte le associazioni, le mamme e i papà che da fuori del palazzo mi hanno dato la forza e il coraggio di andare avanti: #unaleggesubito su Facebook è un luogo dove trovarne molti. Vi invito a leggere le loro storie. Colleghi, vi sono molte ragioni per cui oggi potrei usare l'«io» per rivendicare quanto fatto, ma io in quest'Aula sono nulla senza di voi. Quindi da questo mio discorso emergerà solo il «noi», non perché abbia deciso di non vedere i mille ostacoli che mi sono stati scientemente posti innanzi, non perché non voglia vedere chi vuole strumentalizzare, anche di fronte all'evidenza più palese, che non si può fare campagna elettorale su questo tema, tantomeno non attribuirne il risultato alla sottoscritta e ai 133 colleghi che per primi hanno firmato l'iniziativa. Dalla tenacia con cui abbiamo perseguito e raggiunto questo obiettivo, emergerà solo un «noi», per due motivi: perché in una democrazia la parte si perde nel tutto e perché in politica, come nella vita, occorre saper perdonare. Ma anche perché migliorare se stessi e il mondo in cui viviamo passa e si concretizza nelle azioni che ognuno di noi compie ogni giorno, con il proprio lavoro e con il proprio talento. Le disonestà intellettuali, le appropriazioni indebite non mi appartengono. Quella che noi oggi abbiamo raggiunto *in extremis* in questo disegno di legge di bilancio, senza differenza di colore politico, è una conquista storica per il nostro Paese. Tutta l'Europa ce lo chiede e i nostri cittadini da più di vent'anni: parlo del riconoscimento della figura del *caregiver* familiare. Per risolvere un problema il primo passo è riconoscere che il problema esiste. Ora rivolgo ai membri della Commissione di bilancio uno spunto

un accudimento continuo, assiduo, rigoroso e tenace, ma siete stanchi, distrutti e portate sul vostro corpo i segni della stanchezza. Loro, i *caregiver* familiari non hanno una fine della sessione di bilancio, loro compiono questo lavoro non da settimane, ma da trent'anni e forse più. Trent'anni di lavoro duro, trent'anni passati a fatica, e loro non possono augurarsi la fine: sarebbe chiedere all'amato, alla persona cara, di venire meno e questo è impossibile. Ecco come sono: sono vite di persone che non sono disabili. I *caregiver* familiari assistono i loro cari perché non sono in grado di prendersi cura di sé e non sono in grado di assolvere ai propri bisogni primari. Queste persone li assistono tutto il tempo, privati del diritto al riposo e del diritto alla salute. Come li definisco da sempre, sono innocenti agli arresti domiciliari. Loro non hanno scelto di compiere questa missione, non sono volontari. Loro sono incatenati ai loro assistiti, alle loro abitazioni, spesso rinunciano persino al lavoro o lo perdono per dedicarsi al loro ruolo di cura. Questi eroi, a cui lo Stato sino ad oggi ha negato anche il solo riconoscimento del nome, oggi esistono. Potrà non piacervi il termine inglese, magari difficile da dire per qualche mezzobusto del TG, ma loro sono i *caregiver* familiari. Noi abbiamo reso possibile questo primo imprescindibile passo:

ma ci sono e serviranno a finanziare solo iniziative legislative che entreranno nel merito: chi fa la divisione del totale per un numero, probabilmente non ha letto il testo. Abbiamo il fondo, abbiamo una definizione precisa e puntuale che non lascia spazio ad interpretazioni di fantasia e riguarda una platea di milioni di persone che si prendono cura del loro congiunto. Ecco, quelle leggi cui ci si riferisce nell'emendamento approvato all'unanimità, con le firme di tantissimi di noi e di tutti i Capigruppo - mi dicono che sia la prima volta in questa legislatura e un po' me ne compiaccio - devono guardare a quella figura che ora noi riconosciamo come *caregiver*; devono definire le priorità con cui potranno accedere ai benefici loro riservati in ragione della gravità e durata della malattia del loro assistito, per poter soddisfare i molti bisogni sinora negati. Tra questi penso alle necessità occupazionali, perché molte di queste persone rinunciano alla propria realizzazione professionale perché devono dedicarsi alla cura del loro caro; rinunciano al diritto alla salute perché, per accudire il loro caro, che non possono lasciare solo, rinunciano a curare se stessi, così come rinunciano al diritto alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Per Per coloro che lavorano e hanno parenti ammalati, infatti, la vita spesso diviene un inferno e il rischio di essere ingiustamente licenziati è sempre altissimo, grazie anche alle misure adottate in questa legislatura che hanno annullato i diritti dei lavoratori: basta guardare alla vicenda della mamma sola con due bambini, di cui uno disabile, licenziata recentemente da Ikea. Penso alla possibilità di lavorare realmente da casa, con il telelavoro, al diritto ad una pensione dignitosa attraverso una contribuzione figurativa per coloro che non hanno mai potuto lavorare: non coloro che non hanno lavorato, ma coloro che non hanno mai potuto lavorare o hanno rinunciato al lavoro per assolvere al loro ruolo di cura. Penso al diritto di andare in pensione prima degli altri, perché fare il *caregiver*

Possiamo rinnovare il sistema del *welfare*. Molte iniziative non sono onerose, ma potrebbero modificare sostanzialmente la vita di queste persone. Non vogliono soldi, vogliono diritti finora negati. Per questo ribadisco il mio appello al presidente Grasso, alla presidente Boldrini e al presidente Mattarella, perché ci consentano di chiudere questa legislatura approvando dei provvedimenti che non sono divisivi, come possono essere altri, e che ci permettano di lavorare e di dare il via libera ad una legge quadro sui *caregiver* che, come dimostrato in Commissione bilancio, ha saputo unire tutti, nessuno escluso, anche i più scettici che hanno atteso il voto per sottoscrivere l'emendamento, ai quali pure va il mio grazie. Devo lasciare a voi, voi che tornerete su questi scranni, un appello: non dimenticatevi dei *caregiver*, di coloro che da fantasmi si alienano per un compito gravosissimo, che è un risparmio assolutamente dimostrato per le finanze pubbliche: mandiamoli in pensione, riconosciamo questo lavoro di cura con contributi figurativi, non lasciamo che muoiano,

voi che vantate grande successo e che avete qualcuno che vi rappresenta nell'altro ramo del Parlamento.

perché il voto di fiducia è sempre un voto politico, ma con l'esempio e la dimostrazione che la politica può essere diversa: la politica può essere aggregante e può essere anche l'occasione per una senatrice per caso, sola, ma determinata, di mettere un mattoncino anche in una legislatura sciagurata come questa e, nonostante tutto, degna di essere ricordata per quanto abbiamo fatto per i *caregiver. Ciò rende tutti noi fieri di poter dire che abbiamo fatto qualcosa, un piccolo passo, ma qualcosa; un segno che, volendo, si possono iniziare a risolvere i problemi di tutti. Sì, i problemi di tutti, ricordiamolo: non i problemi dei "poverini", non quelli degli sfortunati, perché nella vita o si cura o si è curati. Quindi, quello che abbiamo fatto ora sarà anche per noi, lo stesso «noi» che, salutandovi, ringrazio.

a parte le pochissime cose buone che sono entrate in questa legge di bilancio, con emendamenti condivisi e votati all'unanimità, come quello a cui faceva riferimento la collega Bignami adesso, la gran parte delle disposizioni e lo stesso impianto della legge di bilancio hanno delle criticità e c'è necessità di disvelare delle menzogne, delle non verità che sono e saranno rappresentate da parte del Governo e della maggioranza che lo sostiene. Ma su questo questo interverranno i miei colleghi, più qualificati di me, che hanno seguito i lavori interamente. Lo faremo in sede di dichiarazione di voto. Personalmente, vorrei impiegare il tempo a mia disposizione per soffermarmi su un altro aspetto, che invece non è stato oggetto di discussione pubblica, ovvero su uno scampato pericolo. Quindi è una buona notizia voglio essere ottimista: l'ottimismo della ragione e della presa d'atto. Parlo di scampato pericolo con riferimento ad alcuni emendamenti di provenienza parlamentare presentati alla legge di bilancio che avrebbero voluto voluto causare sostanzialmente un terremoto nella giustizia civile in questo Paese. Un emendamento era della Lega ed è stato prontamente ritirato, il secondo emendamento, che è stato sottoposto al voto alla fine della seduta di due giorni fa, fa, avrebbe modificato il codice di procedura civile introducendo il cosiddetto rito sommario come rito ordinariamente applicabile a tutte le cause civili che sono di competenza del giudice monocratico (cioè non decise dal tribunale collegiale), che credo rappresentino peraltro l'80 per cento dell'intero contenzioso civile. di quelle lungaggini processuali anche in ambito civile di cui tanto si parla quando si sente ripetere, troppe volte, che vi è necessità di velocizzare la giustizia, quanto il sistema economico italiano sia danneggiato da una giustizia inefficiente, lenta quand'anche ingiusta. pia illusione - perché dobbiamo concedere il beneficio della buona fede a chi ha avanzato proposte modificative di tal fatta - quella secondo la quale, modificando il rito, cioè le regole procedurali delle cause civili, si possa ottenere una velocizzazione dei tempi. È solo una pia illusione, come è stato spiegato e illustrato da chi, resosi conto di questo pericolo devastante, ha fatto sentire la propria voce, una volta tanto unanime: i magistrati

da parte della senatrice Vicari con la singolare circostanza, che ho potuto notare personalmente, essendo presente in quel momento in Commissione bilancio, della recalcitranza dell'altra parte della maggioranza, ossia del Partito Democratico: mi riferisco al senatore Santini che, nel sentire dell'avvenuto ritiro, si è quasi sollevato incitando la collega Vicari a non ritirarlo perché era un emendamento importante.

o di componenti del Partito Democratico non meglio identificati, di riproporre questa modifica - ribadisco: devastante e proverò a spiegare sinteticamente perché

operare questo terremoto nella giustizia civile che, come ho detto, è solo un'illusione di velocizzazione dei procedimenti civili. Infatti, il collo dell'imbuto e i rallentamenti avvengono nella fase decisionale e non nelle modalità con cui con cui una causa viene introdotta e non è il limitare le facoltà della difesa delle parti nel rappresentare le prove, chiedere interrogatori e depositare memorie

di smantellare il sistema giustizia - dice: "Se quelle sommarie durano poco, rendiamole tutte sommarie, così risparmiamo tempo e finalmente avremo una giustizia civile veloce". Senonché, è facile capire che spostando milioni di giudizi civili da un rito all'altro, a parità di risorse disponibili e di numero di magistrati, di cancellieri

operando sul codice di procedura civile: quello che occorre è destinare maggiori risorse. So bene che non è un periodo felice quello in cui, da una parte e dall'altra, si evoca la necessità di impiegare più risorse

su questo aprirei un'altra discussione che non è il caso di fare qui). Cerchiamo di capire come migliorare la macchina giustizia, potenziando ed efficientando i procedimenti e l'amministrazione delle risorse umane disponibili, premiando i giudici che lavorano meglio e più velocemente, punendo ancor più le parti e i loro avvocati che magari incardinano giudizi temerari, applicando la condanna per spese temerarie in maniera più decisa. Non tocchiamo però i codici,

che una volta si chiamavano bolli e oggi contributi unificati per iniziare la causa. Altra follia che è stata fugata. Ma come è stato possibile che siano stati dichiarati ammissibili dalla Presidenza della Commissione bilancio questi emendamenti che, ribadisco, incidevano pesantemente a livello procedurale? di altri emendamenti, tra i quali a me piace ricordare - anzi è doveroso che lo ricordi in questa sede - un emendamento, anch'esso di natura procedurale e ordinamentale, che avrebbe cambiato solo quattro parole a un comma di un articolo del codice di procedura civile. Era un emendamento a mia prima firma e a firma di altri colleghi del Movimento 5 Stelle,

il debito originario, nei confronti per lo più delle banche, ma anche di qualunque altro tipo di creditore, viene inciso in maniera minima, se non nulla, e il ricavato serve a soddisfare le spese della procedura. La morale, il finale della storia, è che il debitore rimane debitore, senza più la casa o l'impresa, il creditore non prende un euro e chi ci guadagna è chi si aggiudica un bene a un prezzo estremamente vile, e questo è già un danno di per sé. Quando, poi, a questo si accompagnano possibili interferenze o vicinanze di torbidezze nell'ambito sociale o anche della malavita, intorno al sistema delle aste immobiliari, capite bene che stiamo creando dei disastri veramente imperdonabili. Come è possibile allora che il nostro emendamento sia stato dichiarato inammissibile e un altro emendamento, che modifica mezzo codice di procedura civile, procedura civile, sia stato dichiarato ammissibile? Ovviamente, devo stigmatizzare i criteri valutativi della Presidenza della Commissione bilancio.

chi avrà la responsabilità di presiedere le Commissioni bilancio di Camera e Senato nella prossima legislatura e le maggioranze che si potranno formare o la maggioranza che si formerà abbiano

interessi di pochi o addirittura incompetenze inconfessabili, perché se l'emendamento sul rito sommario è stato veramente auspicato o sospinto da poteri vicini a Confindustria o da associazioni di imprese che credevano che, con il rito sommario adottato così, si velocizzasse la giustizia, allora vi è un problema di competenza, che evidentemente non riguarda coloro che, quasi quotidianamente, nel *mainstream* mediatico, vengono additati come sommo esempio di incompetenza. *(Applausi

il Parlamento si articola al suo interno, oltre che nei Gruppi, anche in Commissioni di merito. Vi sono Commissioni che trattano questioni che attengono ad alcune materie e altre Commissioni, come la Commissione bilancio, che invece hanno l'obbligo di trattare la generalità delle materie. Lo fa sistematicamente affrontando il problema dei provvedimenti legislativi dal punto di vista dell'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione lo fa anche e soprattutto quando esamina la manovra di bilancio.

triennio, in ragione delle compatibilità finanziarie, si stabilisce di destinare a questo o a quell'argomento che si ritiene più urgente. La manovra di bilancio riguarda tutta la spesa dello Stato, anche la partita delle entrate e quindi il il modo in cui si attingono le risorse e si chiamano i cittadini, il sistema delle imprese e chi lavora in questo Paese a contribuire all'organizzazione della macchina pubblica e alla risposta rispetto ai bisogni sociali. Dico questo perché abbiamo compiuto passi in avanti, in questi cinque in questi cinque anni così turbolenti sotto il profilo politico, con una maggioranza che non esce fuori da un voto chiaro che ha indicato una delle parti come vincitrice

milioni di euro del triennio, perché questo è quello che viene descritto nelle tabelle del bilancio e questa è la spesa che deve affrontare lo Stato per mantenere se stesso, intervenire nell'economia, sostenere interventi sociali, garantire sicurezza,

che lo sviluppo dell'economia e della società del Paese sia adeguato alla sua forza e alla sua capacità

risposte già definite. Quando noi parliamo, ad esempio, del personale pubblico, signor Presidente, non ci riferiamo solo al segmento dei precari di ultima generazione, ma a tutti coloro che già lavorano da decenni all'interno della macchina pubblica e che continuano a lavorarci e quindi il bilancio dello Stato serve a conservare il lavoro di coloro che ce l'hanno, serve a

Il mondo ci dice che dobbiamo dare una risposta in merito alla sicurezza, che i nostri operatori delle Forze dell'ordine

non perché il sistema dell'ordine pubblico in questo Paese sia allo sbando, anzi è uno dei migliori sistemi di ordine pubblico, anche il nostro sistema di tutela della salute. Non c'è bisogno di rifare tutto e se qualcuno ha la pretesa domani di venire qui a dire che bisogna rifare tutto, vuol dire che è nello stadio della follia pura. nello stadio della follia pura. Bisogna stare attenti, perché questo è il ragionamento politico da mettere in campo quando si parla di bilancio.

quando una cosa non funziona, è grazie al fatto che l'insieme funziona e se noi abbiamo un sistema sanitario che ha delle pecche è perché abbiamo un sistema sanitario, non perché non ce lo abbiamo, perché se lo dovessimo fare dalla a alla zeta, saremmo in una condizione di disperazione.

quello che c'è già. Lo voglio dire perché ci sono alcune cose che, ad esempio, rappresentano una conquista veramente innovativa. la senatrice Bignami, intervenendo sulla questione dell'assistenza e del riconoscimento della funzione dei famigliari che si prendono cura dei loro congiunti più sfortunati, un riconoscimento che per la prima volta viene dato, inserendo una figura nell'ordinamento ne riconosce formalmente la funzione come una funzione sociale. Voglio citare un'altra che sembra possa passare sotto silenzio: abbiamo approvato un emendamento che riguarda le procedure di bonifica dei poligoni di tutta Italia, che è esattamente, nero su bianco, quello che bisogna cominciare a fare per evitare che i nostri militari, quelli che difendono il nostro Paese, quando si preparano e sono sul campo di esercitazione non rischino sotto il profilo della salute. È il risultato di indagini parlamentari di primissimo piano svolte in questa e nella precedente legislatura, soprattutto alla Camera dei deputati, deputati, dalla Commissione sull'uranio impoverito. Grazie a quel lavoro, oggi abbiamo un corpo di disposizioni e dotazioni finanziarie perché entro 180 giorni dal momento dell'esercitazione si proceda a fare la bonifica del poligono per tutelare la salute e l'ambiente dei territori limitrofi al poligono, ma soprattutto la salute dei nostri militari. *(Applausi

il munizionamento che si utilizzano sono fatti per ammazzare subito e anche nel tempo. E quando siamo costretti ad utilizzare questo tipo di strumenti, dobbiamo sapere

Questa è la legge di bilancio. Abbiamo lavorato in modo molto trasparente in Commissione, rispondendo ad ogni emendamento presentato dalla maggioranza e dalla minoranza, e sul corpo

Abbiamo avuto sensibilità e rispetto per l'accordo fatto dal Governo sulle pensioni, votandolo convintamente in molti.

Cito in particolare uno fra gli emendamenti da me proposti, e puntualmente respinti, quello a favore dei datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2018 avessero garantito il livello di occupazione medio fatto registrare negli ultimi cinque anni, - a nostro modo di vedere - l'esonero del versamento del 25 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico appunto del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo pari a euro 7.000 su base annua.

state, hanno garantito la stabilità economica dei loro dipendenti e, soprattutto, la professionalità delle proprie aziende. Oppure la mia proposta per sostenere la promozione di forme di imprenditoria in agricoltura, per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali con età inferiore ai quarant'anni, anch'essa respinta. proposte di aiuti concreti fatte da chi sa cosa sia fare attività d'impresa, specie dove è più difficile, ossia al Sud, e quanto sia più importante dare priorità all'economia reale piuttosto che alle alchimie contabili di chi si preoccupa solo di «fare i compiti a casa». Tuttavia la manovra è stata contraddistinta da uno *stop and go* continuo, in attesa che la maggioranza di Governo (maggioranza che - come è di tutta evidenza -non esiste più) si mettesse d'accordo e trovasse una qualche intesa sui vari punti.

come si vuol far credere, guardando all'Europa, quella stessa Europa che, comunque, resta molto critica nei confronti del Governo, specialmente sull'aumento poderoso del debito pubblico avvenuto negli ultimi anni. Questa manovra, dicevo, è il frutto di una precisa scelta politica o, meglio, di una totale inerzia, mista a una drammatica assenza di idee, coraggio e soprattutto lungimiranza in materia di politica economica. Ne abbiamo avuto un esempio anche nel recente decreto fiscale: abbiamo preso atto con soddisfazione che il Governo ha riconosciuto la validità delle nostre argomentazioni inserendo un emendamento per l'introduzione dell'equo compenso. La soddisfazione è stata però, purtroppo, solo parziale perché se ci si fosse mossi in tempo si sarebbe potuto migliorare il testo affinché potesse soddisfare a pieno le legittime aspettative di tutti gli ordini professionali.

mentre la corsa al ribasso del costo delle prestazioni fa inevitabilmente scendere anche la qualità dei servizi offerti e, di conseguenza, la soddisfazione dei cittadini. impegno, dunque, continuerà per estendere all'intera platea degli interessati l'accesso all'equo compenso. Tornando al disegno di legge di bilancio 2018 nel suo complesso, come abbiamo già avuto modo di constatare, su un totale di circa 21 miliardi di euro, miliardi di euro, ben 14,9 sono destinati ancora una volta a evitare l'applicazione degli aumenti dell'IVA, imposti dall'Europa a garanzia della tenuta dei conti pubblici. secondo il Governo, un disegno di legge di bilancio scritto in funzione di quelle clausole di salvaguardia da tempo introdotte a garanzia del rispetto del percorso di rientro dei nostri conti pubblici. Oggi il Governo è qui a chiederci di approvare una manovra molto severa che segue un sentiero stretto che, nel suo complesso, rischia di compromettere seriamente i pur timidi segnali di ripresa in atto della nostra economia. Il ritardo con cui arriviamo a questo appuntamento, con questa legge di bilancio, è la prova lampante delle difficoltà del Governo nel chiudere i conti. Il ritardo è doppiamente colpevole perché pregiudica il diritto del Parlamento ad affrontare una seria discussione sul testo che ci è stato presentato. L'intento ci appare chiaro: chiamarci in questa sede a un estenuante lavoro di ratifica in Commissione, poco più che formale, su un disegno di legge di bilancio che nei fatti è stato discusso e deciso altrove. deciso altrove. Dal novembre 2011, sei anni di Governi, prima tecnici e poi di centrosinistra, hanno dilapidato la nostra credibilità internazionale e portato l'Italia alla totale irrilevanza in Europa. La vicenda dell'EMA è solo l'ultima conferma in ordine di tempo. La politica economica del centrosinistra è sempre stata ispirata ad un'alta imposizione fiscale, ad accontentare i fortunati di turno che, guarda caso, non sono mai le famiglie italiane a cui destinate davvero risorse Da parte vostra c'è la rinuncia a qualsiasi seria politica pubblica di investimento, si va avanti solo alla cieca e l'inserimento del milleproroghe come emendamento nel testo della manovra è la prova provata che ormai non c'è più tempo per rimediare, non c'è più tempo per programmare perché non c'è più il Governo e si aspetta solo lo scioglimento delle Camere. Il vostro ultimo atto è una manovra ancora una volta figlia dell'austerità e di quella stessa visione che ha prodotto politiche economiche sbagliate, che hanno aggravato e allungato la crisi, aumentando ulteriormente le disuguaglianze. Disuguaglianze che non saranno certo ridotte da qualche mancia elettoralistica come gli 80 euro. Disuguaglianze che abbiamo visto perpetuarsi anche sul tema delle pensioni, per cui categorie professionali possono giustamente usufruirne ad un'età più bassa, mentre altre categorie dello stesso livello, che ne avrebbero anch'esse egualmente diritto, purtroppo non possono farlo. Però ci piacerebbe sapere, dal Governo e dalla maggioranza tutta, se hanno almeno fatto una stima del costo complessivo, nonché dell'impatto sui conti pubblici, delle misure prese in questi anni per sterilizzare, di volta in volta, le famose clausole di salvaguardia. E ancora, quanto hanno pesato e pesano decine di miliardi che non si sono potuti impiegare in investimenti, ricerca e sviluppo, misure di contrasto alla povertà in altri modi analoghi? Ve lo siete mai chiesto? E quanto pesa l'impossibilità di mettere in campo politiche pubbliche di sviluppo, dal momento che circa tre quarti della manovra sono bloccati da queste clausole? Un programma di seri tagli alla spesa, a nostro avviso, e di investimenti mirati (non certo *bonus* e mancette a pioggia), unito a un lavoro di diplomazia in sede europea determinato davvero a rimettere in discussione questi limiti ormai sorpassati, avrebbero almeno rappresentato la degna contropartita per quel che oggi ci venite a presentare. Ed è per quello che ho parlato di mancanza di coraggio, quel coraggio che oggi sarebbe necessario per ammettere di aver sbagliato, con scelte che hanno contribuito a mantenere in questi ultimi anni l'economia italiana al palo, mentre quelle degli altri Paesi già ricominciavano a marciare. E invece no, al coraggio s'è preferita la furbesca scappatoia del trucco contabile. Come definire, altrimenti, la scelta del Governo di spostare dal 2019 in poi gli impegni di spesa che avrebbero le maggiori ricadute, in un Paese in cui la disoccupazione giovanile è già oggi quasi al 36 Permettetemi un esempio (ma ne potrei fare tanti, scorrendo gli articoli di questa manovra): avete deciso di stanziare 100 milioni di euro l'anno per la mobilità sostenibile. Una somma importante, che può liberare potenzialità notevoli in un settore che guarda al futuro, tanto per la creazione di posti di lavoro ad alta qualificazione, quanto in termini di politiche industriali e per l'ambiente. Quindi, con la lealtà propria di una forza di opposizione costruttiva, a voi andrebbe il nostro plauso. Peccato, però, che non sia così: i 100 milioni l'anno sono previsti dal 2019 al 2033. Per il 2018, l'importo previsto è zero. Questo era solo un esempio, ma potrei citarne altri, come gli impegni per «l'assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca», anche questo sottaciuto. Ma ormai il tempo è scaduto. Fra poche settimane il potere di decidere tornerà finalmente nelle mani dei cittadini che sapranno giudicare e scegliere. Soprattutto dal Sud, vi assicuro, che voi avete dimenticato, ci aspettiamo una grande spinta di cambiamento: siamo certi che gli italiani premieranno Forza Italia e il centrodestra come unica risposta seria e credibile ai fallimenti della sinistra. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, di questo disegno di legge di bilancio vorrei mettere in evidenza le misure relative agli interventi strutturali in materia di patrimonio culturale, misure che hanno dato l'opportunità alla 7a Commissione del Senato di poter intervenire con proposte che sono state considerate migliorative e, quindi, accolte in fase emendativa. e, quindi, accolte in fase emendativa. Un buon lavoro di interlocuzione con il Governo, e di questo ringrazio i relatori, il vice ministro Morando, ma anche tutti i colleghi della 7a Commissione che hanno attivato un importante gioco di squadra anche con l'altro ramo del Parlamento, al quale la prossima settimana passerà il compito di continuare l'esame. Anche questa legge di bilancio conferma l'impegno del MIBACT nella ristrutturazione dell'articolazione interna e nel rafforzamento delle risorse umane. Con questa ulteriore misura, 200 ulteriori assunzioni, si arriva a quota mille assunzioni che costituiscono, comunque, ancora un tassello, pari a circa i due terzi, rispetto a un percorso ancora più ambizioso di assunzioni e Altre misure intervengono per prorogare i contratti a tempo indeterminato, per stabilizzare (con un emendamento parlamentare) e per dare una maggiore flessibilità nell'avvalersi di figure professionali utili alla programmazione da parte dei poli museali e dei siti archeologici. Anche l'implementazione del contingente dei Carabinieri specializzati nel settore dei beni culturali, così come una risorsa aggiuntiva per la prestazione accessorie dallo straordinario, vanno in questo senso. Importante è la risorsa per l'anno europeo del patrimonio. Il 2018 sarà una grande opportunità per l'Italia e per l'Unione europea per promuovere le diversità culturali, il dialogo interculturale e la coesione sociale; per rafforzare il contributo del patrimonio culturale dell'Europa ad uno sviluppo sostenibile, che avviene mediante il rafforzamento dei settori culturali e creativi, comprese le piccole e medie imprese la promozione del patrimonio culturale, come elemento imprescindibile delle relazioni tra l'Unione europea e gli altri Paesi. In questo senso cito anche il comma relativo alla conferma dei fondi per la Capitale della cultura: sappiamo di Mantova e di Pistoia e aspettiamo, nel 2019, Matera come capitale europea. Sono tutte importanti operazioni volte a imprimere un cambiamento alle città e al territorio circostante con interventi complessivi. molto importante - e non posso non esprimere grande soddisfazione in proposito -, dopo l'approvazione della legge sul cinema e l'audiovisivo e il nuovo codice dello spettacolo, il contenuto del comma 13,

quindi applicata la riduzione dell'IVA anche quando le operazioni dei contratti connessi siano effettuate da un intermediario. Si tratta di una misura molto attesa dal mondo dello spettacolo, che completa le tante contenute nella legge sullo spettacolo. la 7a Commissione, in una risoluzione approvata all'unanimità nel 2015, di cui sono stata relatrice, aveva già indicato al Governo, che abbiamo più volte proposto e su cui era stato presentato anche un ordine del giorno in occasione dell'esame del provvedimento sullo spettacolo dal vivo: sono certa che il mondo delle arti performative l'ha recepita con grande attenzione e soddisfazione. Purtroppo da allora - e mi risulta da molti anni - non si riesce a dare invece alla luce la detrazione fiscale per le famiglie con figli minori che frequentino corsi di musica o di teatro. Si è provato a restringere il campo per far partire una sperimentazione, che avrebbe potuto essere utile per il futuro, offrendo dati di cui non siamo in possesso. Molti erano gli emendamenti in tal senso da parte del superamento di una disequità di trattamento tra sport e cultura. Con questo, naturalmente, esprimo soddisfazione per l'attenzione al mondo dello sport contenuta nell'articolo 40 del provvedimento in esame, ma la richiesta di detrazione fiscale per la frequenza di corsi, avanzata da anni da tantissimi portatori di interesse, è una misura di contrasto alla povertà educativa, è un sostegno alla famiglia, ma è anche un sostegno al terzo settore, è un modo per regolamentare la costellazione di erogatori del privato sociale,

Grazie costituisce una grande opportunità per contrastare un fenomeno, che troviamo ampiamente documentato e che - non possiamo nascondercelo - è di consistente gravità. La crisi della lettura e del libro non ha più un carattere contingente, ma strutturale e va affrontata con una legge quadro, peraltro già in fase avanzata nella 7a Commissione della Camera: una legge che si occupa di tutta la filiera, dalla produzione letteraria, all'editoria, al sostegno della lettura anche nei luoghi pubblici, come le biblioteche. Per questo tema un grande ruolo

un Piano delle arti, che comprende tra le aree della creatività proprio quella della scrittura creativa. D'altra parte, la cosiddetta 18App, la carta cultura per i diciottenni, che in questa manovra di bilancio viene resa strutturale, ci racconta che il 70 per cento delle spese è rivolto ai libri, naturalmente anche di testo e naturalmente anche *e-book.* In fase emendativa è stata inserita quindi una misura intitolata *tax credit* per le librerie, ovvero un credito di imposta nel settore della vendita di libri al dettaglio in crisi da anni e a cui si dà risposta soprattutto alle librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali (fino a 20.000 euro) e per metà alle librerie gestite direttamente dai gruppi editoriali. Queste misure, insieme all'*art bonus* alle biblioteche pubbliche,

importante consumo di libri e che dal 2010 conosce invece una regressione. Tanti i punti su cui riflettere, ma certamente un obiettivo da perseguire con un'attenzione a tutto tondo: una legge quadro che mi auguro si possa realizzare nella prossima legislatura, così come si è fatto per altri settori del Ministero della cultura. Leggo soltanto una frase da un rapporto del 2016 sull'editoria: «I giovani hanno tutti grande familiarità con le tecnologie, ma chi proviene da famiglie in cui i consumi culturali si limitavano a quanto fluiva dagli

Nessuno vuole combattere le nuove tecnologie e lo si rileva anche dalle conclusioni di una risoluzione, approvata in Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza, sui diritti alla fruizione del patrimonio, che, appunto, riconosce come siano importanti gli strumenti tecnologici, ma riconosce anche i limiti dei *device* e l'importanza della materialità, del fare con mani pensanti, integrando corpo e mente. signor Presidente, richiamando un altro importante impulso che noi colleghi della Commissione per l'infanzia e l'adolescenza abbiamo raccolto e che ha avuto un percorso positivo grazie all'attenzione del Governo: mi riferisco ai *care leaver*, i diciottenni che vedono terminare i propri percorsi fuori famiglia - come possiamo immaginare - non sono in grado, nella stragrande maggioranza, di vivere una dimensione di completa autonomia. Un'importante interlocuzione con la loro rete *network* - e qui il *web* assume un grande valore, perché unisce e rafforza le istanze di esigibilità dei diritti - ci ha permesso di entrare in contatto con loro

non solo il merito di dare una risposta al bisogno di accompagnamento verso l'autonomia fino al ventunesimo anno, ma dà modo anche alle politiche di intervento di sperimentare le migliori pratiche a supporto di questi adolescenti, anche se più grandini, che hanno diritto all'autodeterminazione, un diritto impossibile se non sostenuto, perché terminino i propri percorsi di studio e di inserimento nel lavoro.

un altro è l'intervento sulla previdenza; poi c'è un insieme di norme, variamente sparse in diversi articoli, relative ad ammortizzatori sociali e stabilizzazione e, infine, vi è qualcosa sulle politiche attive.

che ci ha coinvolto per dieci anni e che, sulle questioni del lavoro, ha determinato condizioni di disagio fortissimo e una segmentazione della platea dei lavoratori

una presenza molto relativa dei contratti a tempo indeterminato. Se si analizzano le situazioni, c'è però un'esplosione dei contratti a tempo parziale: si tratta di un *part-time* involontario, molte volte

articolati in questo modo: si riducono i contributi previdenziali per i datori di lavoro privati per assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2018 in favore di soggetti tra i trenta e i riduzione che dura al massimo trentasei mesi, con 3.000 euro su base annua. C'è poi la possibilità per alcune Regioni di introdurre misure complementari. Per il lavoro autonomo, invece, ci sono interventi che prevedono l'esonero contributivo triennale per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli di età inferiore a quarant'anni. C'è poi un'ultima misura prevista, quella della riduzione dello sgravio contributivo per le imprese armatrici. Questo è l'intervento dal punto di vista occupazionale. La caratteristica che osserviamo è che un intervento di questo tipo, molto parziale, con una riduzione dei contributi senza nessun tipo di sanzione e di controllo affinché non ci siano licenziamenti alla fine dei contributi,

che hanno le difficoltà più forti. Penso che questo dovrebbe orientare le misure di un Governo; noi, invece, ripetiamo ancora questo tipo di segmentazione, la aggraviamo e, inserendo alcuni elementi, rendiamo molto più rigido tutto il sistema. Farò poi un'altra serie di riflessioni, signor Presidente, ma ora vorrei parlare di come si interviene sulla previdenza.

Quello che abbiamo avuto è quello che c'è: proroga di un anno, dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019, dell'istituto sperimentale dell'APE volontaria. Signor Presidente, sto parlando della previdenza particolare che permette, in certe condizioni, di andare in pensione tre anni prima della scadenza, attivando un mutuo, garantito dal Governo per una serie di situazioni, che i lavoratori restituiranno durante il periodo di pensionamento.

ai lavoratori di andare anticipatamente in pensione senza dover pagare la pensione per questi tre anni. Ci siamo trovati di fronte a situazioni molto particolari perché, per come era stato scritto il provvedimento,

Sei mesi di contributi in più per le donne, per ogni figlio fino a un massimo di due anni, ma solo nel caso di donne che abbiano i requisiti per aderire all'APE *social*, e non come regola generale del sistema previdenziale. Presidente, le donne di questo Paese non vedono riconosciuti dal punto di vista previdenziale né il loro lavoro di cura né il loro lavoro riproduttivo.

settoriale, specifico e parziale, perché genera aspettative e conflitti. Con un emendamento del Governo

di aumento per l'aspettativa di vita nel 2019. Questo significa che nel 2021 per queste categorie si ricomincerà a contare l'aspettativa di vita. Non è una misura strutturale nel tempo,

l'altro, ci sono problemi su come è stato scritto il provvedimento, perché rischiamo che per accedere a questo tipo di intervento ci siano difficoltà come quelle dell'APE *social*. Ci sono delle ambiguità: si parla di anni di lavoro,

fosse stata impiegata in investimenti produttivi diretti, fatti dal pubblico, con la possibilità di riattivare lo sviluppo in Italia con un intervento diretto del pubblico che affrontasse le questioni relative alla ristrutturazione, alla riorganizzazione e alla cura alla cura del territorio, coinvolgendo direttamente gli enti locali. Signor Presidente, il punto fondamentale è la riqualificazione e la rivalorizzazione del lavoro. Noi avevamo proposto una serie di interventi, come, ad esempio, il reinserimento della causale per limitare l'intervento dei contratti a termine.

Però il punto fondamentale è questo: noi abbiamo una situazione nei luoghi di lavoro che sta degenerando. Abbiamo visto tutti i lavoratori di Amazon: è una situazione in cui ritorniamo al vecchissimo terrorismo, con la parcellizzazione e i ritmi fortissimi a cui è impossibile sfuggire. Abbiamo visto anche i lavoratori impegnati nella catena delle carni delle carni della Castelfrigo, a Modena, che sono la rappresentazione evidente dello sfruttamento lavorativo nei nostri giorni. Si tratta soprattutto di lavoratori stranieri, a cui viene imposto un ritmo di lavoro allucinante e che sono soggetti a forme di sfruttamento su cui bisognerebbe proprio intervenire. Signor Presidente, anche per i tirocini è una vergogna

saremo vicini anche in questa fase (saranno infatti essenziali l'intervento e la concertazione con il sindacato) a tutte le mobilitazioni che ci saranno nel Paese. pensiamo che il rischio più grande sia lasciare da soli i lavoratori. Abbiamo bisogno che si manifesti in modo esplicito la necessità di cura, tutela e giustizia sociale per i lavoratori di questo Paese

era prevedibile che l'ultima legge di bilancio di questa legislatura fosse utilizzata dal Governo in vista della campagna elettorale per le prossime elezioni politiche. Si tratta di una tentazione alla quale anche il Governo Gentiloni Silveri non ha saputo rinunciare. Dobbiamo riconoscere che alcuni interventi previsti in questo disegno di legge hanno soddisfatto le aspettative, soprattutto del mondo delle imprese. Dobbiamo però saper porre un distinguo tra le misure economiche necessarie al Paese e quelle che altro non sono che specchietti per le allodole che devono celare quanto l'Esecutivo non ha fatto o ha fatto male. I *bonus* possono riscuotere il favore dell'opinione pubblica, ma di certo sono parte di quelle politiche che fanno comodo al Governo per apparire nella vetrina mediatica e convincere l'opinione pubblica delle sue buone intenzioni. Ancora una volta a mancare è stata una visione d'insieme della situazione economica e sociale del Paese che, senza forzature, sia in grado di suggerire le priorità che devono essere perseguite.

(meno della metà delle risorse che servirebbero) e, di queste, circa 15 miliardi necessitano per coprire le clausole di salvaguardia per gli impegni presi con Bruxelles. In pratica, abbiamo un disegno di legge di bilancio che aumenta il debito e allontana il Paese dal pareggio di bilancio che abbiamo garantito all'Unione europea di raggiungere entro il 2019. Le indiscrezioni di stampa, tra l'altro, parlano di una possibile manovra correttiva dei conti pubblici, non inferiore a 5 miliardi di euro, da approvare in primavera. Ciò significa che dover rimettere a posto i conti che il Governo Renzi-Gentiloni ha messo fuori controllo sarà un'incombenza che spetterà ai prossimi inquilini di Palazzo Chigi. La parola d'ordine che in cinque anni ha caratterizzato l'operato di questa maggioranza è rimandare; posticipare, anno dopo anno, le decisioni più spinose per lasciare ad altri l'onere di trovare soluzioni che al trascorrere del tempo diventano sempre meno percorribili. Se analizziamo nel merito questo disegno di legge, ci accorgiamo che i tanti decantati provvedimenti a favore delle imprese vengono contraddetti ad esempio -dal differimento dell'imposta sul reddito d'impresa, la cui entrata in vigore è posticipata di un anno, al 2019: una decisione che comporterà la mancata riduzione della pressione fiscale sulle imprese, valutata in circa 2 miliardi di euro, che riguarda una platea di 250.000 beneficiari; un danno di grande rilevanza, se consideriamo che le imprese avevano pianificato le loro strategie aziendali sapendo di poter contare sull'entrata in vigore di questa disciplina, che il Governo ha praticamente scippato loro di mano. Due miliardi rappresentano una cifra enorme se raffrontiamo - ad esempio - questa manovra con il rifinanziamento della legge Sabatini, per la quale complessivamente, nel triennio 2018-2020, sono stanziati 330 milioni di euro. sono, poi, le promesse posticipate, come è accaduto per le spese di formazione del personale rientranti nel Piano industria 4.0, per le quali è stata autorizzata una spesa di 250 milioni di euro, ancora una volta a decorrere dal 2019. Sono critiche, queste, non soltanto mosse dai partiti degli schieramenti che si contrappongono alla linea di Governo, ma che arrivano direttamente da Bruxelles. Ben si potrebbe, a questo punto, introdurre subito per finanziare le agevolazioni o riduzioni fiscali alle nostre imprese. È bene rammentare che in meno di quindici giorni sono arrivati dalla Commissione europea ben due moniti. Il Vice Presidente della Commissione europea con delega alla stabilità finanziaria ha ricordato all'Italia che, con le passate manovre, ha esaurito il suo margine di azione per quanto riguarda la clausola di flessibilità per le riforme strutturali e per gli investimenti. A far riflettere, però, è il segnale di pericolo lanciato dal Vice Presidente finlandese con deleghe all'occupazione, crescita, investimenti e competitività, secondo cui i dati mostrano chiaramente che il Governo italiano ha posto una deviazione dagli obiettivi di medio termine. Soprattutto, ha testualmente dichiarato: «L'unica cosa che posso dire a mio nome è che tutti gli italiani dovrebbero sapere qual è la vera situazione economica in Italia». Senza giri di parole, il Vice Presidente della Commissione europea ha detto che il Governo italiano sta nascondendo agli italiani la scomoda verità sui conti pubblici, cioè sta mentendo ai suoi cittadini. un'accusa grave, alla quale il presidente Gentiloni Silveri risponde con un ottimismo fuori luogo, promuovendo l'idea di un'Italia che può «stare serena», poiché ormai si trova fuori dalla crisi. La nostra economia ha cominciato a farci intravedere segnali positivi, ma soltanto perché sta beneficiando degli effetti di una ripresa generale e costante che interessa tutta la zona europea. Altra cosa è dire che ci siamo lasciati la crisi alle spalle. In questa fase, è particolarmente necessario prestare attenzione a quei settori economici che faticano a ripartire e che hanno ricevuto, fino a questo momento, poca attenzione dal legislatore. Mi riferisco ai liberi professionisti, al cosiddetto popolo delle partite IVA, praticamente assenti in questo disegno di legge di bilancio; e ne è esempio la loro esclusione dal beneficio per gli investimenti riferiti a Industria 4.0. Come Direzione Italia abbiamo chiesto dei correttivi, presentando degli emendamenti, che non sono stati né accettati, né discussi. Anche i settori turismo e cultura avrebbero meritato di essere protagonisti di questa manovra; un'opportunità che avrebbe potuto trasformarsi in un'occasione per il Sud, che non ha ancora trovato la modalità per valorizzare l'immensa ricchezza culturale e paesaggistica del suo territorio. Non parliamo poi del comparto degli enti locali, ancora soffocati a scapito degli ignari cittadini da assurdi vincoli di finanza pubblica, che deprimono la spesa corrente per i servizi alle famiglie e alle categorie più deboli e bloccano gli investimenti anche agli enti virtuosi. Il Paese attende un segnale che annunci un radicale ribaltamento in termini di priorità e atteggiamenti tale da ridare credibilità alla politica. Assai poco credibile in questo contesto appare l'emendamento presentato e approvato dalla maggioranza PD che ha stanziato 6 milioni di euro in tre anni per le manifestazioni legate al carnevale. Mi appresto a concludere, signor Presidente, con una riflessione: uno Stato sano mette i propri cittadini nelle condizioni di disporre di opportunità che possono diventare la base su cui costruire un proprio percorso di vita, non di un *bonus* a tempo determinato. In questo senso, è necessario garantire ai giovani il diritto al lavoro. Ma è altresì importante insegnare loro a pensare nella maniera giusta, a camminare sulle proprie gambe e non considerare lo Stato come una stampella a cui aggrapparsi. Uno dei più grandi giornalisti italiani, Indro Montanelli, una volta disse: «Lo Stato dà un posto, l'impresa privata dà un lavoro». Non è un gioco di parole, ma è una distinzione che rappresenta il futuro, che abbiamo il dovere di raggiungere.

gli emendamenti che presentano fossero accolti. Sappiamo però perfettamente che la coperta, essendo un po' corta, accontenta qualcuno e scontenta qualcun altro.

che la salute rappresenta un bene centrale nella vita dell'individuo, per essere un cittadino a pieno titolo. Essa può assumere valore particolare in periodi di crisi economica come quello che con difficoltà stiamo cercando di lasciarci alle spalle. È proprio la crisi economica che ha fatto emergere un fenomeno come la povertà sanitaria, inimmaginabile in un Paese che ha uno dei migliori servizi sanitari nazionali: cioè persone che non possono curarsi, perché prive delle risorse economiche necessarie, che non possono acquistare i farmaci necessari né sottoporsi a esami specialistici. L'impoverimento delle famiglie a causa dei costi per la salute è una realtà sempre più rilevante nell'attuale società, così come lo è il loro indebitamento per fronteggiare i costi sanitari. È per questo che ho caldeggiato l'approvazione dell'abolizione del *superticket*. Aumentano le disuguaglianze di salute, che costituiscono una delle ingiustizie sociali più gravi. La crisi e la povertà sanitaria poi possono portare anche a una modificazione dei percorsi di cura: non si fa più prevenzione e si evitano visite e controlli medici fino a che non se ne può più fare a meno, con conseguenze sia di tipo economico sia sulle possibilità di guarigione e di gestione della malattia, a livello individuale e collettivo. La salute si mostra sempre di più come fatto sociale, oltre che biologico. Pertanto, è necessario riconoscere e studiare i fattori e gli attori esterni al mero ambito medico. È giunto il momento di riflettere su com'è cambiata l'idea di salute e di malattia, alla luce delle trasformazioni sociali in atto e dei cambiamenti epidemiologici, che vedono sempre più individui affetti da malattie croniche degenerative, che necessitano di apparati sanitari adeguati. Ciò riguarda innanzi tutto la capacità del singolo di gestire il nuovo stato di malato, in quanto la malattia sarà sempre meno una situazione straordinaria e sempre più una realtà con la quale fare i conti, specialmente per le persone anziane. Le trasformazioni in atto nel sistema sanitario, il ruolo sempre più attivo del cittadino rispetto alle scelte di cura, la presenza di malattie croniche, degenerative e rare, a partire dal cancro, ci spingono a riflettere sui nuovi temi inerenti la salute e la malattia. Sono proprio le disuguaglianze in salute a costituire una delle più rilevanti forme di ingiustizia sociale. L'aumento della speranza di vita comporta un forte interesse da parte dei decisori pubblici sulle determinanti di salute e su quali interventi mettere in atto per prevenire le malattie, a partire da quelle croniche, che attualmente rappresentano una delle maggiori sfide per la sostenibilità dei sistemi sanitari. La salute è un diritto fondamentale per l'individuo e per la collettività. Solo se l'individuo gode di buona salute potrà essere un cittadino a pieno titolo ed esercitare tutti i ruoli sociali che è chiamato a giocare nel corso della vita. una concezione della salute, quella che emerge dagli studi sociologici, in linea con la definizione fornita dall'Organizzazione mondiale della sanità,

diversi determinanti sociali». Spetta quindi alle istituzioni pubbliche declinare tale definizione in misure di politica sanitaria. È quello che io cerco di far capire da quando sono in Nel dibattito degli ultimi anni emerge anche il concetto di salute come bene comune. Secondo questa accezione, sia l'individuo che i decisori pubblici sono attori con pari dignità. La salute come bene comune è considerata un bene da perseguire mediante azioni finalizzate e sistemi di protezione che vedono al centro tutti gli individui. La salute come bene comune richiede la messa in atto di processi di informazione e anche di formazione, in vista del costituirsi di una coscienza scientifica di massa e di un alto numero di cittadini competenti in grado di dialogare e contare - anche sul terreno delle scelte prioritarie - con i soggetti istituzionali di programmazione e gestione delle azioni di politiche per la salute. Inoltre, è recente la convinzione che l'ambiente non sia semplicemente un dato, ma che esso agisca come fattore decisivo per la vita degli individui e della comunità. Questo lo dobbiamo soprattutto a un medico del lavoro, Giulio Alfredo Maccacaro, che nei primi anni Settanta ebbe un ruolo centrale nello sviluppo della sociologia della salute, focalizzando la sua ricerca sulle cause ambientali e lavorative che incidono sulla salute e la malattia dei lavoratori. Egli pone al primo posto la prevenzione, la vera prevenzione, e cioè individuare, contrastare e determinare le cause di morbosità e mortalità; ma anche lo sviluppo di gruppi all'interno dei luoghi di lavoro capaci di attivare fasi di ricerca, di studio e di lotta sulle proprie condizioni igieniche e ambientali; e infine il recupero della soggettività nel rapporto con i sanitari, il rifiuto di ogni ruolo repressivo e di controllo da parte della medicina. Ecco che assumono peso rilevante la qualità della vita e gli stili di vita e, quindi, anche l'ambiente come elemento essenziale. Spesso lo sguardo dello studente non si spingerà lungo la catena eziologica che dal malato arriva, a monte, fino alle cause delle cause della sua condizione all'interno del sistema sociale, svelandone le responsabilità, ma si fermerà ben prima di doverlo mettere in discussione. La giustizia sociale può essere insegnata, soprattutto cominciando a viverla e ad applicarla, responsabilizzando gli studenti e promuovendo un ambiente in cui si può riflettere criticamente su questioni mediche, sul ruolo sociale e politico della professione sanitaria, su come capacitare il futuro professionista ad analizzare in modo critico il ruolo che la struttura sociale che la struttura sociale ha nella determinazione della salute e nella sua disuguale distribuzione all'interno di una popolazione. Il tutto è finalizzato a più un laureato portatore di un titolo senza competenza, ma un operatore preparato e pronto a essere efficace nella realtà sociale che gli si affida. affida. Signor Vice Ministro e colleghi tutti, quello che io spero facendo questo discorso, apparentemente avulso dai temi trattati nel disegno di legge di bilancio che andremo a votare - sul quale dico sin da ora che l'Italia dei Valori esprimerà un voto che nella vostra coscienza facciate vostre queste mie riflessioni, perché ritengo che siano alla base della costruzione di una società migliore. tenere presente che in uno studio condotto in 26 Paesi dell'Unione europea, nel periodo tra il 1970 e il 2007, si è evidenziato che la crescita della disoccupazione è associata all'aumento dei suicidi e degli omicidi; crescono decisamente l'avvelenamento da alcol, le malattie psichiatriche, le cirrosi epatiche e le ulcere. Sono sempre di più le persone che si rivolgono ai «Banchi Alimentari», strutture sintomo di un'emergenza nutrizionale, che le famiglie si rivolgono a esse come ultima ed estrema risorsa. La continua crescita del prezzo del cibo fa sì che le persone riducano il consumo di frutta e verdura a favore di cibi meno costosi

tutti coloro che saranno seduti a legiferare in queste Aule, di qualsiasi estrazione politica essi saranno, dovranno mettere questi temi al primo posto nella lista dei lavori parlamentari. Spero vivamente che così facendo, nella prossima legge di bilancio, la sanità non sia trattata come un bancomat, ma sia un luogo dove investire risorse da gestire con criterio per cancellare le disuguaglianze sanitarie.

per essere probabilmente l'ultimo e più plateale esempio di assalto alla diligenza. Ci sono stati infatti soldi per tutti. Ci sono stati soldi per i partiti politici; il senatore Sposetti ci stava provando da un anno, come se non bastasse il finanziamento pubblico ai partiti,

ottenere di condonare ai cosiddetti rigassificatori l'onere di pagare l'IMU. E ciò comporterà un risparmio di circa 40 milioni di euro; quindi minori entrate per lo Stato per circa 40 milioni di euro

C'è stato persino il tentativo, molto più grave e importante, che per fortuna non è andato a buon fine, di assegnare qualche miliardo in più - come se ne avessero bisogno - ai concessionari autostradali, che hanno la concessione pubblica senza gara e che notoriamente finanziano la politica. E la concessione pubblica senza gara e il finanziamento alla politica non possono non avere un nesso di causa-effetto.

sono rimasti coinvolti, ma qual è la responsabilità della politica? La responsabilità è di chi ha gestito quelle banche. In parte, ciò è vero. Ci sono stati reati che sono in corso di accertamento da parte delle autorità: reato di aggiotaggio e di ostacolo alla vigilanza. Ma non sarebbero stati sufficienti per realizzare quello che è stato fatto. I banchieri infedeli la faranno franca, perché non è stata fatta la riforma della prescrizione in questa legislatura affinché possano farla franca.

a partire dal decreto per le banche popolari venete che ha reso impossibile per i risparmiatori truffati di adire alle vie legali per avere un risarcimento in virtù del fatto che la banca non c'è. La parte sana della banca, infatti, è stata regalata a Banca Intesa e nella cosiddetta *bad bank* non c'è nulla da aggredire. Quindi, anche se un magistrato

In passato ho visto, quando si è discusso di interventi a favore del sistema bancario, che stanziare miliardi di euro per la finanza pubblica non è mai stato un problema, anche per decine di miliardi di euro. Il solo decreto cosiddetto salva popolari venete, che in realtà non ha salvato un accidente, ha salvato il cosiddetto di tutela dei depositi e, quindi, il sistema delle banche dal tirare fuori di tasca propria entro sette giorni lavorativi, perché così prevede la legge, i 13 miliardi contenuti nei conti correnti e conti depositi. Questo sì è stato un risparmio, una conseguenza importante.

prevedete lo stanziamento di 25 milioni di euro. È lo 0,45 per cento della cifra perduta grazie al decreto sulle popolari venete.

Qualcuno dice che, comunque, è un inizio e che è stato istituito un fondo che prima non c'era. Questa è una novità rilevante. Ne prendiamo atto. I miei colleghi in Commissione ne hanno preso atto. Vice ministro Morando, ricordo però che la legge finanziaria del 2006 aveva già istituito un fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, che avrebbe potuto essere tranquillamente attivato

un fondo ben più importante di 4 miliardi di euro, ma senza pesare minimamente sulla finanza pubblica e sui conti pubblici. Presidente, noi andavamo ad attingere a una a una piccola parte di quelle risorse che in questa legislatura questa maggioranza e questo Governo hanno concesso in più al sistema bancario. Ebbene, non avete voluto farlo. Ve ne assumerete le responsabilità. Il fondo istituito, cosiddetto fondo di ristoro finanziario, è anche di difficile attuazione - come se non bastasse - perché prevede la necessità di una sentenza passata in giudicato. Mi chiedo: a chi dovrebbero far causa i risparmiatori?

Volendosi sforzare comunque, qualcosa di positivo forse lo possiamo anche trovare e dire. Cito un paio di punti. Il primo un fondo - bene o male - è stato istituito. Su di esso si potrà ulteriormente lavorare alla Camera ma, ben più probabilmente, nella prossima legislatura. ovviamente se - e solo se - cambierà questa maggioranza. Ma, se la maggioranza sarà la stessa, allora l'orientamento politico sarà lo stesso: quello di ignorare che un fondo per le vittime di crac finanziari c'era già. Lo hanno ignorato. Esiste dal 2006 e siamo nel 2017. è di ignorare, anzi votare contro quegli emendamenti che come il mio, ma non solo il mio, avrebbero potuto chiudere quel triste capitolo che ha visto la politica veramente implicata nel dramma di 210.000 famiglie. Il secondo aspetto è che questo fondo è, comunque, il riconoscimento della responsabilità della politica e, in particolare, della responsabilità della maggioranza, che ha avuto un ruolo di protagonista nell'aggravare quelle che erano le già critiche situazioni dei risparmiatori truffati nei crac bancari.

- come è notorio - con la fiducia in Senato non ci sarà possibile presentare emendamenti in Aula. E sappiamo bene che non sarà facile modificarlo alla Camera. Questo Governo, a inizio legislatura, si è dichiarato sempre, coerentemente, forte con i deboli e debole con i forti. E in questa occasione è stato coerente con se stesso. Ai più deboli, ai cittadini e ai risparmiatori truffati, a questo punto penseremo noi con il prossimo Governo, se i cittadini riterranno di darci questa responsabilità. Il fondo, signor Presidente, lo alimenteremo cancellando le decine di marchette, di regali, di condoni che avete introdotto in questa vergognosa legge di bilancio. Così, con un solo provvedimento, faremo due atti di giustizia per il Paese, per i risparmiatori e per i cittadini truffati.

Colleghi, valutato l'andamento della discussione e alla luce delle convocazioni delle Commissioni permanenti e delle Commissioni bicamerali, sospendo la seduta fino alle ore 16,30. *(La seduta, sospesa

anticipato dalla relatrice Magda Zanoni e sostenuto anche da altri colleghi, questo - e lo confermo anche nel mio intervento - è un legge di bilancio molto importante, e non solo perché è il disegno di legge di bilancio che conclude questa legislatura, ma perché agisce - e positivamente - in continuità con numerose iniziative inserite in altri strumenti legislativi e innova in molti campi. La collega Parente ha sottolineato le innovazioni intervenute in materia di politiche del lavoro e, in particolare, le iniziative rivolte ai giovani e al loro inserimento nel mondo del lavoro. Aggiungerei le importanti iniziative in campo sociale. Questa mattina la collega Bignami è intervenuta a lungo e con energia sul *caregiver*, una forte e importante iniziativa che innova un principio, quello del riconoscimento, una volta per tutte, dell'insostituibilità del lavoro di cura che viene

per gli orfani delle vittime del femminicidio e tante altre buone iniziative. Si tratta di importanti iniziative richieste e attese: penso

a riempire di contenuti per modificarla nella sostanza. Voglio poi ricordare i tanti provvedimenti fatti sugli esodati e per gli esodati, che, assieme all'APE sociale e all'inserimento

Questi interventi sono il frutto di un lavoro prezioso e importante fatto innanzitutto nel testo del Governo, ma poi dalla Commissione.

smentire il lavoro prezioso fatto nelle Commissioni, come se in quelle sedi non si fossero in alcun modo condivise e posizionate alcune questioni portate avanti anche dalle forze che oggi rappresentano l'opposizione. Negli interventi toni aspri e incattiviti, che nella Commissione francamente non abbiamo ascoltato. Credo che siano importanti e significative anche le iniziative e le proposte condivise poi dalla relatrice e dalla Commissione, che vanno a risolvere ancora ulteriori problemi delle zone che stanno vivendo vivendo il tragico *post* terremoto e la ricostruzione. Approfitto per raccontare - soprattutto alle forze politiche e agli esponenti politici dei territori che hanno più e più volte evidenziato la necessità, ovviamente condivisa anche da me, di una proroga ulteriore della sospensione delle tasse - che ieri ho dovuto affrontare un momento molto difficile nella mia città, assieme a tutti i sindaci e alle categorie produttive. È infatti pervenuta la fredda e cinica comunicazione della Commissione europea che chiede alle imprese aquilane di restituire le somme relative alle tasse sospese nel *post* 2009, a distanza di quasi dieci anni dal terremoto.

conseguenza di quegli errori, ricade oggi come una mannaia sulla testa di imprese e cittadini del cratere sismico. quindi anche in questa occasione a chi rappresenta il Governo di affiancare il lavoro che la Regione ha messo in campo assieme a tutta la rete delle imprese, perché non sia il dunque noi) a pagare gli errori di chi allora governava e non ha pensato ad adottare misure idonee e opportune che non ci facessero incorrere in infrazioni europee.

per illustrare un punto che si ricollega ad un mio emendamento molto utile e importante, che è stato oggetto di una *fake news* da parte di alcuni rappresentanti del Movimento 5 Stelle, dai quali mi aspetto una richiesta

scuola universitaria privata - ma non esistono in questo campo scuole universitarie private - e si dice ancora che questa non solo perché il contributo viene finanziato riducendo per un importo corrispondente il fondo universitario per l'università pubblica,

e che L'Aquila non è un orticello elettorale, bensì una città in estrema sofferenza che questo Governo e questo Parlamento hanno preso in carico

passa anche attraverso scelte di indirizzo che portino nelle città e nei territori colpiti dal sisma iniziative di grande profilo scientifico. Informo che in questa legge di bilancio non solo si interviene sul GSSI, ma anche su una sede del museo

garantire alle aree colpite dal sisma o da calamità naturali di avere una ricostruzione vera, non solo di case, ma anche delle identità personali, dei percorsi di lavoro e del bilancio economico. Approfitto rivolgermi al rappresentante del Governo, auspicando che al passaggio alla Camera si trovi modo di rispondere positivamente a un emendamento da me proposto, sottoscritto anche della collega Bonfrisco nonché da altri colleghi di altre forze politiche, che spinge per una soluzione relativamente alla messa in sicurezza rapida e immediata delle autostrade abruzzesi, sottoposte a un carico di violenza del movimento sismico che ne ha fatto purtroppo delle autostrade insicure. È urgente risolvere questo problema e mi auguro che

lavorato assiduamente per portare oggi in Aula questo provvedimento. Mi riferisco a tutti i componenti della Commissione bilancio, in particolare al presidente Tonini e al rappresentante del Governo, vice ministro Morando.

delle imprese voglio sottolineare alcune misure che per noi sono state fondamentali e che siamo soddisfatti siano contenute in questo provvedimento, ovvero le assunzioni dei giovani con nuovi sgravi per le imprese che assumono *under* 35, che grazie al lavoro della Commissione vengono incrementate per ricomprendere specificamente la decontribuzione per i neoassunti nelle Regioni del Mezzogiorno. Le imprese sono al centro delle misure. Segnalo anche, in particolare, quelle che riguardano il settore della pesca, a noi tanto caro, con il riconoscimento a favore dei lavoratori, anche per il prossimo anno, dell'indennità giornaliera nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto obbligatorio, obbligatorio, purtroppo previsto, e con l'incremento di risorse per il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura nel periodo che va dal 2018 al 2019. Abbiamo risorse per contrastare l'emergenza avicola, con la specifica finalità di favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva delle imprese operanti nel settore avicolo, proprio per agevolare il rafforzamento del sistema di sorveglianza e prevenzione dell'influenza aviaria e, di conseguenza, tutelare la salute umana. Sul fronte famiglia, esprimere un grande ringraziamento al Governo per aver fatto sì che nelle politiche di *welfare* il congedo previsto per le donne vittime di violenza di genere sarà allargato anche alle lavoratrici domestiche, mentre per gli orfani di femminicidio, sempre con approvazione all'unanimità da parte della Commissione bilancio, si istituisce un fondo *ad hoc* con una dotazione di 2,5 milioni di euro l'anno per il triennio.

Penso che ormai sia noto a tutti che senza Alternativa Popolare oggi, in quest'Assemblea, non parleremmo di *bonus* bebè perché, nonostante la legge del 2014 che lo ha istituito, il Consiglio dei ministri non ha poi rifinanziato la misura.

Proprio in riferimento alle coperture, nel 2018 garantiremo la copertura dell'assegno, così come previsto dalla legge istitutiva del *bonus*, ma, vista la scarsità di risorse per il 2019 e il 2020, la copertura rispetto al 2018 sarà pari al 50

consona e rispettosa nei confronti di una misura che ha iniziato a dare i suoi frutti. È ovvio che

non posso non fare un passaggio per noi importantissimo, legato alle diverse ricostruzioni giornalistiche riguardo il *bonus* bebè, che non corrispondono a quell'accordo politico e strategico sulla famiglia che in Commissione abbiamo raggiunto con il Governo. Pertanto, sono a chiedere al Governo di dare in Assemblea, ora, l'interpretazione autentica della portata della norma, per fugare completamente equivoci interpretativi che - ne siamo certi - eventualmente ci fossero, potranno essere modificati in sede di passaggio alla Camera. Per Alternativa Popolare il *bonus* bebè è una norma triennale, che vale per i primi tre anni di vita del bambino, così come era previsto dalla legge che l'ha istituito. Siamo certi che in questa sede il Governo ritenga opportuno chiarire questo punto nodale, che per noi rappresenta - lo ripetiamo - l'accordo politico strategico sulla famiglia, tema che per Alternativa Popolare rappresenta la più importante condizione per votare questa manovra.

penso che per tanti qui dentro sia arrivato il momento di finirla di raccontare frottole e di uscire dalla sfera di cristallo in cui vivono o pensano di vivere. Le condizioni in cui versa il nostro Paese, purtroppo, non sono per nulla buone, a partire - siccome l'hanno citato in tanti - dall'imbarbarimento del lavoro.

Finitela anche di dire che con le poche risorse a disposizione non si poteva fare di più, perché non è vero. Voglio ricordare che, quando avete voglia di trovare i soldi, li trovate. Avete regalato, tra *jobs act* e mancette varie, tra i 30 e i 40 miliardi di euro, che sono soldi pubblici, della gente, senza che essa ricevesse nulla in cambio dai padroni, nemmeno in tema occupazionale (poi vi dirò perché), tant'è vero che la disoccupazione giovanile è attestata al 35,5 per cento: altro che risorse per i giovani! I giovani scappano da questo Paese, perché hanno un lavoro sottopagato,

Solo per dare i dati e per leggerli correttamente (non come fate voi), l'occupazione giovanile è tra i 17 e i 20 punti sotto la media europea e - voglio ricordarlo - voi siete al Governo da cinque anni. Voi, in questo provvedimento, proponete praticamente le stesse cose, sulla scia di *jobs act*, *bonus*, tirocini: soldi a pioggia senza chiedere nulla in cambio. Anzi, aggiungete qualcosa, ancora più triste, su quella scia, che è l'alternanza scuola-lavoro. Spieghiamo, a chi ci ascolta, cosa prevede veramente l'alternanza scuola-lavoro. Riguarderà un milione e mezzo di ragazzi, che dovranno svolgere lavoro gratis, pari a 500 milioni di ore di lavoro, in aziende scelte e senza nessun controllo, tant'è vero che quando emergono le nefandezze è perché sono gli studenti che hanno il coraggio di denunciarle o di manifestare, quindi controlli non ce ne sono.

dopo che avrà lavorato gratis e fuori tema, le aziende avranno l'obbligo di assumere questo lavoratore? Non l'ho visto scritto da nessuna parte. Altro che misure per i giovani! I dati ISTAT bisogna avere il coraggio di leggerli, non di interpretarli a vostro piacimento. Dite che la disoccupazione è scesa grazie al *jobs act* e

chiunque in una settimana abbia lavorato almeno un'ora viene considerato occupato. Questo è per voi l'occupazione

la somma aggiuntiva che prevedete dal 2020. Noi abbiamo osservato che i migliori analisti avevano detto che per far fronte alla povertà in aumento nel nostro Paese, al di là di quello che dite voi, come afferma anche l'ISTAT, servirebbero almeno 7 miliardi di euro; voi avete investito investito la settima parte di 7 miliardi. Adesso, dopo varie insistenze dell'opposizione, dite di aggiungere - se non sbaglio - 400 milioni, che non sono bazzecole (io non scherzo mai sui soldi).

Vorrei fare un'ultima considerazione anche sull'aumento dell'età pensionabile, perché anche su questo, secondo me, parlate a sproposito e continuate a dire inesattezze (voglio essere buono su questo).

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, Governo, dovendo condensare in poche parole e nel tempo di cinque minuti una valutazione complessiva su questo disegno di legge di bilancio, cercherò di dire quelli che mi paiono essere gli elementi salienti che lo connotano. Questo è un provvedimento in qualche modo si colloca in un solco di continuità rispetto alle molte iniziative che i Governi di questi anni hanno intrapreso per intercettare l'esigenza di rilanciare la crescita del Paese e di rimettere in moto le dinamiche di occupazione

i dati che escono in sequenza ormai confermano ogni volta che il *trend* della crescita c'è e che anche sul fronte dell'occupazione ci sono segnali importanti. Insieme a questo - lo sottolineo perché mi pare un elemento politico molto rilevante - questa manovra introduce un segnale certamente non ancora sufficiente, ma dà un'indicazione di forte curvatura verso la domanda di protezione, di contrasto alla povertà, di specificazione nell'incoraggiamento delle dinamiche occupazionali verso i giovani e verso il Mezzogiorno e attraverso i provvedimenti che riguardano la famiglia e l'avvio del superamento del *superticket*. Insomma, questo è un disegno di legge che si colloca, da un lato, nel solco di una continuità positiva, e dall'altro, introduce innovazioni politicamente rilevanti. Lo voglio dire anche con un po' di rammarico perché, pur ovviamente con le sue imperfezioni - e anche con quelle che possono essere ritenute da altre componenti di questo Parlamento le sue inadeguatezze

che segna per la prima volta un'attenzione molto importante - che io credo rappresenti un segnale politico - nel tentativo di riconquistare attenzione e fiducia

sia il tratto distintivo maggiore di questo importante provvedimento. Ho sentito in alcuni interventi fare riferimento - ed è una questione vera - a taluni aspetti e cascami che una legge complessa come questa, che deve essere portata avanti nel contesto di una maggioranza complicata, porta con sé. Qualcuno li chiama mance, qualcun altro usa modi più coloriti. Tutto questo è vero. Parlando con qualche collega stamattina dicevo, per esempio - so che probabilmente non incontrerò il consenso delle colleghe e dei colleghi - che la legge di bilancio in realtà dovrebbe essere la legge in cui più secco è il rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo e in cui l'attività emendativa dovrebbe essere limitata a pochissime grandi questioni. Dopodiché, la rincorsa alle mance - io ho partecipato anche alla seduta notturna, se così la vogliamo chiamare, di ieri - in qualche modo diventa fisiologica in questo contesto e in qualche misura ci rende anche molto più simili

però naturalmente contraddistingue una parte decisamente minoritaria complessivamente del disegno di legge, credo che stiamo per licenziare qui al Senato un buon provvedimento che mi auguro alla Camera possa essere ancora migliorato.

Sottosegretario, che sono rimaste aperte e che io seguo da parecchio tempo. La prima riguarda il destino dei lavoratori del settore delle autostrade di questo Paese, che in questi giorni stanno lottando per difendere il posto di lavoro; ieri in Commissione c'è stata un'importante presa di posizione del vice ministro Morando, che poi non è potuta arrivare a compimento non c'erano le condizioni numeriche per farla approdare in un emendamento e io credo che la questione vada ripresa perché sono in gioco i posti di lavoro di migliaia di persone e condizioni di vita di migliaia di famiglie che vanno guardate con attenzione. La seconda questione riguarda il tema dell'amianto. Ringrazio il senatore Santini per

solo ricordare, tuttavia, che proprio nel fine settimana scorso si è svolta a Casale Monferrato, che è la città tragicamente simbolo della vicenda "amianto", una importante conferenza promossa dal Governo, sul tema

per l'attività di costituzione in parte civile, occorrono risposte più solide, le stesse che il Governo si è impegnato ad assumere non più di qualche giorno fa e che mi auguro nel passaggio alla Camera, per impulso del Governo, possano essere meglio

una legislatura da dimenticare, che ha portato il Paese sull'orlo del baratro sia dal punto di vista economico, che dal punto di vista finanziario. Una legislatura caratterizzata da tradimenti e bugie: sono stati traditi tanti elettori che avevano votato i loro rappresentanti per far parte di uno schieramento e nel corso della legislatura se li sono ritrovati nell'altro. Tradimenti che hanno consentito a tre Presidenti del Consiglio di avvicendarsi, ma nessuno, finita la legislatura, li rimpiangerà. Nel corso di questi anni, i vari Governi hanno tentato, attraverso varie bugie, di tranquillizzare i cittadini, ma nel Paese si è concretizzato un sentimento diffuso di protesta e di reazione che esploderà nella prossima primavera, alle elezioni. Faccio un esempio. Il ministro Padoan ha rilasciato nei giorni scorsi un'intervista al quotidiano «la Repubblica» sulla situazione economica italiana, affermato che il debito pubblico ha smesso di crescere, ci sono un milione di occupati in più e la fiducia delle imprese e delle famiglie è molto più solida. Tre affermazioni completamente prive di fondamento. Se guardiamo in termini assoluti, il debito pubblico in realtà sta crescendo costantemente e da settembre ha raggiunto il valore di 2.284 miliardi di euro. Guardando nel lungo periodo, a partire dal Governo Monti, da quando cioè ha lasciato il presidente Berlusconi, il debito pubblico era di 1.906 miliardi ed è cresciuto di 378 miliardi. Anche se andassimo a guardare il breve periodo, nei primi sette mesi del 2017, il debito pubblico è aumentato complessivamente di 82 miliardi di euro. Un dato in linea con lo stesso periodo del 2016, quando è aumentato di 83 miliardi, ma nettamente superiore a quello del 2015, quando il debito pubblico era cresciuto di soli 64 miliardi. È evidente che nei documenti di programmazione economica il Governo ha fatto previsioni molto ottimistiche e alla fine i conti non sono tornati e ciò ha generato debito pubblico, che continua a crescere.

Siamo andati a vedere, ma non è così. L'Eurostat riporta una percentuale del debito pubblico italiano in rapporto al PIL pari al 134,7 per cento nel secondo trimestre 2017; in crescita rispetto al 134 per cento del primo trimestre

purtroppo evidente che questo rapporto non può diminuire perché non cresce il PIL, ovvero la crescita del PIL non è corrispondentemente adeguata alla

Il calo del PIL obiettivamente è stato molto forte in Italia anche rispetto alla media europea che ha seguito la crisi. Oggi siamo al -7 per cento rispetto al livello massimo del periodo precedente

Purtroppo, dalla crisi ad oggi, in Italia si sono persi 955.000 posti di lavoro. Vero è che nell'ultimo periodo un po' di posti di lavoro sono stati recuperati. Ai cittadini dobbiamo però raccontare tutta Nelle statistiche ISTAT viene considerato occupato anche chi ha svolto una sola ora di lavoro nella settimana di riferimento della rilevazione. Per avere un dato più certo e vero, vi dico che il totale delle ore lavorate è ancora molto lontano dal livello pre-crisi e siamo a ben 680 milioni di ore in meno lavorate. Ciò sta a significare che i nuovi posti di lavoro recuperati sono, perlopiù*, part-time* e, se andiamo a guardare i dati ISTAT, nel 2016 i lavoratori *standard* a tempo pieno rispetto al 2008 sono diminuiti di un milione, mentre quelli a tempo parziale sono cresciuti di 789.000 unità. È vero, quindi, che la quantità dei lavoratori è tornata a livelli pre-crisi, ma è cambiata la composizione dei contratti, con un aumento di quelli *part-time* e un calo di quelli a tempo pieno. Un altro dato che ci consente di vedere come sta andando l'occupazione in Italia è il parametro «unità di lavoro equivalenti a tempo pieno». Dal 2008 abbiamo perso 1,2 milioni di unità di lavoro equivalenti ed è questo il dato che dobbiamo considerare per quantificare l'apporto vero del fattore produzione nella realizzazione del PIL. Se in Italia non c'è lavoro, gli italiani se ne vanno all'estero. Nell'anno 2016 sono 124.000 gli italiani che hanno lasciato l'Italia e sono andati a cercare fortuna nel resto del mondo. Principalmente sono andati in Gran Bretagna e Germania. Di questi 194.000, ben 70.000 sono giovani forniti di laurea e diploma. Ciò determina un impoverimento del Paese anche dal punto di vista intellettuale. Perdiamo anche commercianti, artigiani e professionisti. Dal 2008 ne abbiamo persi 514.000 e il dato è in peggioramento perché nel secondo semestre 2017 la diminuzione del numero dei lavoratori autonomi è stata di 84.000 unità. C'è poi da raccogliere il grido di allarme sulle nascite. In Italia non nasce più nessuno. Proprio ieri l'ISTAT faceva presente che i nati nel 2016 sono 473.000. Le nascite sono diminuite di oltre 100.000 unità negli ultimi otto anni e a farne le spese sono le coppie con entrambi i genitori italiani.

185 milioni di euro, meno di 200 euro a famiglia. Non so cosa ci faranno questi poveri con 200 euro all'anno. Sorvolo sulla fiducia, che è diminuita sia tra le imprese che tra le famiglie e chiudo dicendo che, rispetto a questi problemi che ho elencato, la legge di bilancio fa acqua da tutte le parti. Innanzitutto non ci sono più le risorse. Avete bruciato tutte le possibilità che aveva il Paese. Fate una manovra finanziaria in debito: altri 12 miliardi di euro di debito, cosa che è veramente criminale.

I 20 miliardi che abbiamo in bilancio servono per coprire le clausole di salvaguardia. Scongiuriamo l'aumento dell'IVA nel 2018, ma lo spostiamo al 2019, così se lo ritroverà il nuovo Governo.

Voi avete bruciato le risorse anche della prossima legislatura. Concludo riferendo che anche i lavori in Commissione sono stati vergognosi caratterizzati da confusione, ricatti, decine di fascicoli di accantonamenti ingiustificabili e di mance che fanno vergogna nella condizione disastrosa nella quale si trova l'Italia. Questa è una legge di bilancio da irresponsabili. Nulla per il terremoto. Nulla per i Comuni. Nulla per le Province. Per queste ragioni il nostro giudizio, signor Presidente, è fortemente negativo e fortemente critico e auspichiamo che questa situazione possa finire nel più breve tempo possibile.

sia caratterizzata da importantissimi provvedimenti in essa contenuti, che mirano a dare risposte a questioni economiche ma anche a problemi che investono le nostre famiglie nel quotidiano e che, quindi, sia un provvedimento di grande valenza sociale. Vorrei sottolineare la significatività del fondo destinato alle persone che assistono i malati in casa (i cosiddetti *caregiver*), siano essi familiari (fino al secondo grado oppure al terzo grado nel caso di invalidi non autosufficienti titolari di indennità di accompagnamento), coniugi, *partner* di unioni civili o conviventi di fatto. La copertura finanziaria non è stata debole: si tratta di 60 milioni di euro nel triennio. Un primo importante passo verso il riconoscimento di un'opera assistenziale meritoria, fatta da tante persone "invisibili" che assistono i propri cari

il reddito di inclusione) in questa legge di bilancio. Va sottolineato l'aspetto estensivo della tutela che riguarda l'assegno mensile destinato alle famiglie che ne fanno richiesta entro novanta giorni dalla nascita di un figlio o di ingresso in famiglia di un figlio adottato o in affido preadottivo, dove l'ISEE non superi i 25.000 Ma altre misure sono state veramente buone ed è menzognero quanto detto poco fa: che non è stato fatto niente per le Regioni colpite dal terremoto. Vorrei soffermarmi proprio sull'aspetto dell'introduzione delle zone economiche speciali per le aree del Mezzogiorno e per quelle colpite da fenomeni Sono una sostenitrice di questo strumento, già sperimentato e consolidato in altri Paesi dell'Unione. Io lo reputo utilissimo. Tuttavia, avrei anche in questo caso auspicato una applicazione estensiva di questa modalità anche per quelle aree non necessariamente colpite da emergenze, ma comunque depresse, che vivono in situazioni difficili che comportano un freno alla crescita, allo sviluppo e al rilancio a causa della disparità che subiscono sul fronte della competitività con i paesi contermini.

Passando ad altro tema, nutro un auspicio per un altro emendamento che riguarda le misure previdenziali per i lavoratori che hanno prestato la loro attività in processi produttivi legati all'amianto, argomento di cui prima parlava il senatore Borioli, nei Comuni che presentano un tasso di mortalità per patologie asbesto correlate significativamente

che la scuola sta attraversando e con riferimento alla rivoluzione tecnologica e multimediale, che va governata. I processi di cambiamento vanno governati e non subiti, visti e considerati i rischi devastanti

una situazione sempre più insostenibile, che non si concretizza più in emigrazione interna tra nord e sud del Paese, ma in migliaia di giovani talenti, per lo più laureati, costretti ad andare all'estero per avere un lavoro, una dignità e una qualità della vita, che in Italia diventa sempre più difficilmente raggiungibile. In questi anni riteniamo di aver imparato alcune cose; perlomeno abbiamo verificato che ai rappresentanti di questa maggioranza mancano la capacità e la reale volontà di perseguire le migliori soluzioni. Diversamente dal Movimento 5 Stelle, la maggioranza ha dimostrato di non voler costruire e perseguire quotidianamente, a piccoli passi, il cambiamento. Parlate di sviluppo, di obiettivi, di progresso, ma votate per conservare lo *status quo*, cioè il presente, per tutelare ancora il più forte, per difendere il grande capitale. una pratica che avete applicato in tutti i settori: bancario - bancario - lavorativo e industriale. Dalla parte della domanda e dell'offerta, da quella del produttore o del consumatore, guai a chi tocca il grande capitale speculativo e gli oligopoli, anche se essi distruggono risorse naturali, insidiano Il tema dell'utilizzo e dello sfruttamento delle risorse naturali non trova sufficiente spazio nelle discussioni politiche, figuriamoci nella legge di bilancio.

sarebbe stato un forte stimolo alla creazione di nuovi posti di lavoro, alla crescita dell'economia. Insomma, sarebbero state finalmente misure strutturali di sostegno alla collettività, indirizzando il nostro sistema produttivo verso la *green economy*, l'economia circolare e la decarbonizzazione. Al contrario, siamo invece costretti a constatare che le attività dannose per l'ambiente e la salute, anziché essere adeguatamente penalizzate, sono destinatarie di semplificazioni normative e sussidi da parte dello Stato: sono pari a 18 miliardi di euro i SAD (sussidi ambientalmente dannosi) in Italia e non lo diciamo certo solo noi. Secondo il Fondo monetario internazionale, l'eliminazione dei sussidi al settore energetico a livello mondiale farebbe aumentare il gettito degli Stati di 2.900 miliardi di dollari cento del PIL mondiale), riducendo le emissioni di CO2 del 20 per cento. Tra le proposte del Movimento avete respinto anche quella con la quale innalzavamo dal 50 al 100 per cento della quota del fondo sulle quote delle emissioni per la realizzazione di interventi di risparmio, efficienza e produzione di energia rinnovabile, attualmente utilizzata per coprire il debito, appunto, al 50 Avete invece approvato l'ennesimo favore per i grandi gruppi che operano nel settore energetico delle fonti fossili con gravi ripercussioni sui bilanci dei Comuni di Livorno e di Rovigo: con l'approvazione dell'emendamento 63.4 (testo 4), a la riduzione dell'IMU ai manufatti ubicati nel mare territoriale destinati ad attività di rigassificatori del gas naturale liquefatto. E sarebbe questo il vostro Green Act, tanto pomposamente annunciato, ma mai realizzato? Vi ricordiamo che al rigassificatore OLT di Livorno, in buona parte sottoutilizzato, viene già riconosciuto il cosiddetto fattore di garanzia, pagato attraverso le bollette energetiche per vent'anni. Ogni anno, per vent'anni, paghiamo un sussidio a questi impianti per garantire loro una remunerazione del 70 per cento anche se non svolgono attività. È un emendamento che riteniamo inappropriato e antisociale che metterà sicuramente in difficoltà i bilanci dei comuni di Livorno

le competenze ai rifiuti. È un'operazione inutile, architettata a nostro avviso per due obiettivi: la necessità di sistemare altri due incarichi a 240.000 euro all'anno (a fronte di un incremento di solo 25 unità del personale impiegato) e quella di raggiungere meglio un accomodamento politico che possa escludere il Movimento 5 Stelle da qualsiasi ragionamento sulla nuova composizione del collegio dell'Autorità, che per i prossimi sette anni dovrà occuparsi della regolazione dei settori strategici dell'acqua, dell'energia e dei rifiuti. Noi ci siamo non solo pronunciati contro, ma abbiamo altresì chiesto di prorogare i termini del rinnovo del collegio sino alla prossima legislatura, affinché la nomina sia coerente con la composizione parlamentare che gli elettori decideranno di esprimere con le urne e non abbia nulla a che fare con questo Parlamento ormai al capolinea. In questo provvedimento, inoltre, non si provvede, venendo meno agli impegni più volte assunti dal Governo in ambito parlamentare, a stabilizzare per più anni le detrazioni fiscali per l'efficienza energetica e la ristrutturazione edilizia. Nonostante l'assoluta necessità di intervenire, non si vuole investire per lo sviluppo industriale delle esperienze più innovative che operano nell'ambito della *green economy* e in quello della decarbonizzazione e che vengono invece ostacolate dall'assenza di politiche energetiche e climatiche efficaci, anche con riguardo agli obiettivi europei e internazionali che il Paese deve raggiungere. Inoltre, con le continue modifiche del quadro regolatorio (riforma delle tariffe domestiche e non domestiche, spalma-incentivi, sistemi di distribuzione chiusi, ecobonus, eccetera) e l'incertezza dell'applicazione normativa, sia dal lato dell'offerta di energia, escludendo la partecipazione delle fonti rinnovabili al mercato elettrico, attraverso i servizi di dispacciamento, sia dal lato della domanda, disincentivando il cosiddetto *demand response*, gli aggregatori e il V2G, si vuole conservare il vecchio modello energetico fondato sulla produzione centralizzata con fonti fossili. Ricordo a voi e soprattutto ai cittadini che dal 2014 ad oggi, in Italia, la produzione elettrica da rinnovabili è calata

Questo continuo peggioramento è confermato anche nei primi sette mesi di quest'anno, con una riduzione ulteriore delle rinnovabili di 3,5 terawattora e un aumento delle fossili di 10

Nel 2011, nel settore delle rinnovabili vi erano 140.000 occupati diretti; nel 2016, grazie alle vostre politiche, ne abbiamo solamente 24.000. Ve lo chiedo nuovamente: è questo il vostro *Green Act*? È paradossale che un settore industriale e innovativo come quello delle rinnovabili, anziché crescere, abbia perso oltre 120.000 posti di lavoro in cinque anni e abbia visto un calo degli investimenti di 30 miliardi: una perdita devastante per un settore invece strategico e fondamentale per reggere la competitività internazionale, la crescita e e lo sviluppo economico del Paese. La migliore conferma di quanto dico la trovate nella politica di decine di Paesi esteri, che stanno invece perseguendo questa strada. Non condividiamo, altresì, la riduzione della detrazione dal 65 al 50 per cento per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre, di infissi, di schermature solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, compromettendo così gli aspetti positivi che tali benefici fiscali hanno avuto negli ultimi anni su settori trainanti dell'economia nazionale e rischiando di creare paradossalmente effetti distorsivi di mercato. Per il Movimento 5 Stelle era necessario individuare, tramite questo provvedimento, un piano per l'impiego delle nuove tecnologie, al fine di decarbonizzare il settore produttivo e rendere l'Italia indipendente dalle fossili entro il 2050. A tale scopo sarebbe stato prioritario rafforzare e intraprendere misure per intervenire sugli edifici civili e industriali, con interventi di efficienza energetica, risparmio e autoconsumo e con l'utilizzo di fonti rinnovabili. Bisognava altresì favorire la mobilità elettrica, che vede l'Italia fanalino di coda con l'immatricolazione di soli 2.000 veicoli all'anno (10

su tanti aspetti tecnologici, con tanti giovani che devono andare a lavorare all'estero e che trovano collocazione all'estero proprio in questi settori innovativi, lasciando a noi italiani solo l'onere di aver pagato i loro studi, ma ad altri i benefici di godere delle loro intelligenze. Evidentemente l'importante per voi, però, è non toccare il grande capitale speculativo, non toccare i privilegi costituiti, lo *status quo* e rimanere casta fra le caste. Noi ci opporremo.

questione piccola rispetto alle altre che abbiamo discusso, ma qualitativamente interessante ed emblematica perché, a modo suo, l'AFAM è un piccolo riassunto dell'Italia di oggi. di un settore fatto di eccellenze storiche, ma anche di istituti che fanno fatica a sopravvivere; è fatto di forti identità, ma anche di autoreferenzialità esasperate; è fatto di grandi esigenze di riforme di organizzazione e di ritardi decennali, quasi ventennali, nell'attuazione; è fatto di ampie sacche di precariato e di marginalità del comparto rispetto alla grande questione della scuola. In questo comparto oggi noi possiamo portare due risultati acquisiti dalla discussione in Commissione: un emendamento con il quale fissiamo l'obiettivo della statizzazione di tutti gli istituti ex pareggiati (statizzazione che si può fare in tre anni sostituendo i Comuni che non ce la fanno più a reggerli); inoltre, stanziamo risorse congrue, del MIUR e del MEF, che garantiranno nei tre anni la statizzazione. Quindi non una partita di giro, ma risorse concrete nuove. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, di tutti i Gruppi. Vorrei ringraziare, ovviamente, i Ministeri dell'istruzione e dell'economia, il vice ministro Morando, che ha dato una mano, rappresentanti del Governo e, se mi consentite, soprattutto il mio Gruppo in 7a Commissione, il presidente Marcucci e la capogruppo Elena Ferrara, con i quali abbiamo condiviso con determinazione questo risultato, che non è stato facile né scontato, se pensiamo che da molti anni ci si lavorava senza arrivarci. Vorrei fare due commenti a questo risultato. Il primo è che noi avevamo ambizioni più vaste di quelle che abbiamo raggiunto. Volevamo delineare un percorso per la statizzazione, che vi fossero cioè criteri e modi condivisi. Non c'è stato e il testo è molto stringato. Adesso l'iniziativa sarà del Ministero, che naturalmente ha anche molte altre emergenze e incombenze, e mi auguro che riusciremo a trovare il modo di sostenere il suo sforzo. Il secondo obiettivo era collegare la statizzazione con l'avvio di un riordino dell'intero sistema; obiettivo indispensabile, perché non si può pensare - ed è stato un grande equivoco - che la riorganizzazione fosse soltanto un prezzo chiesto dal MEF per poter finanziare la statizzazione. Non è così, perché è un'esigenza assoluta. Lo dico qui con una frase molto semplice: l'AFAM non vivrà se non si riorganizzerà; rischia di crollare su se stessa se non sapremo innovare e anche riorganizzare l'offerta formativa. Il terzo obiettivo era iniziare a sanare il grande tema del precariato, con coloro che partecipano alla graduatoria della legge n. 128 del 2013, coloro che lavorano da tre anni e i maestri di seconda fascia.

Io credo che si possa intanto vedere se alla Camera il tema possa essere riaperto e in ogni caso, se la soluzione è il regolamento, ora più che mai esso è indispensabile. Il secondo commento è che noi, approvando questo emendamento e ottenendo questi risultati, non abbiamo tagliato il traguardo, né della statizzazione, né del rilancio dell'AFAM. Siamo appena Siamo appena partiti, ed è importantissimo averlo fatto, ma non possiamo ora dimenticare che abbiamo dei compiti immediati davanti a noi. Il primo è avviare bene la statizzazione. Vorrei dire al Ministero dell'istruzione, che avrà il compito di gestire questa fase, di fare tesoro di quanto elaborato in tutti questi anni di lavoro, nei quali abbiamo costruito l'ipotesi di statizzazione senza buttare a mare un lavoro di proposte e anche un clima di concordia che abbiamo costruito attorno a questo obiettivo: arrivarci in tre anni, sgravare i Comuni progressivamente, statizzare tutti insieme, non procedere per assorbimento ma valorizzando le identità. Il secondo compito è impostare un riordino organico, profondo, coraggioso: nessuno pensi che, arrivate queste risorse supplementari, possiamo continuare a lavorare come se niente fosse. io vedo tre filoni di lavoro davanti a noi: una nuova rete territoriale che potremmo sperimentare intanto nella musica;

tema del precariato, dobbiamo assolutamente dare risposta ai lavoratori che attendono di uscire da questa situazione. Ci sarà bisogno di molto lavoro e spirito innovativo il Governo e la politica facciano la loro parte. Diciotto anni di lentezze devono essere ora superati e occorre che anche il settore faccia la sua parte: ci sono state e ci sono troppe divisioni, troppe paure e troppe chiusure. Non è chiudendosi che nascerà l'AFAM dell'eccellenza che tutti noi vogliamo. *(Applausi

Bisogna però dire che il Governo Gentiloni Silveri-Padoan ha lavorato in condizioni difficili, perché, come tutti capiamo, questa è una manovra finanziaria in campagna elettorale.

ha spesso detto di essere abbastanza critico nei confronti dell'Europa e ha ricevuto la Le Pen e anche dei gruppi tedeschi che sono di estrema destra, molto contrari Il presidente Berlusconi è stato fulminato dalla Merkel dopo i dissidi di un tempo e vuole fare una politica di questo genere. Il Movimento 5 Stelle aveva parlato di un *referendum* sull'euro;

sul cosiddetto Italicum. Infatti, i conti dello Stato non sono assolutamente in ordine.

Vorrei ricordare che in Italia non gravano imposte progressive sul patrimonio, mentre si tassano - e troppo - il lavoro, gli stipendi e i consumi. In questo modo le riduzioni che si vantano scontentano persino le categorie che ne fruiscono. Vi faccio un solo esempio: la tassazione delle società, quella sì, è diminuita dal 27,5 al 24 per cento; ma si tratta di un calo che è stato compensato abolendo la riduzione per le aziende che investivano tanto, alla faccia dei contributi alle imprese innovative che vogliono costruire il futuro. Secondo esempio: i tagli ai contributi degli enti locali costringono gli stessi enti locali ad aumentare le loro imposte; quindi, anche modeste riduzioni a livello nazionale delle imposte per noi normali (per noi che non siamo

tutela essenzialmente dalla nostra cattiva politica. Ma naturalmente siamo sotto elezioni e domani i giornali saranno pieni di tutte le marchette che singoli senatori hanno introdotto

cose brevissime su un mio emendamento, che invece era *erga omnes*, nell'interesse del Paese: avevo chiesto di stabilizzare i ricercatori precari

permette l'assunzione forse di un migliaio di persone, creando però altre divisioni nella categoria e una discrezionalità che può essere molto pericolosa.

abbiamo una sanità che protegge davvero in caso di malattie gravi. Questo è assolutamente vero, ma il punto, cara Ministra, è che se, a livello del popolo, si paga troppo per il contributo sanitario pubblico, questo creerà una delegittimazione del Servizio sanitario nazionale, che prima o poi renderà non praticabili e non fruibili neanche le cure essenziali in caso di tumori o di malattie molto gravi. Altra questione riguarda il *bonus* bebè. Ho sentito la collega Vicari di Alternativa Popolare che se ne vantava; ma, collega, si tratta di una mancia: 40 euro a regime. In altri Paesi, la vicina Francia, un bambino che nasce ha dei diritti: ha il diritto a una piccola somma che lo Stato elargisce; ha diritto, se la sua famiglia non è abbiente, alla *crèche*, cioè all'asilo nido; ha diritto alla *maternelle*, che scatta dai tre anni e a una serie di altri contributi per la scuola, per la sua formazione e per le famiglie. Ma la Francia è un Paese molto distante. Sul piano delle imposte, ad esempio, in Francia non si vergognano, come vi vergognate tutti voi, a imporre imposte sul patrimonio. Ad esempio, si paga la tassa sulla prima casa e non solo; in caso di divorzio, il passaggio di una quota della proprietà della casa al coniuge viene tassato nella misura del 2,5 per cento: nel caso di un patrimonio di 500.000 euro sono 2.500 per 5 (fate il conto) di tasse che si pagano allo Stato. Ancora, se vi è un investitore straniero (io abito a Roma in una proprietà di una società spagnola), la *plus-value*, cioè il nuovo valore che la casa assume dal momento dell'acquisto al momento della vendita, viene tassato al 30 Cari colleghi, sappiamo tutti che le tasse non sono bellissime, come ebbe a dire il povero Padoa-Schioppa, ma, intanto, se le pagassimo tutti (se quel 20 per cento che ha il 70 per cento della ricchezza le pagasse), sarebbero meno pesanti; e poi, senza affrontare questi nodi e senza dire la verità alle persone, dove si trovano i soldi per le vostre promesse elettorali? Io vi dico che in ogni caso è bruttissimo;

parli la lingua della verità, che non accetti queste logiche populistiche, demagogiche e sostanzialmente ingannatorie.

Vorrei dunque esprimere inizialmente soddisfazione per i risultati ottenuti per il collegio estero. presentato un emendamento che dava risposte con pochi fondi alle varie istituzioni di rappresentanza degli italiani all'estero, al personale a contratto nei nei nostri consolati, alla diffusione della lingua e cultura italiana, alla stampa italiana all'estero, alle camere di commercio e alle agenzie di informazione; tutto questo per la modesta somma

l'autorizzazione a un concorso per 150 impiegati di ruolo al Ministero degli affari esteri, finanziato non con i fondi del disegno di legge di con l'applicazione del concetto della *spending review*, che faceva riferimento - se ricordiamo il titolo di quell'emendamento - alla riduzione della spesa in invarianza dei servizi. Qualche anno fa avevamo già sollevato il problema dei costi eccessivi dell'indennizzo delle sedi estere per i nostri diplomatici; questa volta, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri, si finanza l'assunzione di 150 persone riducendo quelle spese.

Molti di voi, colleghe e colleghi, mi hanno chiesto cosa prevede l'emendamento 102.0.1, perché avete ricevuto moltissime *e-mail* di protesta contro di esso. Questo emendamento

una cosa allucinante. Solo il nostro Paese permette una cosa del genere. Questo ha creato, soprattutto in America Latina, un vero commercio sulla nostra cittadinanza.

Abbiamo tentato e tenteremo, finché avremo fiato, di moralizzare e sanare questa situazione.

fino al nonno). Questo è il primo attentato. Il secondo attentato è che abbiamo detto che sarebbe opportuno che la persona che riceve la cittadinanza italiana sia in grado di dire «buongiorno» in italiano al console che gli consegna il passaporto.

noi avevamo proposto di portarla a 400 euro. In alcuni Paesi, Presidente, la tassa di soggiorno per lavorare in quel Paese costa molto più di 400 euro

voi avete avuto il disturbo delle varie *mail* che avete ricevuto, allora vi dico che questa era un'operazione di moralizzazione:

Questa proposta viene da persone che vivono all'estero, perché noi abbiamo il senso e il rispetto del valore della cittadinanza, cosa che non riscontriamo sempre sul territorio nazionale. Questo abbiamo proposto, è per questo che siete stati disturbati e per questo noi siamo stati accusati di tentare un *golpe* da una forza politica presente in quest'Aula che, tra i suoi dirigenti, ha un signore che, nei documenti di richiesta di arresto del senatore Di Girolamo, figura almeno quattro volte.

il senatore Di Biagio che hanno sostenuto questo lavoro fino all'ultimo. Non ci siamo riusciti, ma penso che stavamo facendo il nostro dovere di senatori della Repubblica e non di rappresentanti di interessi particolari, come invece credo abbiano fatto molti nostri colleghi dell'America Latina. PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cioffi. Ne ha facoltà.

Con loro ieri ci siamo intrattenuti fino alle cinque di mattina per rimanere sempre sul punto, per cercare sempre di stare attenti e di combattere tutte le cose che sono arrivate in Commissione. Questa legge di bilancio è stata un continuo assalto alla diligenza, in cui ci sono state molte marchette e molte regalie, che in fin dei conti non facevano altro che perpetuare lo *status quo*, come è stato già detto da altri componenti del mio Gruppo. È una politica triste, in cui sembra che tutto possa cambiare, ma poi alla fine non cambia mai niente. D'altra parte, le dichiarazioni di Eugenio Scalfari, che dice che preferirebbe allearsi con Berlusconi piuttosto che considerare il Movimento 5 Stelle, sono

in questo marasma di conservatori di destra e di sinistra. Noi siamo entrati in Parlamento per cercare di dire che questo sistema conservatore non ha più senso, non ha più ragione esistere: noi abbiamo il coraggio di cambiare realmente, di lavorare per l'interesse dei cittadini. Siamo stati, in questi ormai cinque anni, a combattere punto su punto, a evidenziare tutte le schifezze che sono state fatte in questo Parlamento, spesso in combutta tra i due presunti nemici, che sono sempre stati amici (questo lo ricordiamo tutti quanti). Che cosa abbiamo fatto con riferimento a questa legge di bilancio? Abbiamo presentato 400 emendamenti, che non sono tanti, considerando che gli articoli erano 119, e abbiamo visto ieri cose stranissime: abbiamo osservato che il Governo dava parere favorevole a

che è la decima società al mondo per capitalizzazione e che vale alla borsa 355 miliardi di dollari, che non può pagare 60 milioni di euro l'anno per l'IMU e quindi ridistribuire ai cittadini

Una riguarda l'emergenza abitativa ed è assurdo che questo non sia uno dei temi centrali. Abbiamo letto dai dati forniti da Federcasa che l'Italia risulta agli ultimi posti nelle classifiche europee per percentuale di alloggi sociali, con circa il 5 per cento contro una media del 25 per cento

a chi devono essere assegnati questi alloggi, perché abbiamo visto quello che è successo con le analisi che abbiamo fatto al Comune di Roma, da cui si è evidenziato che ci sono persone che vivono negli alloggi popolari e che magari hanno altre otto case, o che hanno redditi superiori agli 80.000 euro l'anno. Allora, forse, sarebbe il caso di rimettere in piedi questo sistema, ma l'emergenza abitativa non è un problema per questa finta sinistra e ovviamente non è mai stato un problema per quelli che si dichiarano di destra. Questa è la rivoluzione sociale che vogliamo fare. Vogliamo rimettere al centro questi temi. temi. Abbiamo poi avanzato proposte riguardo alla sicurezza stradale: il tema della scarsa manutenzione delle infrastrutture è sotto gli occhi di tutti. Tutti infatti sappiamo qual è il problema. E allora, forse, dobbiamo pensare a ripartire dai problemi dei cittadini, da quello che vivono tutti i giorni. È forse il caso di varare un piano straordinario per rimettere in funzione le strade, ma non quelle che passeranno all'ANAS dopo lo sconquasso delle Province, quando l'ANAS si troverà a gestire quell'incredibile buco delle strade provinciali mai perché il ministro Delrio ha detto di aver cancellato le Province ma di fatto le ha solo distrutte: noi pensiamo che dobbiamo ripartire dalle strade delle Città metropolitane. Dobbiamo dare servizi ai cittadini. Anche questo non è stato preso in considerazione. L'ultima proposta che avevamo presentato riguardava i paradisi fiscali,

che hanno una capitalizzazione che varia tra i 500 e gli 890 miliardi di dollari e la sede, ad eccezione di Microsoft, nel paradiso fiscale del Delaware, possano continuare questo sistema. Per non parlare delle società cinesi, che hanno tutte quante la sede nei paradisi fiscali delle Cayman. E noi non affrontiamo questi temi. Chi è allora che che deve pagare le tasse? Sempre i poveri cristi, i cittadini che cercano di galleggiare in questo mare? O forse sarebbe il caso che facciamo pagare le tasse a chi ha potenza economica e finanziaria e non le paga? Forse sarebbe il caso di rimettere al centro questi temi. vede però che non si vuole fare, perché è più importante difendere gli interessi di quei pochi potenti piuttosto che gli interessi diffusi e collettivi. Forse questo dovremmo fare.

Come se la chiesa di Aulla avesse più dignità di qualsiasi altra chiesa d'Italia. Stranamente, però, il senatore Barani è di Aulla; forse il santo protettore di quella chiesa è il Bettino Craxi di cui lui ha messo la statua in piazza. Forse è quella roba lì. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Per non parlare di altri monasteri, sempre di Aulla. Per non parlare del fatto che diamo un contributo un contributo di viaggio ai consiglieri di Stato che, poverini, devono risiedere nella Provincia di Bolzano. Come se i consiglieri di Stato non si potessero pagare un viaggio in treno. Non riesco allora a capire la *ratio* di tutto questo. La *ratio* di tutto questo è di aver visto dei senatori che hanno fatto i comunicati stampa riportati localmente dicendo: «È stato approvato approvato un mio emendamento», «Oh, che bellezza, oh, che cosa importante, oh, quale contributo diamo alla società, al popolo e ai cittadini, perché il mio emendamento è importante».

gli interessi di chi ha il potere in Italia (gli interessi economici e finanziari che dominano la politica) rimetta al centro l'interesse collettivo e diffuso piuttosto che gli interessi particolari. Questo lo possiamo fare solo noi, perché voi non lo avete fatto come non lo hanno fatto gli altri e non siete assolutamente assolutamente in grado di farlo. C'è una sola speranza per questo Paese: che se ne vanno tutti a casa e che il Governo lo facciamo noi. Signor Presidente, lo hanno già detto in molti: siamo all'ultimo atto della rappresentazione della società, del lavoro, dell'economia e del Paese che i Governi del PD hanno allestito per tutto il corso di questa legislatura. Così, anche oggi ci troviamo a commentare, purtroppo, misure asfittiche, senza respiro, che non porteranno ad alcun risultato in termini di risposte serie alle concrete aspettative economiche e sociali che da molto tempo ristagnano nel Paese. Eccoci dunque all'ultima manovra, alla vigilia della campagna elettorale, una campagna tutta piegata, insieme alla sua legge di bilancio, a raccogliere consenso tra molte microcategorie per andare a nutrire il bacino elettorale dell'attuale maggioranza, o almeno questo è il tentativo. Ce la ricordiamo tutti, in quest'Aula, la legge di bilancio dell'anno scorso, che doveva essere uno dei motori verso il sì al *referendum* e tutti ci ricordiamo poi com'è andata a finire. Nonostante questa impostazione tutta criticabile, l'intera opposizione ha mantenuto un atteggiamento responsabile e costruttivo. Alcune delle proposte discusse, infatti, seppur timide, abbiamo valutato andassero nella direzione giusta e le abbiamo sostenute. Lo abbiamo fatto alla presentazione del testo sulla previdenza dei lavori usuranti, cioè dei lavoratori usurati, votando favorevolmente ancorché preoccupati da un testo che rischia,

anche non continuativamente, un lavoro usurante, come quello ad esempio delle maestre di asilo o di altre categorie, possa essere considerato alla stregua di chi invece quel lavoro usurante lo ha fatto davvero tutta la vita. Lo abbiamo fatto sul *bonus* bebè e ci resta però il rammarico, come per gli 80 euro di Renzi, che al massimo serviranno a pagare tasse e tributi, che le famiglie vedono crescere ogni anno di più da quando ci siete voi. Basta un dato:

e rimarrà al 42,9. È più di un punto di pressione fiscale in più a valere sulle famiglie. E, allora, gli 80 euro di Renzi, le sue sperequazioni e le sue ingiustizie, e gli 80 euro di questo*bonus* bebè bebè non basteranno nemmeno a pagare l'aumento di tassazione sulle famiglie che in questi anni si è alimentato.

tolgono dal loro bilancio e dalle loro tasche per versarli allo Stato italiano e sappiamo tutti - lo sanno soprattutto i cittadini italiani - cosa lo Stato

Certo, è ridicola la cifra stanziata, per stessa ammissione del Governo: 25 milioni di euro per tre anni a fronte di centinaia di milioni di euro rubati ai risparmiatori dalle banche prima del loro fallimento. Se a questo aggiungiamo i tempi giudiziari che, come noto, sono lunghi o lunghissimi, il quadro negativo per quei poveri risparmiatori è completo. In compenso però e questo a noi stava molto a cuore - il principio del diritto al rimborso, come da noi richiesto nelle Aule parlamentari grazie alla mozione del collega Augello, sottoscritta da tutti i Capigruppo di quest'Assemblea, ha costretto proprio tutti, Governo compreso, a intervenire in questa legge di bilancio e non in un altro futuribile decreto-legge.

Serviva stanziare di più e sono certa che questa fosse l'opinione di tutti i colleghi, anche perché, ad occhio, questa somma divisa per gli aventi diritto si riduce ad essere di soli sette euro ciascuno. euro a ciascun cittadino che sopporta quel grande, grandissimo, a volte infernale disagio. E invece che caricare su questo fondo tutte le risorse possibili, sacrificando esigenze di qualsiasi altra natura, avete scelto di accontentare altre platee. Certo, non abbiamo potuto votare a favore, esprimendo nettamente la nostra contrarietà, a quel minestrone di norme, alcune delle quali, citandovele come le avete scritte voi, segnalano la vostra totale confusione politica. Certo che non abbiamo apprezzato che in ben due norme lo Stato stesso, dopo aver approvato una riforma del codice degli appalti, sbandierata come chissà quale conquista e che oggi, a distanza di pochi mesi, tutti tutti oramai indicano come sbagliatissima e paralizzante dell'operatività delle imprese, quando però deve realizzare interventi speciali, cioè quando si deve comportare da impresa, come in occasione delle Universiadi a Salerno o dei campionati di sci a Cortina previsti in questa legge di bilancio, deroghi da quello stesso codice che lui ha voluto, disconoscendone la sbandierata funzionalità. Come dire: le imprese devono sobbarcarsi il sempre più pesante carico burocratico per partecipare alle gare pubbliche, ma lo Stato no. Lo Stato si scrolla di dosso questo onere con un semplice emendamento, che consente ad un commissario di derogare e non rispettare quel codice. Avete fatto di tutto contro le imprese. Avete persino bocciato quegli emendamenti che a me sembrava facilissimo approvare e che provavano ad estendere ai professionisti (un'altra parte importante della nostra economia al fianco delle imprese) le norme sul superammortamento o sulla possibilità di accedere alla nuova Sabatini, cioè un aiuto a quel sistema delle professioni per migliorare il proprio reddito e la propria competitività. Oppure, emendamenti che avrebbero dato un po' di sollievo, come la famosa cedolare secca, di cui hanno parlato tutti i giornali, alle imprese commerciali. Una misura, questa, dal costo contenuto, poco più di cento milioni, che invece voi avete preferito spendere in microinterventi a pioggia, una pioggia che cadrà copiosa su manifestazioni su manifestazioni carnevalesche per sei milioni di euro nel prossimo triennio o sull'ippodromo di Merano, dove avete puntato circa tre milioni e mezzo di euro:

al mondo produttivo, alle imprese, che si spera possano trarre vantaggi reali da quel programma 4.0 che andate sbandierando ma che è ancora lontanissimo dal realizzarsi. In questa legge di bilancio non c'è alcun ravvedimento, tanto meno operoso, sulle politiche di immigrazione ed accoglienza, quelle volute da voi finora. Anzi, aggiungete risorse per alimentare l'ingresso di immigrati, seppur universitari, spendendo cinque milioni di euro nel prossimo triennio per accordi con i Paesi dell'Organizzazione di cooperazione islamica. Forse hanno ragione i nostri ragazzi, che se ne vanno all'estero per studiare e lavorare meglio, perché tanto sanno che questo non è più un Paese a loro misura. È un Paese che perde i propri giovani e che non può che impoverirsi, ma per la filosofia del vostro Governo, ci si consola tutti ospitando altri poveri e dividendo la povertà con la povertà.

realizzato una *moral suasion* (e non voglio dire di più) per molti mesi su Cassa depositi e prestiti, il Governo pensa di aggirare l'ostacolo dei vincoli che la nostra partecipazione al sistema finanziario europeo e internazionale ci impone per la salvaguardia del sistema finanziario. Vale un po' come la regola del codice degli appalti: gli altri la devono applicare, invece quando è lo Stato a doverlo fare, può anche non applicarla. Come molti sanno, mi riferisco all'aggiramento dell'ostacolo che ha sempre impedito alla Cassa depositi e prestiti di fornire la propria garanzia agli investimenti in Iran, affidando ad Invitalia lo spericolato compito di utilizzare risorse pubbliche, con una dotazione iniziale di ben 120 milioni di euro, più o meno come la cedolare secca, per fornire al sistema finanziario iraniano la garanzia dello Stato italiano. A poco sono valse le nostre richieste di ritirare quel testo e le nostre critiche, ricordando a tutti, durante i nostri lavori in Commissione, che, secondo l'Indice di Basilea, la Repubblica islamica dell'Iran è il primo Paese al mondo per rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo, addirittura prima dell'Afghanistan. In quel Paese la corruzione del sistema bancario si salda con il ruolo delle guardie rivoluzionarie, i famosi *pasdaran*, che conosciamo da tanti anni, presenti nel sistema bancario e finanziario di quel Paese. E non è finita, signor Presidente: il dato più drammatico, che tutti conoscono e che il nostro Governo fa finta di non conoscere, è che la Repubblica islamica dell'Iran ha tra le proprie missioni la distruzione dello Stato di Israele, come dimostra il grande orologio che campeggia nel centro di Teheran e che segna il tempo che manca alla distruzione di Israele, entro il 2040, cioè tra circa 8.000 giorni, quando si avvererà la profezia di Khomeini. Si tratta di 120 milioni di euro per finanziare l'ambiguità di una politica estera che ha indebolito il nostro Paese nel contesto atlantico e occidentale. Non voglio nemmeno aprire, in questa sede, il capitolo dei diritti delle donne in quel Paese e di qualsiasi altra minoranza, perché è al nostro Paese che dobbiamo pensare. se pagherete il vostro cinismo nelle urne, quando, all'indomani del voto degli italiani, sarete gli unici veri responsabili di derive estremiste o, peggio, della massiccia astensione degli italiani dal voto. Questi sono solo alcuni dei motivi che ci spingono, come Gruppo Federazione della Libertà, ad esprimere un netto voto contrario a questa inutile legge di bilancio.

questo è l'atto finale della legislatura, che ritengo corrisponda anche al vero atto finale del Governo Renzi. Non parlo del Governo Gentiloni Silveri, perché sappiamo da tempo che esso è un paravento della continuità rispetto alla politica del Governo Renzi e lo è anche fisicamente, nelle persone. Abbiamo visto infatti la pseudosostituzione di qualche ruolo interno, ma la Boschi e gli altri Ministri sono per lo più rimasti e sostanzialmente l'impalcatura è sempre la stessa. Alla fine di un percorso bisogna porsi due domande: cosa è stato fatto e cosa viene lasciato in eredità a chi seguirà. Sul cosa è stato fatto, signor Presidente, per essere molto sintetico userei una terminologia straniera, che però in questi giorni va molto di moda: *fake news*. essenzialmente uno sbandieramento di notizie fasulle o quantomeno totalmente incongruenti rispetto alla realtà che vive il Paese, Paese, cercando di creare un'illusione di ripresa economica, di disoccupazione sparita, di situazioni risolte, di capacità del nostro Paese di essere convincente a livello europeo.

della scelta fatta da altri, per convenienza di altri, delle sanzioni alla Russia e siamo ancora qua, purtroppo spettatori delle scelte che fanno altri Paesi nello scacchiere mediorientale e sulla sponda Sud del Mediterraneo, con buona pace del ministro Minniti, che nelle scorse settimane e negli scorsi mesi andava prendendosi il merito di soluzioni che, evidentemente, come vediamo oggi, avevano la durata e la forza di resistenza di una carta velina. Che cosa lascia, quindi, il Governo? Quali sono le eredità? Possono esservi anche progetti iniziati e non conclusi. La bontà di un'amministrazione non sta solo nel fare delle opere, ma anche nel progettare opere che chi verrà dopo continuerà e, francamente, di progetti sul campo di cui poter di cui poter essere soddisfatti e contenti o su cui poter riporre fiducia non ne vediamo. Anzi, vediamo che in queste ore e in questi giorni l'accanimento del Governo e di parte della sinistra, essenzialmente la sinistra PD di Renzi che sta riabbracciando una parte della sinistra massimalista bersanianiana, posizionarsi e riposizionarsi per lo *ius soli*. Questo è il progetto che lascia in eredità il Governo Renzi-Gentiloni Silveri al Governo futuro. Complimenti, non c'è che dire. Gli italiani non ne sentono certamente il bisogno, ma per voi questa è la soluzione di tutti i problemi, perché altri problemi, in Italia, non esistono: non c'è la disoccupazione, la ripresa economica è forte, le imprese sono solide, la buona scuola ha prodotto ottimi frutti, gli studenti vanno con facilità a scuola, anche senza che i genitori li accompagnino. Insomma, Presidente, purtroppo questa è la legge di bilancio che certifica il fallimento di un Governo al quale, non noi di sicuro, una parte degli italiani aveva dato fiducia. Questa fiducia è stata tradita, a partire dalle riforme o pseudoriforme che il Governo Renzi, all'inizio del proprio mandato, aveva dichiarato come fondamentali, salvo impegnare poi, sui mille e rotti giorni del proprio mandato, cinquecento giorni per una riforma costituzionale che ha portato a sfasciarsi quella impalcatura di fondo. Una riforma costituzionale che, a sua volta, è il paradigma del modo di pensare di Renzi: l'importante è che tutto risponda a lui, l'importante era costruire un sistema nel quale l'annuncio

quando i cittadini vanno a votare, non votano sul quesito di un *referendum*, ma sulla persona che l'ha proposto e di questo abbiamo avuto abbondante riprova.

una microcertezza per le famiglie che era il *bonus* bebè e ce lo ritroviamo in bilancio dimezzato, non più 80 euro, ma 40 euro e per di più semplicemente per un anno a seguire. Questo proprio nel momento in cui l'ISTAT pubblica i dati che attestano tutta la difficoltà delle famiglie a svolgere il proprio compito e a dare una nuova generazione al Paese; un Paese che perde addirittura le nascite e registra un decremento demografico; un Paese nel quale i giovani - l'anno scorso più di 100.000 - sono stati costretti a emigrare all'estero per trovare un lavoro; un Paese che invece fa venire nelle proprie città, distribuendole tramite i prefetti, forze che a questo punto definisco di occupazione, o meglio, di sostituzione etnica: gli stranieri clandestini.

La risposta che è arrivata ha raggelato il collega senatore del Partito Democratico, perché l'ambasciatore ha dichiarato placidamente: guardate i vostri numeri,

non corrisponde non solo al *sentiment*, a quello che la gente percepisce, ma alla realtà dei fatti, perché i giovani italiani emigrano e vanno in quel Paese, dove le proposte e le capacità di fare economia sono maggiormente credibili rispetto a quello che il Governo riesce a fare in Italia. Italia. È di queste ore la notizia di una giovane mamma che è stata licenziata da Ikea: è il paradigma esattamente opposto a quanto Renzi ci ha detto negli scorsi anni. Renzi ci ha detto - e Gentiloni Silveri gli va dietro - che dobbiamo incentivare gli investimenti esteri in Italia perché così si crea più lavoro. Noi diciamo da sempre che bisogna fare in modo che gli italiani abbiano fiducia e spendano le proprie risorse in Italia, che le famiglie che le famiglie abbiano ancora voglia di investire in Italia e che le imprese abbiano ancora voglia di fare impresa nel nostro Paese, perché quando arriva una multinazionale assolve ad un interesse finanziario.

e le tutele sociali vanno a calare. Abbiamo bisogno che riprenda fiducia quell'Italia fatta dagli artigiani, dai piccoli imprenditori, da chi con la forza del saperci fare e con la credibilità di chi, quando spende una parola, la mantiene, fa impresa e crea occupazione stabile. Signor Presidente, una delle cose di cui avremmo avuto più bisogno in questa legge di bilancio e in questi ultimi scampoli di legislatura è la riacquisizione di credibilità da parte di chi fa politica.

dà l'idea di una politica che, avvicinandosi la scadenza elettorale, altro non vuol fare che strizzatine d'occhio clientelari e, santo Dio, c'è bisogno di tutto, tranne che di questo.

Noi, al contrario, abbiamo intenzione di andare al Governo per cancellare gli errori fatti dal Governo Renzi, ma, soprattutto, per fare concretamente quelle scelte di svolta che occorrono in un Paese impantanato. Dov'è finita la riforma del sistema giudiziario, Dov'è finita la riforma del sistema giudiziario, così da avere certezza della pena e condanne per chi ha truffato i cittadini con le banche, Presidente?

pochi spiccioli, 50 milioni di euro, che significano poche centinaia di euro divisi per i danneggiati dalle truffe delle banche, che si potranno avere solamente

e ne è sorto, diciamolo, un grande casino. Qui dentro ci avete messo tutto ed è diventato sostanzialmente quello che una volta veniva chiamato un *omnibus*, a cui si è attaccato, volta per volta, un vagone e non si capisce neanche più da che parte andrà questo treno, salvo deragliare.

incapacità da parte della sinistra di Governo di essere critica nei confronti di qualcosa che non fa l'interesse dei cittadini, ma solamente quello delle *lobby*, continuiamo a fare i primi della classe. Continuate a far fare agli italiani i primi della classe applicando su se stessi regole che gli altri Paesi disapplicano, con il risultato che tutti noi paghiamo un prezzo doppio. Noi facciamo i primi della classe in una classe di somari *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)* o addirittura in una classe che si avvantaggia del nostro essere i primi della classe, che però ne pagano poi il prezzo. che Renzi dica che quando è arrivato aveva una quantità naturale di infrazioni delle leggi comunitarie che poi ha risolto. Signora Presidente, se la risoluzione delle infrazioni delle leggi comunitarie significa costringere i nostri commercianti, i nostri imprenditori, il nostro Paese a inginocchiarsi davanti alle banche tedesche o alla finanza di un Paese come il Lussemburgo, che ha una tassazione ancora una volta differenziata rispetto a quella italiana, ciò significa non capire che l'Europa o è un'Europa dei popoli oppure non ha motivo di esistere.

all'immagine di un Paese che è in ripresa mentre non lo è, pensando di illudere che i problemi siano risolti come avete fatto con le zone terremotate, mandando le telecamere a riprendere un taglio di nastro, ma dimenticando che nel 90 per cento di quelle zone ancora oggi si aspetta che siano semplicemente spostate le macerie. Quella macerie. Quella gente, con dignità, chiede di ricominciare ed è la stessa dignità che c'è in tutto il Paese, dove le nostre imprese chiedono di ripartire. Meno burocrazia e lasciateci lavorare: questa è la sintesi estrema che si sente nelle zone terremotate e in qualsiasi angolo del Paese, che si sente dire da qualsiasi commerciante di quelle zone e da qualsiasi imprenditore di questo Paese. Ripeto, meno burocrazia e lasciateci lavorare. Prima vi toglierete dalle scatole e prima daremo noi agli italiani un'alternativa seria di Governo, in grado di essere rispettata anche in Europa. *(Applausi dal

del senatore Candiani mi fa venire in mente un modo di dire delle mie parti, la terra di Lunigiana: a volte chi pensa di andarle a dare, le prende. Quindi, cosa succederà dopo le elezioni sarà il popolo sovrano a deciderlo. A parte questo, onorevoli colleghi, a molti di noi in questi giorni saranno fischiate le orecchie. La grande stampa italiana scandalistica ha guardato ai nostri lavori, rispolverando tutto l'armamentario dal dileggio all'indignazione per quel faticoso lavoro di tessitura che stavamo facendo in Commissione da quindici giorni,

per capire che la gestione del ciclo elettorale rappresenta da sempre, nella storia delle democrazie occidentali, uno dei momenti più difficili da affrontare. Si tratta di una caratteristica che non è solo italiana, ma riguarda la maggior parte di quei Paesi che si affidano a libere elezioni. un sistema tutt'altro che perfetto, ma, come ricordava Winston Churchill, la democrazia è la peggior forma di governo, eccezion fatta per tutte quelle forme che si sono sperimentate fino ad ora. Diceva questo dopo il fascismo, il comunismo, il nazismo e il populismo. Di ciò dobbiamo essere consapevoli se vogliamo avere certezza dei nostri sforzi e giungere a una valutazione serena del nostro lavoro. Infatti, la democrazia si fa non nelle urne

e che questo risultato non era scontato. La stessa Commissione europea ne ha dovuto prendere atto, pur sollecitando il Governo che verrà a una maggiore prudenza finanziaria, alla quale - ne siamo sicuri come Gruppo - saremo in grado di rispondere con la forza di quei numeri che non coincidono con i desiderata della Commissione, fin troppo chiusa in una prospettiva che definirei autarchica. Basti pensare alle misure non convenzionali assunte dal governatore Draghi o alla discussione attualmente in atto presso il Congresso americano sulla riforma fiscale voluta da Trump. Si tratta di un Paese che, a differenza dell'eurozona, ha deciso di puntare tutto sullo sviluppo, anche a condizione di determinare un *deficit* di finanza pubblica pari a quatto volte quello europeo e a un forte *deficit* della bilancia dei pagamenti:

il confronto può essere ancora più illuminante. Scendiamo solo al Governo Amato, che è un autorevole membro della Corte costituzionale, il quale, nel lontano 2001,

Rispetto all'anno precedente, il maggior disavanzo fu quasi di 30 miliardi di euro. Fece indubbiamente meglio il ministro Tremonti. Nel 2007 vi fu un drastico contenimento del *deficit*, dovuto essenzialmente alle maggiori entrate straordinarie a seguito del condono; sì, quel condono condono che è servito molto all'Italia e agli italiani per la ripresa. Quelle misure favorirono indubbiamente gli evasori, ma costrinsero gli stessi all'emersione: li hanno tirati fuori.

Le politiche deflazionistiche indotte dal Governo Monti portarono a un leggero contenimento del *deficit*, circa 4 miliardi di euro, ma gli effetti di quella politica furono devastanti. L'Italia si mosse in controtendenza rispetto agli altri Paesi dell'eurozona, alimentando quella crisi di cui solo oggi, a distanza di cinque anni, si intravede la fine. Tutto grazie a quella legge di deve essere letta. Il paragone con gli anni passati ci permette, quindi, di guardare al nostro lavoro con maggiore serenità. Abbiamo fatto il possibile, tenendo conto del ciclo elettorale, tanto più se consideriamo gli anni di una legislatura che dire travagliata è forse un eufemismo. Le passate elezioni avevano consegnato all'Italia un Paese largamente ingovernabile, caratterizzato da profonde fratture sociali, dovute soprattutto soprattutto agli errori dei precedenti Governi; fratture che avevano determinato l'entrata in Parlamento di forze populiste che avevano profondamente alterato il precedente equilibrio bipolare. Ne era derivata una situazione di completa ingovernabilità, nonostante il ricorso a formule di ingegneria costituzionale, che non avevano, tuttavia, una base programmatica comune. Da qui gli affanni di una maggioranza sempre in bilico, in cui convivevano opposte pulsioni, pronte a esplodere nella voglia catartica di una resa dei conti. Basti pensare alle forzature - il voto a scrutinio palese - che portarono alla decadenza di Silvio Berlusconi, trattato come Craxi: protagonisti della vita politica italiana che si sono voluti eliminare per via giudiziaria, con un vero e proprio colpo di Stato. Per quanto ci riguarda, il mio Gruppo ha sempre cercato di garantire quel minimo di governabilità nell'interesse del Paese (diceva il nostro *leader*, Denis Verdini, che eravamo 14 Ministri senza portafoglio), al fine di evitare il ricorso alle elezioni anticipate (sì, le abbiamo impedite), che avrebbero premiato proprio le forze antisistema e riprodotto in Italia la sindrome spagnola, che nel 1920 aveva già fatto un mucchio di guai, mortali. Era un pericolo che un Paese con il più alto debito europeo non poteva permettersi. Abbiamo fatto il nostro dovere, senza chiedere alcunché in cambio, sopportando stoicamente gli insulti di tanta parte della stampa benpensante, ma aliena dal considerare la drammaticità della situazione italiana; sopportando anche gli insulti che ci sono stati fatti in Commissione e che ci sono stati rivolti in questa sede. Sì, abbiamo permesso di dare soldi anche a delle chiese alluvionate: ne siamo fieri e orgogliosi, perché vogliamo andarci a pregare in quelle chiese; non vogliamo solo andare a guadagnare e a fare i pagliacci

Quando l'ideologia diventa falsa coscienza, non esiste speranza alcuna per un'operazione di verità. Ci vorrà del tempo, ma alla fine meriti e demeriti saranno riconosciuti.

di legge n. 2960** Signor Presidente e onorevoli colleghi!! Per prima cosa voglio mandare un abbraccio solidale, un messaggio d'incoraggiamento alle operaie e alle sarte della CANALI di Sovico, dalle mie parti in Monza-Brianza. Alla Canali quelle lavoratrici stanno conducendo una dura battaglia contro un padronato sordo e gretto che le vuole mettere per strada, pur essendo la Canali un'azienda florida. Analogamente il mio pensiero va ai lavoratori in sciopero della Amazon: Matteo Renzi e il PD stanno con il *managment* dell'Amazon, tanto che il numero 2 di quel colosso lo mettono al Governo. Noi stiamo accanto a chi lavora, senza se e senza ma. E quindi il nostro cuore e le nostre menti sono con i lavoratori dell'Amazon, della Whirpool, della SDA-Express e della Alpitour e di tutte le realtà aziendali che scaricano sui lavoratori scelte manageriali che non hanno a che fare con l'andamento dei ricavi o con la congiuntura. La manovra di bilancio - che rappresenta il principale atto politico per decidere le scelte economiche del Paese - avrebbe dovuto partire da quelle realtà. Partire dalla realtà del Paese, dai suoi drammi e dalle sue speranze. E da questo approccio che si misura il coraggio e la qualità di una classe dirigente. Non dimentichiamo mai che alle disposizioni contenute in una legge come quella di bilancio guardano con preoccupazione e speranza lavoratori, cittadini, giovani e meno abbienti. Il loro futuro per tanta parte dipende dalle nostre scelte. Non dimentichiamolo mai! invece ci troviamo davanti a un provvedimento imposto dalla maggioranza di centrodestra PD-Verdini-Alfano che ci fa fare passi indietro e nelle direzioni più disparate. C'è un velo di propaganda che copre una pletora di interventi di scarso impatto, di localismi e particolarismi nascosti tra le pieghe degli emendamenti. Si tratta in verità di un *collage* vuoto di impegni concreti, con l'unico obiettivo di foraggiare il consenso intorno al progetto di Renzi ovvero al codazzo di liste civetta attorno al suo PdR! Per consolidare il sostegno di ALA sono state approvate proposte *spot*, e stava per rientrare anche il condono. C'è un parziale rifinanziamento del *bonus* bebè, altrimenti un altro pezzo di maggioranza ritorna nella destra; e poi 60 milioni invece dei 600 che sarebbero necessari per il superamento del superticket, per provare a dare una spruzzatina di colore rosso pur sapendo che si tratta di una fregatura! Sono stati presentati e approvati emendamenti della maggioranza scandalosi come la modifica al codice antimafia, che esonera dal presentare la certificazione antimafia le società agricole che ricevono i finanziamenti europei fino a 25.000 euro, nonostante sia risaputo che le mafie hanno forti interessi e fra gli altri sono destinatarie anche di questo tipo di fondi. Ma sono state esentate dal pagamento dell'IMU anche le imprese di rigassificazione ricorrendo ad una sconcertante interpretazione autentica di una norma della finanziaria del 2016. Di conseguenza, è stata tolta la possibilità ai comuni, dove sono stati installati quegli impianti, di introitare milioni di euro a tutto vantaggio di grandi società italiane ed internazionali. Il fatto, oltre ad essere sconcertante in sé, è in palese contraddizione con quanto sostenuto dalla stessa Guardia di finanza, secondo la quale queste società dovrebbero essere tenute a pagare l'IMU. C'è anche poi un'inspiegabile deroga al codice degli appalti. Che riguarda segnatamente i campionati mondiali e la coppa del mondo di sci a Cortina d'Ampezzo, come anche le Universiadi del 2019 a Napoli. Tutto avverrà senza indire gare pubbliche, in sprezzo del fatto che ciò produrrà inevitabilmente un contenzioso, data la palese violazione di ogni canone di trasparenza e di lotta alla corruzione. Si istituisce poi anche un Parco interregionale sul Delta del Po. Il tutto senza aver coinvolto i territori, le associazioni e le popolazioni residenti. Sono ben 21 le società ambientaliste riconosciute che hanno espresso la loro contrarietà, ma siete andati avanti senza ascoltare nessuno. Ci sono poi milioni e milioni di euro di "marchette" a vari enti e fondazioni. Finanziamenti dati a pioggia, prebende necessarie ai vari senatori per la futura campagna elettorale: 400.000 euro per tre anni per un'anonima chiesa ad Aulla; altri 100.000 per il 2018 e 400.000 nel 2019 per un'altra abbazia sempre ad Aulla; 400.000 a una fondazione di Trieste, soldi peraltro sottratti al fondo per la ricerca; 1 milione di euro nel 2019 e 2020 all'università di Padova e alla Federico II di Napoli, emendamento equamente condiviso e sottoscritto da senatori veneti e campani. Per non dire degli oltre 3 milioni di euro per l'ippodromo di Merano e via cantando. Così si pensa di conquistare consenso nel mercato elettorale, mentre la credibilità di questa classe dirigente crolla! Non ci si lamenti poi del populismo e dell'antipolitica, perché la via maestra è quella che voi avete tracciato! Il testo che oggi arriva all'esame dell'Aula è infatti insoddisfacente, non risponde alla necessità di determinare una svolta nell'economia e non fa le scelte radicali di cui si avverte da tempo la necessità. Manca cioè qualsiasi disegno progettuale per l'Italia dei prossimi anni. Manca una strategia, un progetto, una visione della società italiana! Non si adottano misure strutturali di carattere universale, che diano sostegno, in primo luogo, alle parti più povere del Paese. Al contrario! Questa manovra è ispirata unicamente a finalità contingenti e puramente elettoralistiche! Il nostro punto di vista è esattamente opposto! Bisogna partire da una fotografia delle condizioni economiche e sociali dell'Italia reale. Solo su questa base poi fare le scelte, decidere le priorità, valutare l'effettivo impatto delle misure inserite nella legge di bilancio! A dieci anni dall'inizio della crisi, il PIL italiano è ancora sotto al livello del 2007 di circa 8 punti. La perdita cumulata è di circa 800 miliardi di euro. Tutti i principali dati macroeconomici ci parlano di un profondo impoverimento del Paese, di una pesante difficoltà di numerosi nuclei familiari, anche nelle aree storicamente meno fragili da un punto di vista sociale. E noi tutti sappiamo che sarà drammaticamente difficile recuperare nei prossimi anni il crollo dell'occupazione patito dal Paese in questi anni. I problemi investono sia il lato della domanda (consumi inferiori del 5 per cento, investimenti di quasi il 30 per cento), sia il lato dell'offerta con una perdita ulteriore di produttività del lavoro. Negli ultimi anni, sia da parte del Governo Renzi che di quello Gentiloni, c'è stata una rigida insistenza nel perseguire una politica dell'offerta basata sulla contestuale riduzione della spesa e delle imposte come via per recuperare la crescita. Così l'Italia ha incredibilmente sprecato anche i margini di flessibilità ottenuti in sede europea. Gli interventi di decontribuzione fiscale, presenti soprattutto nel *jobs act*, non hanno consentito di recuperare i posti di lavoro persi, come dimostrato anche dalla grande diffusione dei contratti a tempo determinato. Una tendenza confermata peraltro, nel corso delle nostre audizioni, anche dai rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio. A questo Paese, che continua a soffrire dopo anni di crisi, servono risposte concrete e coraggiose: non si può continuare con i tagli e le sofferenze sociali! Articolo 1 ha presentato perciò una serie di proposte precise, alcune fra le più qualificanti costruite insieme ai colleghi di Sinistra Italiana. Tutte quante hanno il segno dell'equità sociale. E solo per questo avrebbero meritato un esame più rigoroso e puntuale! Ad esempio abbiamo immaginato un diverso utilizzo delle risorse del Fondo per gli investimenti di cui all'articolo 95, centrato su un'azione sinergica costruita su più interventi: risanamento e manutenzione del territorio; rischio sismico; miglioramento delle periferie urbane, bonifica dei territori, recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale e o produttivo. E ancora: investimenti nel campo dell'efficienza energetica degli immobili della pubblica amministrazione, potenziamento del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile, soprattutto per il pendolarismo regionale e il trasporto su ferro. Infine investimenti per la costruzione di asili nido o per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Ma poi c'è il tema per noi decisivo della promozione e della dignità del lavoro. È un carattere decisivo della nostra identità e della nostra azione politica. Proponiamo politiche strutturali di incentivo al lavoro e segnatamente alle assunzioni a tempo indeterminato. Le nostre proposte sono serie, sostenibili e molto articolate. Tanto per cominciare: reintrodurre la causale per potere fare ricorso ai contratti a tempo determinato. E poi: introduzione di un condizionamento per il *bonus* assunzioni, nel senso di prevedere sanzioni nel caso in cui i datori - che usufruiscano del *bonus* contributivo del 50 per cento per le assunzioni - licenzino poi i lavoratori nei tre anni successivi a quello della fruizione del beneficio dello Stato! Questi sono speculatori, non datori di lavoro! Ancora: sanzioni per l'uso improprio dei tirocini. L'ammontare della sanzione deve essere proporzionale alla gravità dell'illecito; particolarmente se viene violata la finalità formativa o se si pretende di sostituire personale in malattia, maternità o ferie. Abbiamo pensato inoltre di riconoscere la decontribuzione per le assunzioni dei giovani a tempo indeterminato solo per le assunzioni a tempo pieno. C'è poi il tema grave e ricco di implicazioni economiche e sociali della delocalizzazione delle attività aziendali che ricevono aiuti dallo Stato. Personalmente me ne sono occupata per la vicenda K-Flex, azienda italiana specializzata nella produzione di materiali elastomerici per isolamento termico ed acustico. Una azienda *leader* mondiale per qualità e innovazione tecnologica dei propri prodotti, che ha deciso improvvisamente di traslocare la produzione nello stabilimento in Polonia. Un nostro emendamento al riguardo non costava nulla. Era virtuoso, sostenibile e molto preciso: le imprese che operano sul territorio, italiane o estere, che abbiano ricevuto aiuti dallo Stato, devono restituirli in caso di delocalizzazione (anche all'interno dell'UE) delle attività nei tre anni successivi alla ricezione del contributo. L'emendamento prevedeva inoltre specifiche sanzioni per le imprese sopra i 1.000 lavoratori che non rispettino il vincolo dei livelli occupazionali e della continuità aziendale. Per questo abbiamo anche proposto la costituzione di un Fondo (finalizzato ad esempio alla concessione di incentivi fiscali) a favore delle aziende che assumano lavoratori posti in mobilità proprio dalle imprese che delocalizzano in Stati esteri, anche dell'Unione europea. Sempre in materia di lavoro abbiamo chiesto l'incremento del fondo per le vittime dell'amianto, con l'estensione della platea dei beneficiari, ma anche del fondo per il risanamento degli edifici pubblici che richiedano bonifica dall'amianto. Abbiamo inoltre proposto sanzioni più severe ed efficaci per chi ricorre in modo fittizio a rapporti di lavoro *part time* che però occultano lavoratori a tempo pieno, ma anche sanzioni incisive per combattere la piaga dell'evasione contributiva. veniamo al tema delle pensioni. Dal 1996 il regime pubblico ha visto aumentare forme di sperequazione e di esclusione sociale di cui sono stati vittime molti anziani in condizioni di fragilità e povertà; fasce di cittadini che spesso non riescono neanche ad accedere all'assegno sociale. Il nostro Gruppo ha fatto diverse proposte, tra cui anche quella in cui si prevede che i risparmi di spesa risultanti dal monitoraggio delle domande dell'APE *social* vengano utilizzati per finanziare il Fondo sociale per la formazione e l'occupazione di cui al decreto-legge Il Governo per parte sua ha proposto un intervento più articolato, introducendo misure previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori addetti

Si tratta di un intervento provvisorio, non strutturale e insoddisfacente! A nostro avviso si doveva fare molto di più. Si è infatti scelto di coinvolgere una platea inferiore al 5 per cento del totale dei lavoratori, e soprattutto mancano norme atte a garantire effettiva dignità al futuro previdenziale dei giovani. Per questo insieme di motivi Articolo 1 sostiene con convinzione la mobilitazione della CGIL indetta nelle piazze per il 2 dicembre! Ma c'è un'altra materia davvero decisiva per il nostro futuro, quella ambientale. Manca quindi del tutto, ancora una volta, una strategia complessiva in grado di coniugare le esigenze di sicurezza ambientale e contestualmente di crescita economica. Siamo intervenuti poi sul diritto allo studio, proponendo nuovi finanziamenti a livello sia regionale e statale. L'obiettivo è rafforzare il fondo di funzionamento ordinario delle università, anche al fine di garantire nuovi scatti stipendiali ai docenti universitari, oltre a misure per il personale Ata. In verità questa manovra avrebbe potuto rappresentare un'occasione per un effettivo rifinanziamento del Sistema sanitario nazionale. Questo tanto più che la nostra spesa sanitaria sul Pil è più bassa della media europea e sta ulteriormente decrescendo. Senza dire della necessità di rendere possibile l'assunzione di personale sia medico sia infermieristico con l'abolizione dei vincoli al tetto di spesa per personale. Davvero gravi sono poi le agevolazioni fiscali per società di capitali nello sport dilettantistico. In pratica si è scelto di introdurre la logica del profitto, di fatto facendo pagare - con il dimezzamento dell'IRES a loro vantaggio - la palestra dei ricchi nei centri cittadini ai disoccupati di periferia. E invece dalla parte migliore del mondo dello sport veniva la richiesta di riconoscere il valore sociale dello sport. che costerà caro a molti investitori privati. Cari colleghi, alla luce di queste considerazioni, è chiaro il senso politico delle principali battaglie del nostro Gruppo. La nostra è una impostazione radicalmente alternativa alla vostra! Attraverso numerosi emendamenti e proposte di merito, e con un lavoro molto intenso fatto in Commissione la posizione di Articolo 1 è chiara di fronte al Parlamento ed al Paese! A questa legge di bilancio diciamo no perché siamo accanto alla sofferenza sociale del Paese!! NO, perché ci opponiamo a una politica di bonus, regalie e mance elettorali! NO, perché abbiamo un'idea precisa per il futuro: l'Italia può cambiare solo, con politiche più giuste e solidali a favore del lavoro con nuove tutele e diritti, con maggiore equità nella sanità, nella scuola e nella ricerca, e con nuove politiche ecologiche! Votatela voi, questa pessima legge! **Testo

la legge di bilancio è l'atto conclusivo di questa legislatura; dalla sua struttura possiamo comprendere l'azione politica dei cinque anni trascorsi. Ripercorriamoli brevemente: la legislatura iniziò sull'onda del Governo Monti, quello che per i *media mainstream* e quindi per l'opinione pubblica «salvò l'Italia dal baratro». In realtà oggi sappiamo che quella fu una clamorosa *fake news*. Da anni la Commissione europea nel suo *report* annuale sulla sostenibilità fiscale dei Paesi dell'eurozona ci ricorda che la sostenibilità dei conti italiani è la migliore di tutti sul lungo periodo, frutto delle politiche di contenimento della spesa pubblica e di preparazione all'ingresso nell'euro che l'Italia adottò fin dagli anni Novanta. Ma allora perché il Governo ha continuato, e con il Governo Renzi ha accelerato, il contenimento della spesa pubblica? Semplice: lo impose la BCE con la famosa lettera Trichet-Draghi dell'estate 2011. Quella lettera rappresenta tuttora la guida politica dell'Italia. Lì dentro c'era scritto tutto quello che è stato avviato da Monti e realizzato in questa legislatura: l'abolizione dell'articolo 18, la precarizzazione strutturale del mercato del lavoro, la riforma del sistema pensionistico, il contenimento degli stipendi dei lavoratori, attuato mediante una disoccupazione strutturale superiore al 30 per cento, considerando i lavoratori scoraggiati, cioè coloro che hanno smesso di cercare lavoro, ma che non vengono conteggiati mai nei dati ufficiali, e quindi la privatizzazione dei servizi pubblici primari. Una terribile *spending review*. Queste politiche hanno creato 5 milioni di poveri e il fallimento di oltre 100.000 imprese. Sono numeri da guerra. Mai dalla fine della Seconda guerra mondiale l'Italia si è trovata in una situazione così drammatica. E con la legge di bilancio in discussione, il Governo di questa legislatura, traghettatrice verso un'Europa che ci fagociterà, persegue l'identica linea politica cristallizzando una presunta ripresa che non è altro che stabilizzazione del ciclo economico all'interno di una lenta ed inesorabile spirale deflazionistica. L'unica preoccupazione è quella di soddisfare le prescrizioni dell'Unione europea, volte unicamente alla distruzione della domanda interna, celata dal contenimento dei conti pubblici e, quindi, non allo sviluppo del Paese. Negli ultimi cinque anni sono successi, però, due avvenimenti, peraltro previsti e prevedibili, che renderanno vani gli sforzi governativi di stabilizzazione. Il primo è la crisi bancaria Contrariamente a quello che ci raccontano i *media* *mainstream*, le responsabilità del sostanziale fallimento di numerosi istituti di credito italiani non sono da addebitare a un inefficace controllo degli enti preposti alla vigilanza, Banca d'Italia e Consob *in primis*. Se pur le mancanze di questi organi nella vicenda sono gravi e andranno accertate le rispettive responsabilità, sappiamo che molto dipende dall'Unione bancaria europea, che ha affossato il nostro sistema creditizio.

Queste politiche, creando disoccupazione e fallimenti diffusi, hanno impedito alle banche di rientrare dei prestiti e degli impieghi accordati, destabilizzando l'intero sistema bancario. In secondo luogo, si è proceduto all'adozione del *bail in*, oltretutto anticipando le norme comunitarie, quasi a voler farsi vanto di essere

che vietano l'intervento dello Stato nella risoluzione delle crisi bancarie. Il secondo avvenimento è la reazione della società a queste politiche, incompatibili non solo con la Costituzione, ma soprattutto con il buonsenso comune. All'estero lo abbiamo visto soprattutto con la Brexit e l'elezione di Trump negli USA: il popolo e, in particolare, la classe media - il grande pollo da spennare - rifiuta le politiche anti lavoro e pro mercati. Lo vediamo proprio oggi in Germania, incapace di creare una compagine governativa che non contempli forze politiche fortemente contrarie alla cosiddetta integrazione europea. Insomma, il fallimento dell'ordoliberismo nell'Unione europea a trazione tedesca - e sotto altri aspetti, nell'intero mondo occidentale - è sotto gli occhi

prodotti creati dalle multinazionali? Ecco che diventa fondamentale invertire la rotta delle scelte economiche e produrre un'autentica politica dei redditi, unico modo per far ripartire i consumi. E questa legge di bilancio non lo fa, compromettendo il tessuto socio-economico e produttivo italiano

Signora Presidente, colleghe, colleghi, rappresentanti del Governo, la manovra finanziaria per il 2018 prende le mosse dai migliori auspici, ma rimane fortemente condizionata, nonostante i segnali di una ripresa ormai consolidata, dalla ristrettezza delle risorse disponibili. È una manovra che contiene diverse misure positive, che cercano di favorire da una parte lo sviluppo e dall'altra l'inclusione sociale, ma che purtroppo non riesce ancora a soddisfare in pieno le esigenze del nostro Paese. Sul testo presentato dal Governo è stato fatto uno scrupoloso lavoro da parte della Commissione bilancio e dal presidente Tonini, che ringrazio anche per aver accolto diversi nostri emendamenti che sono strategici e non solo per il nostro territorio. Un grazie sincero va anche al vice ministro Morando, così come a tutti i rappresentanti del Governo che si sono succeduti nei lavori in Commissione e dimostrati disponibili al confronto e a comprendere l'importanza delle nostre richieste. Registro con soddisfazione alcune misure che vanno nella direzione auspicata dagli autonomisti. Mi riferisco, in particolare, al rinnovo dell'ecobonus, con le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e di recupero edilizio e per le misure antisismiche. di interventi che avevamo sollecitato con una specifica mozione approvata da questa Assemblea. Registro con soddisfazione anche l'estensione di tutte le detrazioni energetiche ed edilizie agli IACP e agli enti assimilati, novità particolarmente importante per la Provincia di Trento e l'introduzione della detrazione per il recupero degli spazi verdi. Fra le misure positive, cito anche il rinnovo delle misure per i giovani che si occupano di agricoltura; l'istituzione dei distretti del cibo per favorire la qualità e la competitività del nostro agroalimentare, un ambito strategico per la crescita del Paese; il Piano straordinario nazionale per la realizzazione di invasi multiobiettivo e per la diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua per gli usi agricoli e civili; e civili; la sterilizzazione dell'incremento dell'aliquota IVA e delle accise per il 2018, la proroga delle cosiddette misure di superammortamento e iperammortamento, che consentono alle imprese e ai professionisti di maggiorare la quota di ammortamento dei beni strumentali a fronte di nuovi investimenti effettuati. Importanti sono anche il rifinanziamento della cosiddetta *card* cultura per i giovani; l'innalzamento da 7.500 a 10.000 euro del limite che non concorre a formare il reddito imponibile per i dirigenti sportivi e artistici che operano a titolo non professionale; gli sconti fiscali per le librerie. Per il settore della cultura noi e altri colleghi del Partito Democratico avevamo proposto alcune misure a favore del volontariato, che peraltro erano state promesse sia in Commissione che in Aula in occasione dell'approvazione della legge delega sullo spettacolo, con precisi ordini del giorno approvati. Mi riferisco alla possibilità di detrarre le spese per la formazione musicale, teatrale e coreutica, esattamente come accade per chi esercita un'attività sportiva; alla richiesta di ripristinare il 2 per mille dell'IRPEF per le associazioni culturali, inspiegabilmente cancellato per quest'anno, o alle richieste per sgravare burocraticamente il volontariato, che in molte realtà rischia di cedere sotto la pressione di adempimenti che talvolta sono insostenibili per una piccola associazione. Al Governo rinnovo la richiesta di valorizzare maggiormente la qualità culturale e il ruolo sociale del volontariato che, con passione e competenza, opera gratuitamente in ogni realtà del nostro territorio e che, se andiamo avanti così, rischiamo di scoraggiare irreversibilmente e di metterne a repentaglio la sopravvivenza, soprattutto nelle realtà più periferiche e disagiate. Per quanto riguarda gli interventi a sostegno dell'impresa, sottolineo il rifinanziamento della cosiddetta nuova Sabatini per i finanziamenti agevolati sui nuovi macchinari e il sostegno agli investimenti del Piano industria 4.0, oltre al sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo e al Piano straordinario per il *made in Italy*. Cito ancora gli sgravi contributivi e previdenziali per le nuove assunzioni a tempo indeterminato; le misure per promuovere la formazione professionale e l'apprendistato; gli interventi volti ad ampliare l'ambito di applicazione di alcuni ammortizzatori sociali; la proroga antincendi per gli alberghi approvata con il nostro emendamento; e poi l'istituzione - richiesta dalle organizzazioni operanti nel settore della disabilità e che anch'io ho sostenuto convintamente - del fondo per il cosiddetto *caregiver* familiare, finalizzato al giusto riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale ai disabili o agli invalidi. Significativo per la realtà da cui provengo è anche il sostegno ai carnevali storici e tradizionali, che da noi sono particolarmente diffusi. Prendo poi positivamente atto che, finalmente, è stata introdotta la tassazione per le imprese operanti nel settore del digitale, dando una prima risposta a esigenze emerse da tempo anche in ambito internazionale ed europeo. Positivi sono anche il fondo di ristoro ai risparmiatori danneggiati ingiustamente; il taglio parziale dei *superticket*; il *bonus* per i nuovi nati; le agevolazioni pensionistiche per i lavori gravosi. Per finire, nei giorni scorsi avevo apprezzato l'inserimento nel decreto fiscale della norma che esenta le imprese agricole che usufruiscono di fondi comunitari fino a cinquemila euro dalla presentazione del certificato antimafia. A maggior ragione, oggi esprimo orgogliosamente la mia soddisfazione per l'approvazione da parte della Commissione bilancio di un mio subemendamento, sostenuto dal Gruppo Per le Autonomie, con il quale si proroga al 1° gennaio 2019 l'obbligo del certificato per i fondi europei di importo inferiore a 25.000 euro. È un impegno che va incontro alla nostra richiesta di arrivare a un definitivo superamento del problema che - come abbiamo più volte denunciato - preoccupa fortemente le organizzazioni agricole e le stesse istituzioni, perché interessa un numero molto elevato di aziende, determinando un forte ritardo nei pagamenti. Il subemendamento approvato, però, risolve solo in parte il problema. Io spero vi sia lo spazio per rendere definitivo l'esonero per tutti o, almeno, per aumentare la soglia di esenzione. Voglio ora richiamarmi a quanto ha detto la collega Ricchiuti, invitandola ad approfondire meglio le sue parole. Io vengo da una realtà come il Trentino dove non esiste una sola situazione mafiosa, e men che meno esiste nella mia valle. Se si vogliono controllare gli atteggiamenti mafiosi delle imprese, basta chiedere agli enti pubblici di controllare direttamente tramite

anche a frequentare qualche agricoltore, per capire che cos' è un'azienda agricola. Il codice antimafia è uno dei provvedimenti importanti di questa legislatura e le azioni di contrasto e prevenzione non devono mai venire meno. Le istituzioni, però, tramite l'autorità giudiziaria, possono controllare automaticamente la posizione dei singoli richiedenti, senza costringerli a gravose perdite di tempo, che possono essere evitate. Lo stesso vale per la richiesta, contenuta nel mio ordine del giorno approvato, di esentare le particelle fondiarie delle zone montane, inferiori a 5.000 metri quadrati di superficie, dalla registrazione dei contratti di comodato, per poter ottenere i carburanti agricoli. Si tratta, solo per il Trentino, di più di 100.000 particelle e, se le aziende agricole dovessero fare un contratto di comodato registrato per ognuna, si troverebbero a dover chiudere, perché andrebbero sicuramente in perdita. Per quanto riguarda le autonomie speciali, segnalo l'approvazione di alcuni nostri emendamenti finalizzati a valorizzare esperienze virtuose messe in campo dai nostri territori e che potrebbero essere utili anche ad altre Regioni, soprattutto a quelle che aspirano a una maggiore autonomia. Mi riferisco, ad esempio, al riconoscimento della piena operatività locale dei fondi complementari e integrati regionali. Si tratta di un risultato per noi particolarmente importante, atteso da anni e fortemente sollecitato dalle istituzioni e dalle organizzazioni sindacali e datoriali. L'emendamento introduce significative e fondamentali novità anche per i fondi integrativi sanitari territoriali, prevedendo la possibilità per i lavoratori di aderire, tramite accordi territoriali o aziendali, a fondi sanitari diversi da quelli nazionali. I fondi, peraltro, funzionano anche da volano per lo sviluppo economico e sociale, attraverso il versamento dell'imposta sostitutiva e gli investimenti effettuati a favore del territorio. Sulla stessa linea si trova l'emendamento che riconosce ai nostri territori la competenza sulle concessioni idroelettriche. Si tratta di un ulteriore passo in avanti per proporre politiche innovative in ambito energetico e quindi, indirettamente, nel contesto economico e ambientale. La norma, introdotta in Commissione, rafforza il ruolo degli enti locali anche in termini di ricaduta delle risorse finanziane derivanti dalle concessioni. Infine, accanto alle novità positive introdotte nella manovra di bilancio, devo sottolineare come altre richieste avanzate dalle categorie produttive per semplificare l'enorme peso della burocrazia e ridurre l'eccessiva pressione fiscale, così come le sollecitazioni delle realtà sindacali e sociali, che chiedevano una più incisiva revisione del sistema pensionistico, non si siano nemmeno potute prendere in considerazione o non abbiano potuto trovare accoglimento, per carenza di risorse. La direzione presa dal Governo e dalla 5a Commissione è però quella giusta e mi auguro che le prossime manovre di bilancio, che saranno adottate in un contesto spero finanziariamente più favorevole, possano affrontare anche altri problemi cruciali per il Paese che in questa sede non si sono potuti considerare.

alcune delle impressioni che ho ricavato frequentando, insieme a tantissimi miei colleghi, la Commissione bilancio nelle lunghe maratone che ci hanno visti impegnati nei giorni scorsi, fino a stamattina presto, quando i lavori si sono conclusi.

Ho visto mettere tante toppe, qua e là, a problemi anche giusti; toppe corrette - per carità - alle quali è difficile opporsi,

alla ricerca di una vera e propria missione, e non per se stessi, ma per il Paese intero. Questa è la ricerca: non una missione per se stessi, ma un servizio al Paese e alla comunità intera.

opporre all'obiettivo di ricavare qualche spicciolo in più per i ricercatori? Questa è l'attività a cui ho assistito con i miei occhi, ben lontana da quella che deve essere una programmazione per obiettivi; ben lontana

Partiamo quindi dai numeri: ci sono nelle università italiane in questo momento 13.350 assegnisti di ricerca. Ricordo che l'assegno di ricerca è un contratto assolutamente debole, con bassissime tutele lavorative e senza alcuno sbocco professionale

A fronte di questo esercito di precari senza alcun futuro, abbiamo appena 2.295 ricercatori di tipo "B", la cosiddetta *tenure track*, quelli che effettivamente hanno una possibilità, una volta ottenuta

senza nome e senza volto, la durata di una forma contrattuale che - badate bene - noi stessi crediamo debba essere abolita dal panorama delle figure pre-ruolo. Si trattava di un emendamento costruito in modo tale che soltanto gli assegni che andavano in scadenza dei sei anni - e solo quelli - potessero essere rinnovati temporaneamente fino

81 della Costituzione. Forse bisognerebbe spiegare al vice ministro Morando, che rappresenta il Governo, e quindi al Governo tutto, che gli assegni di ricerca non gravano sui fondi ordinari: non c'è bisogno di alcuna copertura, perché gli assegni di ricerca gravano su fondi a progetto che gli stessi ricercatori si vanno a trovare su base competitiva.

Dalla riforma Gelmini, dal 2010 al 2017, le università hanno assunto solo 2.295 persone come RTD-b - come ho già detto - a fronte di 14.492 pensionamenti: 12.000 posti evaporati nelle nostre università. Si può parlare a tutto titolo, senza timore di essere smentiti, di un vero e proprio attacco E non finisce qui, signora Presidente.Il

poi il capitolo dell'abilitazione scientifica nazionale, signora Presidente: 12.600 abilitati a professore ordinario, 24.500 abilitati a professore associato, per un totale di 36.000.

per gli enti pubblici di ricerca, con l'obbligo degli stessi enti di ricavarne un altro 50 per cento in più, e quindi fino all'ipotetica cifra di 75 milioni. Ebbene, a quanti ricercatori corrispondono 75 milioni? Se andiamo a vedere la relazione tecnica dell'articolo 56, in cui si sono stanziati 13,5 milioni per 300 ricercatori negli enti pubblici di ricerca, facendo la divisione il risultato è pari a 45.000 euro per ricercatore. E, in effetti, questo è un costo giusto, perché le tabelle ci dicono che 47.000 euro è il costo di un ricercatore di terzo livello negli enti pubblici di ricerca.

è totalmente insufficiente per venire incontro alle esigenze della massa di precari, con i numeri che ho denunciato proprio in questo mio intervento. Naturalmente apprezzo il fatto che nell'emendamento si faccia menzione specifica dell'articolo 20 del decreto legislativo

Per il resto si tratta ancora una volta di un provvedimento tampone del tutto insufficiente a dare le giuste risposte a persone - parliamo di persone, e lo sottolineo ancora una volta che hanno dedicato la loro vita al Paese, per intraprendere una carriera, nelle università e nella ricerca, a fronte della continua incertezza che stanno vivendo e patendo sulla loro pelle. Abbiamo visto le mobilitazioni che si sono susseguite in questi giorni e l'occupazione del CNR

Hanno patito più di ogni altra categoria le disposizioni, le mannaie cadute nel 2010 per fare cassa sul pubblico impiego; non stati recuperati gli scatti e ancora una volta l'articolo 55, in maniera del tutto insufficiente, prevede il ritorno alle biennalità a partire dal 2020. totalmente insufficiente, tant'è vero che c'è ancora una volta un emendamento sia della maggioranza che delle opposizioni. Ebbene, qual è la soluzione di cui stiamo discutendo? Un *una tantum* nel solo anno 2018, peraltro, facendo i calcoli, pari a circa un terzo di quello che hanno perso con il blocco perdurante dei loro scatti stipendiali. È un blocco valevole - lo ricordo - anche agli effetti giuridici, e non solo economici: è come se non avessero lavorato per cinque anni,

Grazie dei Governi che si sono succeduti in questa legislatura, quello Renzi prima e Gentiloni Silveri poi, a dare qualsivoglia risposta in termini strategici e strutturali al settore dell'università e della ricerca. Io penso che questo sarà un prezzo che voi pagherete alle prossime elezioni, perché non si può mortificare per tanti

pregnante: questa legge di bilancio, per quanto riguarda la cultura, mi è sembrata più un film sugli indiani che attaccano la diligenza piuttosto che quello di un Ministro che ha una visione organica su ciò che dovrebbe essere il finanziamento alla cultura e sulle misure che ancora devono essere prese nel campo dei beni e delle attività culturali.

Il sistema di non avere una visione organica del finanziamento degli istituiti e degli enti di cultura nel nostro Paese e di continuare ad alimentare un sistema che fa sì che il tale istituto di cultura o il tale ente si debbano affidare alla generosità del parlamentare, non fa altro che alimentare quel circolo vizioso, per cui quegli enti non sono "liberi", ma continuano a essere dipendenti magari dalla bontà e generosità del parlamentare che si prende a cuore la loro causa. Voglio essere buona e non voglio parlare di prebende o marchette.

però, c'è di tutto, a partire dal finanziamento per la ristrutturazione di chiese a seguito di eventi alluvionali. Per l'amor di Dio, un evento alluvionale è importante e può portare anche alla degradazione di una struttura. Mi chiedo,

che impegnava il Governo a trovare i fondi per acquistare la parte ancora in mano ai privati, che si sta degradando e sta intaccando la parte di proprietà della Curia, che si sorregge sulla buona volontà di don Carlo, un prete meraviglioso che sta tenendo in piedi un gioiello del nostro patrimonio medievale. Troviamo i soldi per la chiesa di Aulla, mentre il Governo si dimentica di trovare un milione di euro per mantenere

apre la via a degli istituti culturali dipendenti dalla volontà politica. Queste fondazioni, infatti, percepiscono finanziamenti pubblici e non si possono reggere su finanziamenti privati e, quindi - gioco forza - diventano dipendenti dalla bontà del politico di turno, con tutto quello

per le biblioteche, dimenticandoci in quali condizioni versano le nostre periferie e di quanto le biblioteche servano per contrastare il fenomeno delle sale videolottery, con tutto il bagaglio di degrado sociale che si portano dietro. *(Applausi

si è sbloccato finalmente il bando per i 500 funzionari, ma i restauratori sono ancora fermi alla partenza, e forse alla partenza dell'ippodromo di Merano, quello a cui abbiamo dato i soldi facendo un favore a Zeller. Non c'è niente, invece, sul piano delle assunzioni per il personale e sappiamo quanto sia necessario provvedere a nuove assunzioni. Avete respinto un mio emendamento sulla digitalizzazione e catalogazione e a tale proposito si è aperto un giallo sui fondi. L'emendamento è stato respinto dicendo che i fondi c'erano già, mentre dal MIBACT mi dicono che non ne

Pompei, con un emendamento avverto il Ministro che si è dimenticato, nella proroga che propone, di prorogare gli organici che sono dentro la struttura della segreteria generale del progetto. Se si proroga il progetto, ma non gli incarichi a chi ci lavora all'interno, si crea un problema a marzo 2018.

è stato bocciato perché non segnalato tra i subemendamenti, cosa che non era stata chiesta. Se la vedranno Franceschini e Morando e magari parleranno anche dei famosi soldi per la catalogazione e la digitalizzazione, che non si capisce se vi siano o meno. Ma voi

Dopo i beni culturali, passiamo alla scuola. Sull'alternanza scuola-lavoro abbiamo definitivamente decretato che non è un momento di formazione e di affiancamento, ma è un momento in cui proprio si va a lavorare. *(Applausi stipendi dei docenti della scuola pubblica sono fuori dai *radar*, come sempre, e continuano a essere i peggiori pagati in Europa. Noi avevamo avanzato molte proposte per quanto riguarda il diritto allo studio, proposte che non sono state accolte. L'emendamento Verducci stanzia delle risorse per il diritto allo studio. Anche noi avevamo una proposta per stanziare più risorse, ma ci compiacciamo che almeno sia stato accolto l'emendamento Verducci, il quale però avrebbe dovuto avere un po' più di coraggio.

Ma sì? Ma dove? Nessuno ha aderito al bando e adesso possiamo utilizzare quei fondi per coprire altro. Concludo velocemente. C'è la proroga dei servizi di pulizia e manutenzione nelle scuole, sempre con le esternalizzazioni, che sappiamo non dare un maggiore risparmio e a cui maggiore risparmio e a cui sono legate anche vicende giudiziarie per quanto riguarda i bandi di assegnazione. Continuiamo quindi. E non avete voluto accogliere una nostra proposta. Le maestre delle scuole dell'infanzia, dimenticate dalla buona scuola, poi illuse e sacrificate da un provvedimento del 2016, oggi sono di nuovo dimenticate e speriamo che torni la memoria alla Camera. L'AFAM: benissimo la statizzazione, abbiamo votato favorevolmente, ma la stabilizzazione dei docenti, anche quella, resta *missing* e continua a navigare in un limbo di anni e anni. Sul riordino del comparto siamo rimasti fermi alle *slide* e al bel nome

ci dispiace che l'emendamento Verducci, che metteva un correttivo agli scatti stipendiali per i docenti, sia stato ritirato, pare, pare, per problemi di copertura e speriamo che si possa approvare alla Camera. Infatti anche su questo veglieremo, perché siamo in clima natalizio e quindi veglieremo come il bue e l'asinello su tutte queste cose. siamo contenti che ci sia stato questo timido passo in avanti per la stabilizzazione dei ricercatori negli enti pubblici di ricerca. Bisognava avere un po' più di coraggio (sappiamo infatti che in realtà l'obiettivo era molto più ambizioso) perché c'è un intero comparto che da anni aspetta questo passo, sul quale si regge il nostro futuro.

Noi dobbiamo decidere se vogliamo essere un Paese fanalino di coda, destinato a diventare un bacino di approvvigionamento di manodopera a basso costo, o se intendiamo investire risorse adeguate nella ricerca e lanciarci nel futuro tra i Paesi che traineranno le comunità internazionali verso il futuro con idee e proposte innovative, per cercare di superare le sfide complesse che questo presente impone a tutti noi.

infatti dare uno sguardo complessivo alla manovra; una manovra iniziata con l'impostazione del DEF, passata attraverso il collegato fiscale e che adesso arriva al disegno di legge di bilancio, che la maggioranza sviluppa tra il Senato e la Camera.

non applicare meccanicamente l'elevazione dell'età pensionabile, come è previsto dalla normativa vigente, e, insieme con le forze sociali e con il sindacato, riaprendo un dialogo con essi, di individuare 13 categorie per le quali questo meccanismo non è automatico. Quindi facciamo una scelta importante sul piano dell'equità. Allo stesso modo è una scelta sul piano dell'equità, soprattutto verso il futuro, quella di continuare a sostenere

e neanche l'immigrazione sta riuscendo a colmare questo dato. Certo, non è quella l'unica soluzione, ma, siccome sappiamo - perché questo ci dicono i dati - che, purtroppo, all'aumentare dei figli aumenta il rischio di povertà, soprattutto nelle classi medie, anche l'intervento economico va preservato. Dico di più: questo aspetto rafforzato nei prossimi anni; andrebbe stimolato e garantito, anche per la fatica che questo Paese ha di guardare al futuro. Così come sta sullo stesso filo strategico, secondo me,

tra chi dà e non poteva ricevere niente fino a questo momento. Pensiamo anche alle scelte che abbiamo fatto verso i cittadini nel decreto fiscale; allo *stop* alle bollette ogni ventotto giorni, per dirne una:

restituire a chi ha pagato di più la crisi qualcosa del di più che quest'anno, l'anno scorso, sta iniziando a emergere. Non siamo ancora usciti dal *tunnel* ma, in fondo, il lavoro fatto inizia a dare risultati sui quali si possono costruire fondamenta solide per un'uscita di questo Paese dalla crisi e una ripresa del ruolo e del compito che il nostro Paese ha in Europa.

ha disciplinato le procedure per accedere alle prestazioni di mobilità in deroga erogate dall'INPS. Il Ministero del lavoro, il 4 novembre 2016, ha emanato la circolare n. 34, con la quale sono stati attribuiti alla Regione Molise 52 milioni di euro per il pagamento della mobilità in deroga per il triennio 2014, 2015, 2016 a una platea di circa 2.000 lavoratori. Nel frattempo, la Regione Molise, in data 23 dicembre 2016, ha pubblicato nuove istruzioni operative sulla mobilità in deroga, ampliando questa platea ad altri lavoratori ed estromettendo di fatto i circa 2.000 lavoratori che non hanno potuto fare domanda per l'anno 2016. In pratica, la Giunta regionale del Molise, con delibera n. 638 del 30 dicembre 2016, ha pensato bene di utilizzare i fondi già destinati a finanziare le politiche attive del lavoro per l'area di crisi Chiedo pertanto al Governo di provvedere al pagamento delle spettanze relative agli anni 2015 e 2016 ai lavoratori che ne avevano diritto, e di stanziare le risorse necessarie per il sostegno alla nuova platea di lavoratori.

si è creata nei Comuni di Bardonecchia e Oulx, in alta Val di Susa. Sono ormai decine i migranti che arrivano in queste due località per cercare una strada verso la Francia. La strada possibile per andare via dall'Italia passa attraverso due colli, il colle del Monginevro in particolare, che ormai è già pieno di neve e, purtroppo, in molti casi, c'è il tentativo di queste persone, di questi disperati, di attraversare il confine Italia-Francia passando nel *tunnel* ferroviario del Frejus, molto pericoloso, realizzato nel 1870, in questo *tunnel* laddove dovessero incrociarsi due treni e ci fosse una persona a piedi,

nella giornata di ieri RFI ha chiuso le sale d'attesa delle due stazioni di Bardonecchia e Oulx che erano di notte occupate da questi migranti. Naturalmente c'è l'intervento della Croce Rossa, c'è un'azione

Minniti un intervento soprattutto di rafforzamento della presenza delle Forze dell'ordine, perché scaricare su RFI la responsabilità dell'accoglienza, cosa che naturalmente

e si stanno diffondendo voci incontrollate secondo cui questi migranti sarebbero mandati dalla Francia verso l'Italia, cosa del tutto falsa, perché ci sono migranti che sono in Italia e che stanno andando in quei Comuni con l'aspettativa di andare in Francia. supportare la disponibilità che pure RFI ha dato di trovare altri locali riscaldati, che non siano le sale d'attesa delle stazioni, dove ospitare di notte queste persone, ma è necessario che la vigilanza e la sicurezza siano in capo alle Forze dell'ordine. Il prefetto di Torino ha convocato un comitato per l'ordine e la sicurezza lunedì, ma è evidente come sia necessario rafforzare la presenza di Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza in un momento in cui sta per iniziare anche la stagione sciistica e si rischia una situazione di tensione del tutto inopportuna dal momento che siamo di fronte a persone che versano in una situazione davvero drammatica e molto spesso

rivolgendomi al Governo, ai Ministri, alle Commissioni. Nei miei interventi, ho cercato di portare a conoscenza quello che succede realmente al di là dei cancelli di quelle fabbriche,

agli spazi di democrazia sempre più ridotti (tanto che agli operai - lo voglio ricordare - viene negata anche la possibilità di scegliere da chi farsi rappresentare). Ora credo che ci sia un problema che dovrebbe interessare tutti (so che quando parlo di altri temi tutti si voltano dall'altra parte), che è il tema occupazionale. Nonostante sia stato concesso praticamente tutto da questo Governo a FCA (ma non solo a FCA),

Pomigliano, Mirafiori, Cassino, Brugliasco, Cento, Pratola Serra, tra cassa integrazione e mancate riconferme di giovani operai la situazione è a dir poco preoccupante. Questo silenzio, che continua a essere non innocente da parte del Governo su questo tema, è veramente poco dignitoso. Spero seriamente che qualcuno abbia un sussulto

La seduta è tolta